il 19 marzo di diciassette anni fa un vile agguato di matrice brigatista colpì uno straordinario servitore dello Stato: Marco Biagi. Un uomo mite, un uomo colto e un uomo per bene, che stava tornando a casa in bicicletta dopo aver speso un'altra giornata lavorativa per il suo Paese, perché in realtà è questo che Marco Biagi faceva incessantemente, da quando giovanissimo aveva terminato gli studi e intrapreso il percorso accademico e professionale. Fu ascoltato consigliere di vari Ministri, oltre che un prezioso consulente per gli enti locali e per le istituzioni europee. I suoi studi nell'ambito giuslavoristico furono sempre ispirati alla possibilità di favorire l'adozione di politiche attive in grado di conciliare sviluppo economico e sviluppo sociale, competitività e sicurezza, flessibilità e benessere. Nel suo ricordo continua una fruttuosa e qualificata attività di approfondimento scientifico, portata avanti dalle università di Modena e dalle associazioni e i centri di studi che si ispirano che si ispirano alla cultura riformista di Marco Biagi, con un impegno significativo nella formazione delle nuove generazioni di ricercatori sociali. Alla famiglia di Marco Biagi e a tutti i suoi studenti di ieri e di oggi vorrei rinnovare la nostra gratitudine, la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Vi invito ad un minuto di raccoglimento.

ha comunicato le dimissioni dal Senato a seguito dell'elezione a Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo. Trattandosi di dimissioni motivate da incompatibilità, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, l'Assemblea non può che prenderne atto. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è autorizzata a convocarsi per l'individuazione del senatore subentrante.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 La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha stabilito su richiesta di alcuni Gruppi che, nell'ambito delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, all'ordine del giorno della seduta odierna, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca altresì sul *memorandum* Grazie cui seguiranno fasi uniche per la discussione e per le dichiarazioni di voto, con possibilità di presentare risoluzioni distinte per entrambi i temi in discussione. Dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio la seduta proseguirà con le relazioni e l'avvio della discussione generale del documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernente l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'interno.

potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori Segretari fino alle ore 19. Successivamente sarà proclamato il risultato. Il pomeriggio di domani sarà dedicato al sindacato ispettivo. Restano confermate, per giovedì 21 marzo, le mozioni di sfiducia individuale nei riguardi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: per le votazioni saranno indette due chiame. Alle ore 15 si svolgerà il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'economia, delle politiche agricole e della salute.

Europa, vorrei dirle che l'Europa si chiede anche se l'Italia, con questo Governo, stia perdendo quei valori che l'hanno contraddistinta nella sua storia millenaria. oggi non può non dire nulla, per l'ennesima volta, su quanto sta accadendo sulla nave Ionio al largo delle coste di Lampedusa.

costrette a rimanere al largo con le persone imbarcate sulla nave non avendo indicazione su cosa fare. I porti non dipendono dal Ministro dell'interno, ministro Toninelli: lei è qui e come Ministro delle infrastrutture i porti dipendono da lei.

verranno perseguite, sarà la magistratura a farlo, non lo può fare il ministro Salvini, ma lei oggi non può consentire che delle persone ancora una volta vengano tenute in ostaggio per fare la faccia feroce a fronte, in realtà, di politiche sull'immigrazione che sono deficitarie per quello che riguarda i rimpatri. *(Applausi dal Gruppo PD).* Faccia scendere quelle persone dalla nave, signor Presidente, le faccia scendere per la dignità del nostro Paese.

Sì, ancora. Ho tutto il diritto di parlare in quest'Aula e di chiedere, visto che oggi abbiamo il Presidente del Consiglio, un'assunzione di responsabilità, finalmente, su questa vicenda. Per l'ennesima volta, ci troviamo di fronte a un conflitto, che viene in qualche modo ratificato, tra il salvare le persone, e quindi tra il primato Presidente, mi rivolgo a lei - della salvezza delle vite umane e le regole e controregole (potremmo discutere a lungo sulla

presidente Conte, che in questo momento è quella di far entrare la nave, che è territorio italiano. Poi, una volta per tutte, su questa storia della chiusura dei porti,

Grazie intervengo per capire cosa sta succedendo in Assemblea, perché non ho ben capito se abbiamo aperto un dibattito sulla politica italiana in tema di immigrazione, di ONG, di contrasto all'immigrazione clandestina. In questo caso, chiediamo di rivedere i tempi di discussione e allungare il tempo a disposizione dei Gruppi, perché avremmo molte cose da dire su questo e sulla vicenda della nave Mare Jonio, su chi la capitana, sui personaggi dei centri sociali resisi protagonisti, in un passato non troppo lontano, di episodi di violenza gratuita ai danni degli avversari politici. *(Applausi dai

molto volentieri, però vogliamo avere il tempo sufficiente per farlo, per argomentare, per parlare di blocco navale e di mille altre cose. Altrimenti chiedo che la discussione si limiti a quanto previsto dalla Conferenza dei Capigruppo: Consiglio europeo, politiche commerciali con i cinesi e accordo Via della Seta.

seguiranno fasi uniche per la discussione e per le dichiarazioni di voto. I tempi del dibattito sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive due ore. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte.

A questo riguardo, vorrei dire che si è parlato di assunzione di responsabilità. Chi vi parla, a nome del Governo, si è sempre assunto dall'inizio la responsabilità che compete al Governo e continuerà a farlo.

perché su questa vicenda - come ho già detto - c'è una chiara linea politica in tema di migrazione che questo Governo sottoscrive e il responsabile dell'Esecutivo sottoscrive per primo. di una politica che può piacere, può essere opinabile. Diversi indirizzi politici sono stati espressi in passato e non tocca a me, oggi, valutarne gli esiti. Da parte nostra, noi li Da parte nostra, noi li abbiamo giudicati insoddisfacenti, partendo da un presupposto concettuale e pratico fattivo: il concetto di accoglienza è diverso da quello di sbarco. Consentire sbarchi indiscriminati senza limiti non equivale a offrire accoglienza.

senza nulla togliere a chi l'ha pensata diversamente e ha fatto valutazioni diverse. Abbiamo ritenuto che occorresse un diverso approccio per quello che a me piace chiamare non il fenomeno della migrazione, ma il problema politico, giuridico, economico e sociale della regolazione e della gestione dei flussi migratori. Il presupposto è che questo problema complessivo vada affrontato con un approccio strutturale e in modo da non rimanere schiacciati dal caso emergenziale.

Per rassicurarvi - perché comprendo le premure e sono stati evocati anche interessi fondamentali della persona - vorrei ricordare che, in tutti i casi emergenziali (anche quelli più drammatici, che hanno avuto gli onori delle cronache nei *mass media* per vari giorni), noi abbiamo sempre tutelato i diritti fondamentali delle persone e siamo sempre tempestivamente intervenuti per assicurare assistenza sanitaria ai bisognosi. Anzi, visto che si sta parlando di questo caso emergenziale, vi preciso che è stato prestato un soccorso sanitario (che si è poi rivelato superfluo, perché non sono state accertate patologie) anche a uno dei migranti della nave Mare Jonio. così continueremo a fare anche perché - attenzione - riteniamo che disincentivare gli sbarchi non solo contrasta più efficacemente il traffico di esseri umani (che è una cosa indegna per qualsiasi Paese civile), ma - ovviamente - evita anche il pericolo.

sul prossimo Consiglio europeo, che è il quarto a cui prenderò parte da quando ho l'onore di presiedere il Governo italiano e il quinto se consideriamo anche il Consiglio straordinario che si è tenuto lo scorso 25 novembre, nel corso del quale abbiamo approvato l'accordo di recesso con il Regno Unito e la dichiarazione politica. Questo quarto Consiglio europeo assume una valenza politica peculiare perché si svolge due mesi prima delle elezioni per il nuovo Parlamento europeo e deve al contempo confrontarsi con sfide cruciali per l'Europa di oggi e domani. C'è un *trait d'union* tra i principali temi in agenda al Consiglio europeo. Mi riferisco alla capacità dell'Unione europea di affrontare unita, da *leader* globale, temi che sono in agenda: l'epilogo della Brexit, il rapporto dell'Unione europea con la Cina, la priorità della crescita, del lavoro, dello sviluppo industriale e dell'innovazione, a fronte del rallentamento internazionale dell'economia e, infine, il cambiamento climatico. Se non saprà rimanere unita, l'Unione europea non potrà essere né forte, né competitiva, prima di tutto sul piano politico, nel definire e perseguire la propria posizione in ordine alle priorità appena menzionate, menzionate, rispetto alle quali è evidente che nessuno Stato nazionale, muovendosi isolatamente, potrà mai assicurare e garantire una compiuta ed efficace tutela dei propri interessi nazionali. In questo senso l'Italia si riconosce pienamente in un approccio europeo, come l'unico foriero di un futuro migliore per i nostri cittadini e per i cittadini dell'intero continente. L'esigenza di un'Europa unita al suo interno e forte nel mondo va tenuta a maggior ragione presente nell'attuale fase di fine legislatura europea. In vista dell'avvicendamento del Parlamento europeo e della Commissione europea viene ancora più in rilievo - se mi permettete - il ruolo del Consiglio europeo e quindi dei Governi. Occorre dunque che questo organo primario dell'Unione abbia discussioni prenda decisioni con vero spirito europeo, capace di mantenere coesa l'Unione, che adesso si è dilatata - siamo arrivati a 28 Stati membri - e che necessita, ora più che mai, di unità di intenti e di spirito solidale al suo interno. Per essere forte nel mondo - tornerò su questo punto quando ragionerò di rapporti con la Cina e con il Regno Unito - l'Europa deve essere un attore di respiro globale già al suo interno, elaborando adeguate strategie in materia di crescita, lavoro, sviluppo industriale e innovazione. Vedo purtroppo confermarsi - questo mi preoccupa molto - un approccio europeo prociclico e procedurale, che negli ultimi si è mostrato evidentemente inadeguato rispetto alla sfida della crescita e all'esigenza di equilibrio tra la riduzione e la condivisione dei rischi. Il rallentamento economico globale sta avendo un impatto sulla congiuntura economica in Europa e necessita di una risposta europea, con un rafforzamento della domanda interna e con un impulso alla crescita attraverso maggiori investimenti più coraggiose riforme. In particolare, l'esigenza di un rilancio della domanda interna è supportata da nuove evidenze empiriche, autorevolmente prodotte e argomentate, che in questo rilancio individuano la giusta risposta alla necessità che la crescita economica europea non sia eccessivamente dipendente dalla domanda esterna, vale a dire dall'e*xport*, e al rischio di una possibile tendenza strutturale dell'economia mondiale alla stagnazione. In questa prospettiva, soprattutto gli Stati membri che hanno spazio fiscale o *surplus* commerciali dovrebbero usarli a sostegno della domanda degli investimenti pubblici, in modo da permettere all'Europa di crescere a pieno potenziale e di reagire alle tensioni provocate dagli altri, rafforzando e rendendo più resiliente la propria economia. La continua sollecitazione alla crescita e alla competitività è da accogliere se è finalizzata ad accrescere gli *standard* di vita dei cittadini europei, ma è da respingere se nasconde un mero spirito mercantilista: lo vietano le regole europee, che non possono essere invocate solo quando ritenute convenienti. Per essere più espliciti, crediamo che la crescita della produttività del lavoro

piuttosto che favorire l'accumulo dei *surplus* commerciali, che peraltro, oltre una certa misura, sono vietati dalle stesse regole europee. Questi aspetti devono essere al centro della discussione di un Consiglio europeo che guardi alla realtà di un continente che soffre tuttora di troppe asimmetrie sul lavoro (lo dico soprattutto con riguardo ai giovani) e sulla crescita e deve ancora completare quel pilastro sociale adottato a novembre 2017 al vertice informale di Göteborg. È in chiave di impulso europeo alla crescita, al lavoro, alla sicurezza sociale che auspico sia orientata la discussione che il Consiglio europeo avrà sul mercato, rispetto al quale occorre promuovere la rimozione delle barriere ingiustificate, in particolare nel settore dei servizi, con sollecitazioni per la Commissione a prospettare e realizzare una visione di lungo periodo per il futuro industriale dell'Europa; maggiori investimenti nella ricerca e nell'innovazione; una più equa competizione al suo interno e a livello globale, con una politica commerciale ambiziosa e che protegga l'Unione europea contro le pratiche scorrette. L'Unione europea, anche nella prospettiva della nuova legislatura dopo le elezioni per il Parlamento europeo, deve lavorare a una vera strategia industriale europea, capace di creare crescita e occupazione attraverso il sostegno, con adeguate risorse, alle nuove tecnologie, alla ricerca e all'innovazione e capace di tutelare imprese e mercati europei da strategie aggressive di Paesi terzi. Questi impegni e l'obiettivo primario di sostenere crescita, lavoro e inclusione sociale sono al centro dell'azione del Governo italiano, ma la sfida di un'economia che cresca e crei posti di lavoro richiede uno sforzo europeo, come dimostra la recente polemica in materia di tecnologia delle comunicazioni. Dovremmo domandarci come mai uno spazio economico affollato da mezzo miliardo di persone, con livelli di istruzione tra i più elevati, con *standard* di vita tra i più alti al mondo, non sia stato capace di sviluppare sul tema delle telecomunicazioni un'infrastruttura alla frontiera della tecnologia, capace di soddisfare a pieno tutte le proprie e nuove esigenze. Non credo francamente che sia dipeso da carenze di intelligenze o di risorse destinate alla ricerca; credo piuttosto che questa inefficienza riveli un'altra manifestazione della mancanza di visione di lungo periodo dell'Europa a cui l'Italia può porre rimedio rilanciando l'idea di un'Europa protagonista nel mondo. Si tratta di un percorso in cui l'Italia, Paese fondatore e potenza industriale europea e globale, intende fare la sua parte e adoperarsi affinché la politica industriale, anche nel sostegno alle piccole e medie imprese e nella regolazione degli aiuti di Stato alle imprese europee, sia accompagnata da un approccio equilibrato e da politiche di convergenza, senza le quali solo alcuni Stati membri potranno sostenere i costi della citata politica industriale. Quanto alla politica commerciale, è fondamentale preservare la coesione dell'Unione europea nei confronti degli altri attori globali, dagli Stati Uniti (con cui l'Unione deve proseguire il dialogo e l'agenda commerciale positiva che è stata definita tra il presidente Juncker e il presidente Trump lo scorso 25 luglio) alla Cina, su cui ovviamente mi soffermerò tra breve. Prima di farlo, considero doveroso richiamare il sostegno italiano a un approccio ambizioso dell'Unione europea ai cambiamenti climatici, che considero componente essenziale di un'economia europea moderna e che saranno oggetto di un breve paragrafo delle conclusioni del Consiglio europeo, volto a consolidare un linguaggio unitario rispetto a un'intensa agenda del Consiglio ambiente dell'Unione. Alla sfida dei cambiamenti climatici l'Unione europea deve dedicare il meglio della sua capacità di adattamento ai mutamenti globali. Anche in questo caso gli sforzi nazionali da soli non bastano per garantire un futuro migliore. Il tema della sostenibilità è centrale anche ai fini della crescita del continente. Il potenziale di crescita dell'Europa - e questo spesso viene trascurato potrebbe tornare ai livelli sperimentati nel passato, se solo decidessimo di accelerare la transizione verso un'Europa decarbonizzata. Un grande piano di investimenti pubblici, finalizzati a questo scopo, darebbe un grande impulso anche a quelli privati, garantendo una robusta crescita ecocompatibile all'intero continente. Questa visione è coerente con il recente richiamo autorevolmente effettuato dal presidente Mattarella il 12 marzo scorso a Belluno, in occasione della cerimonia commemorativa dell'alluvione che ha afflitto la Regione Veneto lo scorso ottobre. La sessione economica del Consiglio europeo non avrà, a differenza del Consiglio europeo di dicembre scorso, un corrispettivo in forma di Eurosummit; rimane non di meno oggetto della nostra attenzione il percorso verso l'Eurosummit di giugno che, con una legittimazione in parte attenuata, a seguito delle elezioni per il Parlamento europeo di fine maggio, dovrà attuare, preparate dall'Eurogruppo, le decisioni dell'Eurosummit dello scorso dicembre. Sono in gioco, tuttavia - e conviene su questo soffermarsi un attimo - argomenti di fondamentale importanza per il futuro assetto economico e finanziario dell'Unione europea. Mi limito a richiamare, tra gli altri, i temi del *budget* dell'Eurozona, dello schema europeo di garanzia dei depositi (il cosiddetto EDIS) e degli emendamenti al Trattato sul meccanismo europeo di stabilità. In particolare, è attualmente aperta in seno all'Eurogruppo la discussione sulla definizione di uno strumento di bilancio per la competitività e la convergenza, appunto il *budget* dell'Eurozona, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. La questione è molto delicata per i nostri interessi nazionali: come sempre, ogni nuovo strumento può tornare utile ed efficace per rafforzare il nostro sistema economico-finanziario, ma, al contrario, può rivelarsi anche molto insidioso, a seconda di come venga concepito e concretamente strutturato. Per l'Italia - lo voglio chiarire subito - è prioritario che tale strumento sia di dimensioni adeguate, prevedendo anche una sua capacità di prendere a prestito sui mercati finanziari, offra un vero supporto a investimenti e riforme, che abbia funzioni anticicliche e di stabilizzazione e, soprattutto, non sia sottoposto a condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti. La discussione sulle relazioni esterne, prevista alla cena di lavoro del Consiglio europeo di giovedì 21, riguarderà i rapporti tra l'Unione europea e la Cina, in vista del vertice Unione europea-Cina, previsto che potrebbe seguire di pochi giorni - e l'argomento, comprendete bene, non è da trascurare - la conclusione del negoziato economico-commerciale in corso tra Washington e Pechino. Il vertice Unione europea-Cina a Bruxelles avverrà, inoltre, a poco più di due settimane dalla conclusione della visita di Stato del presidente Xi Jinping in Italia. Agli omologhi europei, giovedì, potrò quindi ribadire la piena coincidenza tra la visione italiana del rapporto con la Cina e la strategia seguita dall'Unione europea, che sarà persino rafforzata dall'approccio italiano. Confido che il 9 aprile il nostro *memorandum* con Pechino sull'iniziativa Belt and Road - una delle tante intese che verranno firmate, voglio precisare - non desterà più grande attenzione.

Ho avuto già modo di evidenziare e dichiarare pubblicamente: non è un accordo internazionale. Non crea vincoli giuridici. Se proprio volessimo definirlo da un punto di vista tecnico, potremmo, più correttamente, ragionare di una mera intesa programmatica che, ribadisco, pur non dando luogo a impegni giuridicamente vincolanti, delinea obiettivi, principi, modalità di collaborazione nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road, che è un grande progetto di connettività euroasiatica e che, sin dal suo lancio, nel 2013 (quindi, non ieri e neppure l'altro ieri), ha attirato l'interesse dell'Italia e dei suoi Governi. La nostra attenzione economico-commerciale nei confronti di queste infrastrutture e della Cina stessa è pienamente legittima ed è giustificata proprio alla luce dei nostri interessi nazionali. Per questa via - attenzione - potremo potenziare il nostro *export* verso un mercato di enormi dimensioni. Le nostre imprese avranno la *chance* di poter direttamente partecipare alla realizzazione di nuovi e importanti investimenti infrastrutturali. La nostra penisola, e segnatamente i nostri porti, i nostri scali commerciali, non saranno così bypassati dai nuovi traffici, ma potranno anch'essi godere a pieno titolo dei vantaggi economici e valorizzare la loro posizione geografica di terminali naturali di questa nuova Via della Seta. Attenzione: il perimetro del *memorandum* sulla Belt and Road è squisitamente economico-commerciale. non mette minimamente in discussione la nostra collocazione euroatlantica. Il suo contenuto, che è stato negoziato per lunghi mesi con Pechino, coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate, non presenta alcun rischio per i nostri interessi nazionali ed è pienamente in linea con la strategia dell'Unione europea, promuovendola, anzi, come nessun Paese membro ha fatto sinora nel suo dialogo con Pechino. Il *memorandum*, infatti, imposta con estrema chiarezza la collaborazione sulla Belt and Road, in raccordo con i principi espressamente richiamati dall'Agenda 2030, dall'Agenda 2020 di Cooperazione Unione europea-Cina e dalla strategia dell'Unione europea per la connettività euroasiatica, capisaldi dell'approccio dell'Unione europea verso la Cina. Esso promuove, inoltre, con forza, i principi, condivisi in ambito europeo, di mutuo vantaggio, reciprocità, trasparenza, sostenibilità, tutela della proprietà intellettuale e prevede la creazione di un vero *level playing field.* Posso rivendicare, quindi, a buon titolo, e a ragione, che il nostro approccio alla Belt and Road è tra i più lungimiranti ed efficaci che siano mai stati applicati in ambito europeo. Vorrei poi anche rimarcare, perché la questione non è trascurabile e, quindi, la offro anche al dibattito pubblico, che altri Stati membri, pur non avendo stipulato analoghe intese con Pechino, già collaborano, molto più di noi, su questa iniziativa. La verità è che l'Italia ha scelto un approccio trasparente, formalizzando la collaborazione con la Cina in una cornice ben definita, preferendo così esplicitare con chiarezza i pilastri fondamentali di matrice europea da cui ci lasciamo ispirare. Rispetto al *memorandum of understanding* firmato da altri Paesi, fuori e dentro l'Unione europea, il nostro stabilisce un raccordo molto più esplicito con le linee e le norme dell'Unione europea e promuove con più forza i valori e gli interessi dell'Italia. E, se mi permettete, questo è un gran vantaggio per l'Europa stessa. Su quest'ultimo aspetto vorrei precisare che l'attenzione del Governo non si è esaurita con il negoziato sul *memorandum*. Come nelle collaborazioni con altri Paesi, il Governo italiano opererà, nell'ambito della Belt and Road, un attento monitoraggio delle singole iniziative di collaborazione che saranno avviate a valle del *memorandum* per garantire che anch'esse siano promosse con attenzione alla difesa degli interessi nazionali, alla protezione delle infrastrutture strategiche, anche quelle nel campo digitale, e prevenendo il trasferimento di tecnologie in settori sensibili. Alla discussione al Consiglio europeo, al vertice Unione europea-Cina del 9 aprile, seguirà poi la mia partecipazione (ho già anticipato la mia adesione) alla seconda edizione del *forum* Belt and Road in programma a Pechino il 26 e il 27 aprile. Il Forum, che riunirà un numero elevato di Paesi, mi offrirà un'ulteriore occasione per promuovere, in uno spirito di collaborazione con Pechino, quella che deve essere la visione italiana ed europea sull'iniziativa Belt and Road. Alla discussione sui rapporti con la Cina, il Consiglio europeo arriverà dopo una sessione - quella di apertura, giovedì 21 pomeriggio - in cui, in formato 27 (senza il Regno Unito evidentemente), si discuteranno gli ultimi sviluppi relativi alla Brexit. Nonostante gli sforzi negoziali aggiuntivi sulla questione irlandese e l'intesa raggiunta da May e Juncker l'11 marzo scorso, la settimana scorsa - lo sapete - c'è stato un secondo voto negativo del Parlamento britannico sulla ratifica dell'accordo di recesso. Questa decisione è avvenuta a pochi giorni dalla data stabilita per l'uscita dall'Unione europea lo ricordo, è il 29 marzo 2019. Nonostante il poco tempo a disposizione, dobbiamo cogliere i messaggi positivi emersi dai voti successivi a quello sulla ratifica, con cui il Parlamento britannico ha espresso la volontà di evitare una Brexit senza accordo, e dobbiamo lavorare insieme ai *partner* europei per garantire un'uscita in termini chiari e amichevoli, chiedendo un differimento dei tempi di uscita dall'Unione europea. È molto probabile, quindi, che i 27 Capi di Stato e di Governo al Consiglio europeo saranno chiamati a discutere una possibilità di proroga della data di uscita. Come anticipato dallo stesso Governo britannico, non si tratterà, però, di una proroga in bianco ma, se del caso, di un differimento funzionale all'obiettivo di garantire un recesso ordinato. Come abbiamo sempre fatto durante questo faticoso - permettetemi di dirlo - negoziato, dalle dinamiche molto complesse, continueremo a lavorare per una Brexit ordinata, nel pieno rispetto della volontà del popolo britannico e delle decisioni del Parlamento di Londra, ma anche ribadendo la necessità di maggiore responsabilità e di maggiore chiarezza nell'interesse dei nostri cittadini e delle nostre imprese. L'auspicio è che le decisioni di questi giorni a Londra garantiscano un'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza strappi, in maniera ordinata, in modo da poter costruire una relazione futura tra Unione europea e Regno Unito che sia all'altezza dei profondi, speciali rapporti che abbiamo costruito con i britannici in oltre quattro decenni di comune partecipazione al processo di integrazione europea. In un contesto che mantiene ancora forti elementi di incertezza, il Governo italiano continuerà a lavorare per garantire la tutela dei diritti dei cittadini, delle nostre imprese e della stabilità finanziaria, anche nell'ipotesi, che davvero è poco auspicabile, di un'uscita senza accordo (il famoso *no deal*) per il 29 marzo 2019. Ai temi sinora citati, si aggiunge anche un breve paragrafo, nelle conclusioni, riservato ad uno stato dell'arte sulle azioni poste in essere a contrasto della disinformazione, con un invito alle piattaforme *on line* e ai *social network* ad assicurare elevati *standard* di responsabilità e di trasparenza. A giugno il Consiglio europeo riceverà un rapporto sulle elezioni apprese, che verrà predisposto dalla Presidenza con la Commissione e con l'alto rappresentante dell'Unione Per l'Italia, uno sforzo europeo coordinato su un fenomeno ormai percepito in molti Paesi europei come una minaccia alla democrazia è necessario, proprio in virtù della natura complessa e plurale del problema e delle relative insidie. La disinformazione, venendo da una molteplicità di soggetti statuali e non, richiede un approccio strategico multidimensionale e di ampio respiro, che accanto ad una rafforzata cooperazione internazionale preveda anche un investimento di lungo periodo nella formazione dei giovani e non trascuri, naturalmente, i delicati profili di necessaria garanzia della libertà d'informazione, fondamento essenziale delle nostre democrazie. È proprio la piena tutela della democrazia, anche sul piano del diritto al lavoro, alla sicurezza e al benessere, che rende necessari nei *leader* europei una visione strategica e un impulso a politiche europee di più ampio respiro. Con questo spirito, il Consiglio europeo potrà affrontare la transizione verso la fase successiva alle elezioni del Parlamento europeo, ponendosi in sintonia con una domanda di cambiamento che - attenzione - attraversa l'intero continente e merita risposte urgenti, che possano realizzare le premesse per un futuro migliore per i nostri cittadini. Vi sono davvero grato per l'attenzione.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio:

come unico foriero di un futuro migliore per i nostri cittadini e per quello dell'intero continente, signor Presidente, il Gruppo per le autonomie, che qui ho l'onore di rappresentare sicuramente sottoscrive in pieno tali dichiarazioni.

dice cose largamente condivisibili, ma la percezione che c'è in Europa e in generale dell'approccio europeo del nostro Governo è totalmente diversa. allora sono due: o lei - legittimamente, come persona ragionevole - si presta in qualche modo a fare una plastica facciale della politica vera del Governo o - seconda ipotesi - è in atto una revisione, che personalmente mi sentirei di auspicare, della politica europea del Governo.

Il posto dell'Italia è nella critica a questi Paesi o nella condivisione, nella complicità e nella collaborazione con questi Paesi per dare nuovo smalto a un'Europa che certamente ha problemi che non riesce a risolvere? Signor Presidente, noi riteniamo con molta sincerità e speriamo che ci sia una revisione critica della politica del Governo e che l'Italia riprenda il posto che ha sempre avuto. Lei ha Lei ha detto in gran parte cose condivisibili e, peraltro, noi non abbiamo gli elementi sulla Brexit non perché non ce li fornisca lei o non ce li abbiamo noi, ma perché non li forniscono gli inglesi, perché hanno una situazione molto difficile.

la collocazione atlantica dell'Italia - e lei ha fatto benissimo a spiegare che questa collocazione non è in discussione - questo avviene perché ci sono degli antefatti. Noi abbiamo avuto un Ministro della difesa che dal mattino alla sera, senza aver interpellato su questo il Ministro degli esteri che si era dichiarato del tutto ignaro, ha spiegato che l'Italia si ritirava dall'Afganistan; poi abbiamo una polemica altalenante sul tema degli F-35, che è non solo un insieme di commesse negoziate, ma anche un insieme di impegni presi a livello internazionale. Andiamo avanti: Andiamo avanti: sul Venezuela la comunità europea ha preso una posizione assieme agli Stati Uniti e noi, anche in questo caso, ci siamo distinti. ci sono delle motivazioni che stanno alla base di una diffidenza che sta crescendo nei confronti dell'Italia da parte della comunità internazionale. Lei stesso ha parlato della necessità di un'Europa più unita sotto il profilo dei commerci. Sappiamo che questa è la competenza specifica dell'Unione europea, ma noi auspichiamo che la concertazione la concertazione che il suo Governo porti al tavolo dei *partner* europei è di lavorare assieme sul tema della Via della Seta. Non servono fughe in avanti, anche se evidentemente il Governo, in queste ore, ha lavorato per limare i trattati e e lei ci può giustamente venire a dire che questo *memorandum* di intesa non ha impegni giuridicamente vincolanti. Sappiamo bene che gli altri Paesi europei hanno una penetrazione commerciale e rapporti con la Cina più forte di noi. noi. Siamo amici della Cina e crediamo che il Governo faccia benissimo a lavorare per accordi commerciali nella direzione corretta, ma vi chiediamo di essere parte di un disegno europeo perché le fughe in avanti - detto sinceramente - non siamo - non siamo neanche in grado di farle, perché gli altri, se vogliono, le fanno meglio di noi. Noi siamo il Paese d'Europa più interessato a un'Europa che decolli. Se le sue parole oggi in quest'Aula sono il segno che c'è una revisione rispetto alle scellerate polemiche di questo primo anno contro l'Europa a giorni alterni da parte dei Ministri del suo Governo, non non guardiamo al passato. Tra il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno tengo il bicchiere mezzo pieno perché sono un patriota e perché sono interessato a che l'Italia vada nella direzione giusta, indipendentemente da chi governa. I Governi passano, ma l'Italia rimane. Il punto vero è che mi auguro fortemente che la direzione si corregga finalmente e che con questa sua relazione si segni una discontinuità tra una prima parte del suo Governo e una seconda parte. Sappiamo che c'è la campagna elettorale, ci sono le elezioni europee, ci saranno mille polemiche: speriamo che non inquinino inquinino e non avvelenino più di tanto i pozzi della politica. Abbiamo bisogno di trovare una congiunzione di intenti e di destino comune con gli altri Paesi europei,

ci rendiamo conto di come non possiamo permetterci di procedere in ordine sparso, perché diventiamo irrilevanti tutti. Ma il nostro Governo deve recuperare quello spirito europeo che noi non abbiamo visto in questi mesi. mesi. Altre considerazioni le faranno i colleghi. Io voglio solo dirle che mi auguro che questo Consiglio europeo possa essere produttivo e foriero di risultati positivi. Voglio esprimere un auspicio anche rispetto al Regno Unito: noi abbiamo un destino comune con il Regno Unito; credo personalmente che sia stato un errore enorme il voto sulla Brexit, a dimostrazione che non ci sono vie di fuga solitarie, e questo lo dico a tutti i sovranisti. Noi dovremmo sì essere sovranisti, ma essere sovranisti europei. Per noi, il nostro vero sovranismo è tornare a identificarci in un destino comune con i nostri *partner* europei: questo è il sovranismo positivo che io voglio evocare. E mi auguro che il Regno Unito possa recuperare, con queste trattative in zona Cesarini, un senso di un destino comune che inevitabilmente ha con il resto d'Europa. Le auguro buon lavoro e speriamo che il vertice europeo possa essere positivo per tutti i cittadini del nostro continente.

I temi che verranno trattati nel prossimo Consiglio europeo sono la sintesi delle problematiche su cui i nostri *partner* europei discutono già da molto tempo. La questione del rilancio economico, la questione ambientale, la questione dei rapporti della UE in questo caso sono

È anzitutto fondamentale, signor Presidente, agire sul fronte del cambiamento economico. Come sappiamo, le regole imposte dall'Unione europea sui bilanci degli Stati hanno inibito l'espansione economica e, con le riforme del lavoro approvate negli ultimi anni, hanno anche aumentato precarietà e disoccupazione. Per questo è necessario compiere quello che lei, signor Presidente del Consiglio, ha definito uno sforzo di responsabilità collettiva, e affrontare la questione del lavoro e della disoccupazione giovanile perseguendo un'efficace tutela della dignità della persona, che protegga sia il salario dei cittadini, sia i disoccupati, prevedendo ad esempio un'assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l'introduzione di un salario minimo europeo. Il Governo del cambiamento ha già dimostrato che è una strada percorribile con l'introduzione del reddito di cittadinanza e le riforme collegate, come ad esempio quota 100. Sono misure che - lo ricordo - oltre a sostenere le fasce più deboli della popolazione, permettono anche di introdurre nuova liquidità nel mercato interno e di conseguenza aumentare l'occupazione. Ma occorre per questo superare il dogma del pareggio di bilancio, che stride con l'esigenza di rilanciare un ruolo pubblico dell'economia con investimenti e opere infrastrutturali. Per questo questo è il momento di uscire dal dilemma crescita-stabilità. Questo non esime l'Italia e i *partner* europei ad attuare riforme coraggiose anche dei meccanismi di funzionamento politico dell'Unione, a partire dalla centralità del Parlamento europeo, che oggi, come sappiamo, incide relativamente nei processi decisionali interni dell'Unione europea. Non basta. L'Unione europea deve avere una strategia industriale di sostegno alla ricerca e all'innovazione comune, seppur nel rispetto delle peculiarità delle singole realtà. Un esempio su tutti è la tecnologia 5G, sulla quale l'Unione europea non è in grado in questo momento di produrre una risposta sotto il profilo tecnico-economico.

Sul tema dei cambiamenti climatici è necessario infatti andare oltre i limiti evidenti del cosiddetto sviluppo sostenibile ed anche qui è necessaria una linea comune, che faccia dell'Unione europea un attore globale nella promozione della decarbonizzazione e delle fonti rinnovabili.

di stamattina alla Camera che in quello di oggi pomeriggio al Senato. Grazie Presidente, buon lavoro.

che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Nicola Calandrini. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Nicola Calandrini. Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

è un piacere crescente di volta in volta, perché lei acquisisce dimestichezza sempre maggiore, e soprattutto è un sollievo, dopo le picconate che i suoi Ministri danno a quella politica tra un Consiglio europeo e l'altro. Questo è penoso per lei e per il Paese, perché è uno schema che ormai conosciamo bene, secondo il quale suoi Ministri "rompono ma non pagano", anzi lucrano o pensano di lucrare in termini di consenso, mandando in frammenti una politica europea dell'Italia costruita nel tempo e i "cocci" non sono loro ma sono suoi, e nostri come cittadini italiani, perché malgrado i suoi sforzi - lo dico sinceramente - molto lodevoli, mai è stata così in basso e così incompresa la politica estera del nostro Paese, nostro Paese, in particolare in Europa. Mi trovavo a Berlino la scorsa settimana, invitato a un'audizione al Bundestag su un documento che avevo preparato per incarico delle tre istituzioni europee sul bilancio settennale dell'Unione e ho visto poi varie personalità che conoscevo da tempo e anche nuove, come la nuova Presidente della CDU, e inevitabilmente la conversazione andava anche sull'Italia, anche se io davo considerevoli colpi di freno, perché non era quello l'obiettivo della mia missione a Berlino. Ho però proprio constatato il loro totale sconcerto, che probabilmente quando si incontrano con lei, essendo, come lei, uomini e donne di mondo, riescono abbastanza a mascherare. C'è una situazione molto delicata, che mal si concilia con le presentazioni che lei ci fa e che, come ha detto il presidente Casini, sono coerenti - non diciamo convenzionali - ed in linea con l'europeismo dell'Italia. Vorrei concludere chiedendomi chiedendomi come potremmo noi aiutarla a trasformarsi in architetto progettista della politica estera europea dell'Italia da quel restauratore *ex post* della politica europea dell'Italia che è costretto ad essere oggi.

guardando agli ultimi sei-otto mesi - e siamo ancora prima dell'infuocarsi dei dibattiti per le elezioni europee - la politica estera dell'Italia e quella europea sono state teatro del trionfo dell'incompetenza. La linea è stata fissata da estemporanee uscite verbali - o digitali - di questo o quel membro del Governo, meglio se impreparato nel merito e incompetente nel ruolo. Lei e il Ministro degli esteri, in più occasioni, siete stati smentiti da questo o quel Vice Presidente del Consiglio, in altre occasioni avete abbozzato e rammendato, ma sono gli interessi e la considerazione dell'Italia ad andarci di mezzo. Ora che a mio giudizio - e credo a giudizio di molti - il Presidente del Consiglio appare rafforzato e apprezzato

«Il Presidente del Consiglio ricorda che ogni dichiarazione di membri del Governo, inclusi i Vice Presidenti del Consiglio, che non riguardi le materie di loro rispettiva competenza, non rappresenta la posizione del Governo italiano. Se tali dichiarazioni vengono rilasciate da esponenti di partiti, questi dovranno indicare che la dichiarazione viene rilasciata a tale titolo. Si invitano in particolare le sedi diplomatiche a non considerare le dichiarazioni di cui sopra come espressione di posizioni della Repubblica italiana». Di fronte a una tale innocenza cristallina voglio vedere chi potrebbe divergere da lei nel Governo che lei presiede. Questo è scolastico e velleitario, ma scusi, Presidente, perché noi italiani dovremmo accettare che il nostro Paese e la nostra bandiera vengano imbrattati e spesso coperti di ridicolo proprio da politici che ogni giorno richiamano noi ai valori ai valori della Nazione, della patria, della sovranità? Lei, a mio avviso, è sulla buona strada per mettere fine a questa fiera della incoerenza e del disprezzo degli italiani si invoca «prima gli italiani», ma prima gli italiani nel senso del ridicolo, spesso - per dare dignità, coerenza e di nuovo rispetto alla politica estera ed europea dell'Italia. Anche in questo lavoro, signor Presidente,

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in queste settimane si discute molto di clima e aumento delle temperature e dei risvolti negativi, ambientali e sociali del problema. Una relazione speciale dell'IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, ha mostrato come una delle conseguenze negative del riscaldamento globale sarà il calo della produzione di cibo nel mondo a fronte di un aumento della popolazione. Il documento riporta chiaramente dei possibili rischi legati proprio alla scarsità di cibo e alla possibilità che si verifichino conflitti dovuti a un aumento delle persone che soffrono la fame e la sete. Le aree più colpite saranno quelle dove già insistono ed esistono problemi di sicurezza alimentare. Da diverse analisi è emerso come il Mediterraneo sia un *hot spot* del cambiamento climatico, dove saranno più evidenti le variazioni di temperature e regime idrico. Per quanto riguarda l'agricoltura, i dati dimostrano che ci saranno problemi di approvvigionamento: per ogni grado di riscaldamento il raccolto dei cereali (riso, mais, grano) calerà dal 3 al 10 per cento. Ne deriverà una riduzione del quantitativo di mangimi per gli allevamenti con riduzione di carne, uova e latte. Ci sarà, inoltre, un incremento di malattie e parassiti e il pescato calerà del 10 per cento. Considerato ciò, il percorso verso un'agricoltura a misura d'uomo è la chiave necessaria per affacciarsi su un futuro nel quale la tutela di ambiente e salute e il rispetto dei diritti primari delle comunità devono tornare ad avere la priorità che spetta loro nella nostra scala di valori. È ormai inderogabile la scelta di soluzioni sostenibili, che riportino al primo posto i reali bisogni delle comunità e la tutela dell'ambiente, scalzando gli interessi di forme imprenditoriali sempre più aggressive. È dunque urgente tornare a pratiche agricole che non debbano essere sostenute dall'uso di pesticidi, privilegiando colture a destinazione alimentare, produzioni commisurate a reali fabbisogni delle comunità, fertilizzanti organici derivati da compostaggio aerobico, tecniche agronomiche che incrementino la fertilità dei suoli, incentivino la biodiversità e preservino la qualità delle acque e degli alimenti; soprattutto interventi che vadano verso la riduzione del consumo dei suoli destinati alla produzione di cibo, provvedimento al quale stiamo già lavorando a livello nazionale nelle Commissioni competenti. Ma ciò non basta: le scelte devono essere fatte a livello mondiale per rimanere al di sotto della soglia di 1,5 gradi centigradi di aumento della temperatura. Per questo bisogna intervenire in modo forte e deciso. I cambiamenti climatici attuali, infatti, per rapidità e caratterizzazione, sono solo ed esclusivamente collegati agli interventi antropici e questa posizione è stata riconosciuta dalle maggiori agenzie scientifiche internazionali. Gli Stati e le organizzazioni sovranazionali devono sanare, *in primis*, la grande frattura che esiste tra le risultanze scientifiche e il mondo politico e proprio dalla scienza farsi guidare per trovare dei rimedi ai gravi ed irreparabili danni che stiamo arrecando al pianeta e al genere umano. Chiediamo che anche in agricoltura si proceda nella direzione di arrivare alla modifica di tutte quelle pratiche che attualmente favoriscono, determinano e accelerano in modo irreversibile le variazioni climatiche. Bisogna procedere su questa strada, altrimenti si arriverà alla scomparsa del genere umano e alla fine del pianeta. In questo scenario l'Italia può e deve essere parte attiva di tutte queste politiche di protezione del clima e dell'ambiente. Il sistema europeo inizialmente vedeva come unica soluzione alla questione dei cambiamenti climatici quella di ridurre le emissioni di gas serra, di cui anche l'agricoltura è responsabile, in misura pari al 15 Negli ultimi anni ci siamo resi conto che a queste strategie di mitigazione si devono associare tutta una serie di strategie di adattamento. Bisogna fare in modo che l'agricoltura si possa adattare a queste variazioni climatiche. Ecco perché chiediamo espressamente che nei nuovi

Il primo ha a che fare con quello che ha detto prima il presidente Monti. Lei, presidente Conte, ha misurato, anche recentemente, nelle sedi europee la diffidenza nei confronti dell'Italia, a volte marcata anche da stereotipi. Non voglio alimentare un dibattito che rischia di essere esagerato, ma quella diffidenza va dissipata, perché attraverso l'Europa passano le sfide principali. Pertanto, il primo invito che vogliamo farle, presidente Conte, è quello di provare faticosamente a ricucire lo strappo che è avvenuto con alcuni Paesi storicamente alleati con noi nelle sfide principali. Se ci sarà un fuori sacco sul Venezuela o si parlerà di Russia, è importante mantenere il consenso europeo, essere compatti e dare l'idea che noi investiamo sulla dimensione comunitaria. È importante perché, se lo facciamo su quei *dossier,* è più facile affrontare anche il tema della gestione dei flussi migratori. Presidente Conte, l'ho ascoltata con grande attenzione quando ha detto

la Gran Bretagna decida di uscire senza un accordo. Stiamo parlando di 23 miliardi di *export*, più del doppio di quanto importiamo dalla Gran Bretagna. Rischiano di scattare le clausole MAC e non ce lo possiamo permettere. Vorremmo capire - so che ci state lavorando - quali sono i piani di emergenza in caso di *no deal*. Questo è un punto per noi fondamentale. L'altro punto riguarda un monito per i sovranisti e gli

negli ultimi anni, proprio grazie ai Governi Renzi e Gentiloni Silveri, si è costituito il *business forum* Italia-Cina e si è accorciato il *deficit* commerciale, portandolo sotto i 15 miliardi di euro. Quindi, bene le intese settoriali: aumentiamole e permettiamo al nostro sistema Paese di essere competitivo e presente con le piccole e medie imprese, perché quelle più grandi grandi ce la fanno anche da sole. Ma sa di cosa siamo preoccupati? Siamo preoccupati per un'adesione ad un progetto globale senza un'interlocuzione approfondita con i nostri *partner* storici all'interno dell'Alleanza atlantica e all'interno della dimensione perché questo non è solo un progetto economico-commerciale, ma è una visione alternativa nella geopolitica e nella costruzione di un nuovo ordine internazionale, in cui la Cina, legittimamente, aspira ad essere punto di riferimento dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi non allineati. Dunque, attenzione: possiamo stare dentro questo progetto, ma definire la cornice europea. C'è un vertice, il 9 aprile, tra Unione europea e Asia: definiamo la cornice europea, parliamo con i nostri *partner* storici dentro l'Alleanza atlantica e poi andiamo avanti su questo percorso. Lo dico perché Lo dico perché la Cina ha costruito in quella via marittima una serie di punti strategici che contrastano con il principale alleato che abbiamo dentro il Patto atlantico. Vediamo gli investimenti sugli Stretti principali,

con il riferimento principe del Patto euro-atlantico. Questo è allora un punto fondamentale: lo abbiamo discusso con i nostri *partner* storici? Questa è la domanda fondamentale e via via, con le dichiarazioni più ancora che con i fatti concreti, si dà la sensazione che con l'attuale Governo ci si stia allontanando dai riferimenti storici e cioè dall'atlantismo e dall'europeismo. Noi, dall'opposizione, non lo permetteremo.

ideologie, salutata da molti come l'apertura di spazi di libertà e di azione politica svincolati da schemi concettuali preordinati. In Europa la morte delle ideologie si è tradotta nel considerare ammissibile un'unica ideologia: l'europeismo. La morte delle ideologie sta diventando l'assassinio del pluralismo e l'arma di questo assassinio è la criminalizzazione della propaganda. Di quale propaganda? Ovviamente di quella degli altri, di chi non aderisce all'europeismo liturgico, di maniera, che qui spesso viene celebrato. Questa evidenza si impone alla lettura della JOIN(2018) 36, uno dei documenti in esame al quarto punto dell'ordine del giorno del Consiglio. Lo scopo dichiarato è apparentemente nobile: la lotta alla disinformazione. Chi vorrebbe più disinformazione, così come chi vorrebbe, ad esempio, più inquinamento? Nessuno, naturalmente. Il diavolo però è nei dettagli e mi permetto, Presidente, di attirare l'attenzione sua e dell'Assemblea su alcuni di essi, nonostante vi siano, in questo ordine del giorno, anche ben altre priorità.

ed è totalmente opaco sul reclutamento e la valutazione dei cosiddetti *fact checker* indipendenti, gli alacri funzionari del ministero della verità europeo. Andiamo al primo punto: perché mai si dovrebbero combattere contenuti legali? Nel mondo in cui io e lei siamo cresciuti, i comunisti facevano propaganda per il comunismo, i socialisti per il socialismo e i liberisti per il liberismo, a meno di errori. legittimamente trovare discutibile l'idea che i mercati sanino ogni male del mondo, ma non per questo vorrà considerarla disinformazione: la considererà o una sciocchezza o propaganda. Personalmente sono lieto di essere vissuto in un mondo in cui a nessuno era ancora venuto in mente di criminalizzare la propaganda, che è legittima in un contesto di dialettica politica. Criminalizzare la propaganda per assicurare elezioni democratiche è una contraddizione in termini, una delle tante cui ci ha abituato l'europeismo liturgico. Quanto al ruolo dei *media* tradizionali non si contano le informazioni fattualmente false propalate dai *media* tradizionali, cioè giornali e televisioni. Faccio tre esempi: il 13 marzo scorso Massimo Nava, giornalista in un prestigioso giornale, ci diceva che l'Italia è un percettore netto di fondi dell'Unione europea; è un falso, Il 27 gennaio 2015, durante «Ballarò» un altro giornalista, Massimo Giannini, diceva che il debito pubblico della Grecia era al 125 per cento, poi è salito al 300 per cento, ma con la cura della *Troika* è sceso al 175 per cento. Peccato che al 300 per cento non ci sia mai arrivato e che quella cura

La propaganda sui *media* tradizionali è più e non meno insidiosa di quella condotta sui *social* per due precisi motivi: intanto perché si ammanta di un'aura di posticcia credibilità (normalmente chi disinforma sui *media* tradizionali è iscritto a un albo o a qualcosa e poi perché è indirizzata a fasce di popolazione che sono intrinsecamente più fragili, come ad esempio gli anziani, proprio perché la distanza dal *web* non consente loro di accedere alle fonti primarie. dobbiamo chiederci chi sono i *fact checker.* Se il buongiorno si vede dal mattino c'è da rabbrividire. Basta pensare a chi c'è nel comitato di alto livello dell'Unione europea per la lotta alla disinformazione: Gianni Riotta e Federico Fubini, due giornalisti che hanno attivamente promosso una propaganda politica ostile a questa maggioranza, anche con delle cadute nella *fake news.* Basta pensare a quando Gianni Riotta negava che il secondo comma del primo articolo della Costituzione menzionasse la sovranità popolare, una *fake news* con l'aggravante dell'odio ideologico. La sollecito quindi, presidente Conte, ad analizzare il tema del contrasto alla disinformazione partendo dalla serena constatazione del fatto che questo compito, il contrasto, viene affidato a persone che hanno attivamente fatto propaganda contro il suo Governo e questo dovrebbe suscitare in lei e in tutto l'Esecutivo una qualche attenzione. Da cittadino italiano rifiuto con sdegno l'idea che il nostro Paese abbia bisogno di tutele esterne per vivere una democrazia compiuta. Lei che si è dichiarato nostro avvocato difensore saprà difendere non solo l'interesse, ma anche la dignità del popolo italiano da chi implicitamente lo assimila a una massa di decerebrati influenzabili da algoritmi sul *web (Applausi dai

Presidente, onorevoli colleghi, giungiamo a questo nuovo Consiglio europeo con il consueto *spread* tra dichiarazioni, fatti e risultati che contraddistingue ormai l'agire di questo Governo e dei suoi azionisti. L'Italia si presenta a questo appuntamento ancora una volta sotto veste di osservata speciale, tanto dal punto di vista economico che per le sue determinazioni sul piano internazionale che costruiscono una sorta di Torre di Babele che getta una luce inquietante sul Paese. Si dice che la diversità è un valore. È vero, ma quando essa diventa confusione, quando essa assume contorni dell'incoerenza, dell'avventura e dell'improvvisazione, tanto più in un campo delicato quale quello della politica estera, un Paese perde di credibilità, mette a rischio le proprie alleanze, che sono di ordine culturale prima ancora che politico, e pregiudica il suo ruolo internazionale. Purtroppo è quello che sta avvenendo con una certa e preoccupante costanza. Non c'è una strategia, ma non si naviga neanche a vista. Continuate a parlare di un'Unione

Ci sono solo generiche dichiarazioni di cambiamento che equivalgono, come nella miglior letteratura, a non cambiare nulla. E di cambiamento, anche sul tema dell'immigrazione e del necessario approccio europeo, francamente si è visto ben poco. Eppure si ripete che tutto è cambiato. Il Consiglio affronterà, tra le tante questioni - dalla Brexit al tema dei cambiamenti climatici - il nodo dell'economia. Per noi non è proprio un capitolo delle gioie. Dovrà infatti approvare, o meno, le priorità politiche strategiche dell'analisi annuale sulla crescita che gli Stati membri dovranno inserire nei propri programmi. Mi chiedo, e chiedo al Governo, con quale forza e credibilità l'Italia siederà a quel tavolo e dirà la sua Ma soprattutto, visto che il Governo critica le ricette comunitarie in materia economica - aggiungo non senza ragione - avrà la coerenza di votare contro questo *dossier*, o magari di cambiarne i contenuti previsti? Temo che, come nei precedenti casi, seguirà la corrente, salvo poi dichiarare a favor di telecamera l'esatto opposto. Ma, così facendo, non si fa il bene dell'Italia, né dell'Europa, tantomeno si diventa attori credibili. L'unica cosa che realmente è cambiata in questo lasso di tempo, ma in peggio, sono le previsioni economiche, che annunciano per l'Italia tempi bui e questo grazie anche ad un Governo - il vostro - che ha varato una manovra tutta a debito, priva di investimenti e di sviluppo. Non è un caso che il country report dello scorso febbraio, base per la discussione in materia economica che affronterà il Consiglio europeo, annoveri l'Italia, insieme alla Grecia e a Cipro, tra i Paesi che presentano «squilibri macroeconomici eccessivi». Grazie a voi nel Consiglio si parlerà della nostra Italia come un Paese "untore", che rischia con le sue politiche economiche balorde di travolgere l'intera Unione europea, che pure sui temi della crescita non è esente da gravi responsabilità. Di tutte le raccomandazioni al vaglio del vertice, il Governo italiano nella sua azione non ne ha recepita nemmeno una: non fa niente sul debito, niente per sostenere la produttività e non fa niente per far fronte a quelle che nel *dossier* europeo vengono chiamate le «sfide specifiche». In questo contesto il tema del *memorandum* con la Cina rappresenta la ciliegina sulla torta. Abbiamo assistito - in questo caso sì - ad un cambio di rotta silente, ma epocale, per la nostra politica estera, un cambio che finirà per scontentare tanto i nostri alleati storici (Europa ed USA, cui non ci lega solo un rapporto economico-commerciale, ma anzitutto di civiltà e di valori), tanto i nuovi "compagni" di avventura. Anche con quale credibilità il Governo parlerà nel prossimo Consiglio europeo, che dovrebbe pronunciarsi a favore di ulteriori passi sul tema digitale, quando volete consegnare le nostre infrastrutture, anche quelle digitali, in mano ad una potenza straniera. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ma sapete che cos'è l'interesse nazionale? Non è un tema per dichiarazioni, ma è la libertà di un popolo e di un Paese. Francamente, non so se attribuire le vostre affermazioni sulla firma del *memorandum* a dolo o ad incompetenza: in entrambi i casi è grave e dimostra improvvisazione e inadeguatezza. Non aver ben chiaro l'orizzonte è preoccupante, poiché è un presupposto necessario per sedersi con consapevolezza al tavolo delle discussioni, avendo chiari obiettivi, rischi e strategie da adottare. adottare. Dunque, cari amici del Governo - e concludo - più serietà, più coerenza, meno dichiarazioni e meno avventure. Siamo alla vigilia di una fase economica e geopolitica delicata

come rappresentante dell'Italia è per questo Parlamento un valore aggiunto, che scaturisce evidentemente dalla sua personale credibilità, fermezza, nonché lungimiranza ed equilibrio, attitudini da lei dimostrate in diverse occasioni, come oggi. Queste doti le permetteranno, al Consiglio europeo, di manifestare, senza remore, il profondo convincimento di questa maggioranza dell'urgenza di un cambiamento di visione e di direzione politica, non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa. Dato che il dibattito verterà, tra gli altri temi, anche sul futuro del mercato unico e del mercato dei capitali, sono certa che ella riterrà utile ricordare che l'origine della parola «mercato» viene dal latino,

quel poco che valga, al Consiglio europeo dica che non tutto ha un prezzo, ma che molte sono le cose che, invece, hanno un valore. Dica, per esempio, che non è più in vendita la dignità dei lavoratori, né è più negoziabile lavoratori, né è più negoziabile il prezzo che il pianeta deve pagare a vantaggio del profitto di un'economia non lungimirante. Questo vale anche per la programmazione della politica digitale, per la quale sarà necessario prevedere misure urgenti per la tutela e la difesa dei diritti della nuova cittadinanza digitale, per permettere alle persone di restare tali anche nel mondo digitale e di non diventare, cosa che in parte stanno già diventando, dato prodotto da svendere. Che non si applichi più il paradigma, già applicato (e fallimentare, tra l'altro) nel passato, di una politica industriale rivolta a misure esclusivamente a favore del profitto. Non è retorica,

Siamo certi, presidente Conte, che ella saprà indicare la nuova strada, che l'Italia ha già cominciato a percorrere grazie a questo Governo, non perché sia la strada più facile da percorrere o che porta consenso, ma perché è la strada giusta e urgente, l'unica che possa, nonostante la volontà di crescita di cui abbiamo bisogno, ridimensionare i danni irreversibili che ha prodotto l'azione degli uomini che fino ad oggi hanno governato. Noi Noi siamo consapevoli che alcune azioni e alcuni provvedimenti non hanno portato consenso mediatico: come fermare le trivellazioni nel mare, come fermare come aver imposto l'ecotassa sulle auto, come la decisione di investire 11 miliardi di euro per prevenire disastri idrogeologici. Questi provvedimenti, però, che non hanno portato consenso, li abbiamo fatti lo stesso, e prima

il Movimento non è mai stato per una decrescita felice, ma per una crescita felice, equilibrata e in rapporto e in relazione ai diritti degli uomini e dell'ambiente. Una citazione, si sa, non si nega a nessuno e, quindi, abbiamo lasciato che dicessero «decrescita felice» più volte. A questo punto, mi prendo il tempo di una citazione anch'io, perché sono certa che lei porterà in Europa questa riflessione dentro di sé. Il re Mida,

Ahimè: anche il cibo, che lui voleva accostare alla bocca per mangiare, diventava oro. In questo momento in cui spesso si parla di tramonto dell'Occidente - molti intellettuali ne parlano facendo riferimento anche all'Europa - sono certa che lei, il 21 marzo (siamo praticamente in primavera), porterà una nuova primavera europea, voluta dall'Italia per un'Europa unita e più forte.

il Consiglio europeo rappresenta un'occasione per portare le istanze del nostro Paese in sede europea. Siamo stati abituati per troppi anni a vedere gli interessi italiani messi da parte dai nostri governanti in nome di un europeismo che altro non era che puro assoggettamento nei confronti di Bruxelles. Con questo Governo l'aria è cambiata: il rapporto con l'Europa è tornato ad essere un rapporto alla pari e la voce del nostro Paese non rimane inascoltata come succedeva in passato. Nel prossimo Consiglio si tratterà di temi fondamentali per il futuro dell'Unione: crescita dell'occupazione, la grande tematica relativa ai cambiamenti climatici e le relazioni esterne dell'Unione europea. Sul tema della crescita economica e dell'occupazione ribadiamo con forza l'impegno del Governo italiano nel superamento delle politiche di austerità europee, causa delle ricette economiche fallimentari adottate dai precedenti esecutivi. L'impegno dell'Italia in Europa deve perseguire il superamento del modello di promozione della competitività basato sulla deflazione salariale e puntare con decisione a politiche in grado di stimolare la domanda interna. Va prestata, inoltre, particolare attenzione ad una delle principali sfide che si apriranno nel breve termine: la sfida della digitalizzazione del mercato delle imprese, in grado di dare il via ad una vera e propria nuova era industriale, elemento essenziale che permetterà alle imprese italiane ed europee di stabilizzarsi come attori primari sul mercato internazionale. Sempre riguardo alla crescita economica e la tutela dell'occupazione italiana, va portato in Europa il tema della lotta alla contraffazione, un fenomeno che arreca decine di miliardi di danni al nostro sistema economico. La tutela del *made in Italy*, garanzia di qualità e di riconoscibilità per le nostre imprese operanti nel mercato europeo ed internazionale, deve rappresentare un obiettivo primario dell'impegno italiano in sede europea. Un secondo punto che verrà attenzionato dal Consiglio europeo è quello riguardante il clima: è importante ribadire la centralità dell'Accordo di Parigi che deve rappresentare la cornice all'interno della quale operare per il raggiungimento di obiettivi concreti, ben consapevoli della portata globale della lotta al cambiamento climatico. Bisogna agire promuovendo misure a sostegno di alternative tecnologiche innovative che permettano non solo un reale apporto alla tematica ambientalista ma che rappresentano anche uno strumento di rilancio economico e un'opportunità per le aziende italiane ed europee. Sulle relazioni esterne, il *focus* del Consiglio verterà sui rapporti dell'Unione europea con la Cina e sulla situazione Brexit. Entrambi gli argomenti sono certamente rilevanti ma non dobbiamo dimenticare, soprattutto in sede europea, l'importanza della situazione del Nord Africa, area geografica di importanza fondamentale per gli interessi italiani in merito a sicurezza, immigrazione e approvvigionamento energetico. È nostro dovere, presidente Conte, rimarcare l'importanza della promozione di un processo di pace di carattere inclusivo in Libia al fine di raggiungere i requisiti essenziali per l'indizione di nuove elezioni e per terminare così il difficoltoso processo di transizione politica. L'obiettivo è quello di evitare l'acuirsi di una nuova *escalation* di violenza nel Paese che risulterebbe deleteria in termini di interessi energetici e di sicurezza. Il livello di attenzione deve rimanere alto e deve essere allargato anche al monitoraggio della crisi politica in atto in Algeria. Bisogna ricordare che il Paese nordafricano rappresenta il secondo fornitore di gas dell'Unione europea e che condivide 2.500 chilometri di confini con il Niger e il Mali, stati nei quali transitano alcune tra le principali rotte migratorie africane. L'Unione europea deve rimanere vigile sul tema della stabilità del Nord Africa, per non rischiare l'acuirsi delle ondate migratorie cui abbiamo assistito negli ultimi otto anni. Proprio sul fenomeno della migrazione vorrei sottolineare che questo Governo ha smentito tutte le falsità che abbiamo sentito a inizio legislatura. Ci veniva detto che i flussi migratori erano incontrollabili, mentre gli ultimi dati che ci giungono dal Dipartimento della pubblica sicurezza evidenziano un risultato straordinario: nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 18 marzo 2019 sono sbarcate 348 persone

Per concludere, la strada da fare è ancora molta, ma la rotta è quella giusta. Il cambiamento in atto in Italia rappresenta anche la speranza che ne avvenga uno in Europa, perché i nostri obiettivi sono gli stessi, in Italia come in Europa: far sì che le azioni e le decisioni politiche siano realmente siano realmente a beneficio dei cittadini e a tutela dei loro interessi e della loro sicurezza. Un Governo vicino ai bisogni dei cittadini che fa sentire la propria voce in Europa è la migliore garanzia di un reale cambiamento delle istituzioni comunitarie.

e allora, ancora una volta, le riproponiamo la necessità che queste discussioni, se vogliamo che il Parlamento svolga effettivamente la propria funzione d'indirizzo, luogo in tempi utili affinché il lavoro del Governo sia in grado di interloquire sulla costruzione del Consiglio europeo; questo diventa un rito, anche abbastanza formale, che non consente al Parlamento di svolgere fino in fondo la propria funzione. I tempi a mia disposizione, che abbiamo presentato, non mi consentono di affrontare tutti i temi. Stiamo comunque discutendo di questioni rilevantissime per il nostro Paese e per ora, signor Presidente, non siamo in un anno bellissimo per l'Italia,

ci preoccupa che la dinamica delle nuove assunzioni sia legata a un dato di precarietà, dato che la media delle assunzioni è sotto i dodici mesi. Sarà il Governo del cambiamento, si saranno realizzate e starete realizzando grandissime cose: tuttavia,

dato che lo abbiamo già detto più volte nelle discussione precedenti, siamo convintissimi della necessità di un cambiamento profondo delle politiche europee. L'austerità, le politiche sul credito e quelle bancarie hanno prodotto danni e non risolto problemi per il nostro Paese. Tuttavia, la domanda che già le hanno rivolto altri colleghi è anche la mia: per attuare il cambiamento nelle politiche europee, come intendete rapportarvi agli altri Paesi europei? Qual è la vostra politica di relazioni? Come intendete rilanciare un diverso europeismo? Ogni giorno, non ci facciamo mancare la dichiarazione di un rappresentante del Governo o di un Vice Presidente del Consiglio che mette in discussione quanto lei ha detto in

Presidente, si deve porre questo problema in nome di tutti noi italiani. Deve risolvere questo problema; diversamente le nostre

perché qui ci potrebbe essere un impegno comune a lavorare per cambiare quella politica europea. Lo utilizzi; chieda più coerenza al suo Governo; sia coerente.

Ci sono state - sono state evocate da altri colleghi - grandi manifestazioni. Bisogna dare una risposta. Prenderete una posizione per dire che la programmazione sulla riduzione dei gas della Commissione è troppo timida? Chiederete che si riesca ad arrivare - come è indispensabile - per il 2030 al dimezzamento? Diversamente nel 2050 non arriveremo mai Presidente, farete anche un piano energetico in Italia che ci consentirà di gestire questa politica? Infine, sulla Cina

chiarendo che ci sono aspetti tuttavia che non riguardano le politiche commerciali europee. I porti, infatti, in Europa si fanno concorrenza e noi abbiamo diritto di tutelare gli interessi italiani e a fare

proprio il posizionamento dell'Europa nei confronti della Cina e una serie di misure - io ne ho elencate almeno dieci - che riguardano la nuova politica dell'Unione europea per tutelare le imprese e la sicurezza del Continente europeo rispetto alla nuova Cina. Signor Presidente, sono stato in Cina decine di volte quand'ero delegato al commercio, nei primi anni del 2000; ero anche a Doha al WTO quando fu accolta la Cina. Ma quella Cina non era questa Cina.

la Via della Seta, che lei ha derubricato a un fatto economico-commerciale, non ha invece più nulla di commerciale. Infatti - come lei sa bene - la politica commerciale è esclusiva competenza dell'Unione europea. Non c'è alcuno di questi accordi che sia commerciale; invece, sono ben altro. Nel MOU sono citati diversi settori strategici. Le infrastrutture, l'energia, le telecomunicazioni sono citate nel MOU perché riguardano questa materia, non avere valore legale per noi, come non ce l'hanno nemmeno i bandi della TAV, per dissolvenza giuridica, e come non ce l'ha il contratto di Governo tra voi; ripeto che non ha valore legale giuridico, ma per la Cina ha un valore strategico fondamentale. Nel 2017 Xi ha imposto una riforma dello statuto del Partito Comunista Cinese che ha posto la Via della Seta come obiettivo strategico del suddetto Partito per cambiare le sorti del mondo.

i concetti del leninismo, ma la Via della Seta come strumento strategico per imporre il dominio della Cina, ribaltare il quadro delle alleanze e far soccombere l'Occidente. Subito dopo, non a caso, la Via della Seta è diventata pertinenza del Ministero per la sicurezza nazionale. Nel contempo, dal 2015 in poi, con quattro revisioni legislative è stato imposto che qualunque cittadino e qualunque azienda cinese nel mondo hanno l'obbligo - non la facoltà, ma l'obbligo - di rispondere ai Servizi di sicurezza e militari, fornire loro informazioni e assistenza. Quindi, lei si sta confrontando con una potenza di questo tipo che ha il monopolio dei trasporti tra l'Asia, l'Africa e l'Europa, e avrà le chiavi

dopo tutte le trattative segrete, e direi anche oscure, al punto tale che, signor Primo Ministro, la stessa maggioranza le presenta un documento anomalo. Nel documento della maggioranza c'è scritto che il Governo si impegna «a confermare che sono state effettuate le necessarie verifiche». Oggi? Deve confermare che sono state effettuate le necessarie verifiche: quindi non l'avete comunicato né ai Ministeri né alla maggioranza? Il Governo si impegna «ad assicurare che gli accordi ad esso collegati non interessino aspetti economico-commerciali di valenza strategica». La maggioranza chiede al Governo di impegnarsi in questo senso? Quindi, voi per primi ben sapete e siete consapevoli che riguarda gli assetti di politica strategica del nostro Paese! Nello stesso documento di maggioranza che bisogna «garantire che ognuno degli strumenti bilaterali in via di sottoscrizione sia compatibile col mantenimento delle tradizionali relazioni transatlantiche». Garantirlo oggi? Non li avete esaminati in questi sette mesi? E poi c'è l'ultimo impegno che riguarda i nuovi rapporti. Bene, signor nel documento in Consiglio europeo ci sono dieci punti, il primo dei quali era stato portato all'attenzione di questo Parlamento dal rapporto dei Servizi di sicurezza che lei stesso ha firmato poche settimane fa. fa. Lì c'è scritto che una delle azioni fondamentali per tutelare gli interessi nazionali è il regolamento - lo ha firmato lei il rapporto - sullo *screening* degli investimenti esteri in Europa. Mi chiedo allora: perché il suo Governo si è opposto decisamente al regolamento che la stessa relazione al Parlamento dei Servizi di sicurezza ritiene fondamentale? Ha già una postura filocinese che contraddice i suoi stessi documenti e i rapporti sulla sicurezza nazionale al Parlamento? Perché il Governo si è posto in una posizione insieme alla Grecia, di fatto filocinese, sul Venezuela? Perché il Governo si è opposto, a differenza di quello che dice - perché questo a me risulta - che siano riprese le relazioni transatlantiche, a cominciare dall'abbattimento delle tariffe industriali di prioritario interesse del nostro Governo? Perché il Governo non sa quello che fanno i suoi rappresentanti in Europa? Aggiungo che nell'elenco del Consiglio europeo si parla di argomenti fondamentali: si parla di economia digitale, di tassazione dell'economia digitale, di nuove regole sulla cibernetica, cibernetica, sulla sicurezza nazionale e sulle imprese straniere che investono in Europa e che devono rispettare la legge sugli aiuti di Stato; si parla di nuove regole per quanto riguarda l'intelligenza artificiale con un piano dell'Europa per diventare finalmente la prima potenza globale sull'intelligenza artificiale. Si parla anche del Fondo sovrano per tutelare le industrie europee dalla Cina. Di tutto questo lei non ci dice nulla. Noi vorremmo sapere come si comporterà l'Italia in Europa in tale contesto e su queste argomentazioni vitali per la sicurezza nazionale e per la tutela del nostro sistema industriale.

la prima minaccia è quella cibernetica - e lei non ci dice nulla su questo e abbiamo alla porta il bando dei 5G che viene invece tutelato in sede europea - e la seconda è l'azione predatoria di alcuni Paesi che stanno comprando gli assetti strategici del nostro Paese.

Non avete verificato, oppure, se lo avete fatto, è perché condividete la strategia imperiale e predatoria della Cina in Europa.

Signor Presidente del Consiglio, al secondo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio europeo vi è la questione dei cambiamenti climatici. Il Consiglio dovrà fornire gli orientamenti sulla direzione generale e sulle priorità politiche che serviranno a definire, entro il 2020, la la strategia di lungo termine che l'Unione europea dovrà perseguire per restare in linea con i parametri previsti dall'Accordo di Parigi. di Parigi. L'Italia arriva a questo appuntamento a dir poco con una posizione non chiara. Anzi, possiamo senz'altro dire che su moltissimi aspetti è una posizione assolutamente contraddittoria. D'altronde, le premesse erano inequivocabili e non lasciavano alcuna speranza per una inversione di tendenza. La Lega a guida di Matteo Salvini

e ha respinto da par suo il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sottoscritto da 195 Paesi.

sui provvedimenti per l'efficienza energetica, sulle emissioni di CO2 delle automobili, sul regolamento per la contabilizzazione dei gas effetto serra per gli obiettivi climatici 2030, nonché sulla direttiva per la riduzione della plastica monouso. Non finisce qui: finisce qui: il 14 marzo scorso il Parlamento europeo si è già espresso nei contenuti del prossimo Consiglio europeo e sulla questione dei cambiamenti climatici ha approvato - come immagino sappia - a larga maggioranza, con esplicito riferimento alla mobilitazione Fridays for future, le risoluzioni sul clima e sull'aria pulita. Ebbene, Presidente, anche in quel caso, in particolare sulla risoluzione più importante, che è quella sul clima, la Lega ha votato ancora una volta contro quello che nel testo descritto va ad individuare un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'Accordo di Parigi.

Il risultato, Presidente, è che abbiamo fatto zero con l'operazione del Parlamento europeo e rischiamo di fare lo stesso il 21 e il 22 marzo su punti imprescindibili che erano presenti in quella risoluzione. Mi riferisco - per esempio -tra i tanti punti, alle politiche energetiche, alle politiche industriali e alle politiche di ricerca e innovazione. Zero non è soltanto un riferimento algebrico per significare la nullità delle scelte e delle azioni intraprese per fronteggiare il contesto globale e dunque il mutamento climatico; ma zero, Presidente, è il voto che si meritano questo Governo e questa maggioranza per l'assenza in tematiche così importanti e decisive per il nostro Paese. Signor Presidente, la sua maggioranza dice un giorno sì e l'altro pure che vuole incentrare tutte le politiche sulla giustizia sociale. Ebbene, Presidente, c'è un nesso fondamentale tra la questione dell'ambiente e la questione della giustizia sociale: la maggior parte dei migranti che premono alle nostre porte è rappresentata da esuli ambientali che fuggono dalla siccità,

Se lo faccia spiegare dal ministro Costa, se avrà la grazia di venire a rispondere a qualche interrogazione in quest'Aula o almeno in Commissione. Questi dati sono stati forniti da centinaia di studiosi raccolti in questi giorni, fino al 15 marzo scorso, nel rapporto sottoscritto e presentato all'Assemblea dell'ONU di Nairobi.

a Belluno. Ha portato la testimonianza sulla tempesta Vaia, che non si era mai vista in Veneto. Guardi, Presidente, il 7 dicembre, nel cuore delle Dolomiti, a Pieve di Cadore, si sono ritrovati relatori, studiosi e amministratori e tutti hanno concordato che quel fenomeno cataclismatico dipende fondamentalmente dal cambiamento climatico; eppure, ci sono ancora i negazionisti. L'assessore all'ambiente della Lega della Regione Veneto, in un dibattito con il sottoscritto, ha detto qualche giorno dopo quel cataclisma che non c'è alcuna evidenza scientifica che leghi il mutamento climatico con l'azione antropica. Di questo stiamo parlando. Dite di esserlo anche voi, soprattutto i colleghi del MoVimento 5 Stelle, ma non è con gli *slogan*, con le bugie e con gli equilibrismi che lo si dimostra, ma con i fatti. Signor Presidente, il piano energia e clima è assolutamente inadeguato per 10.000 motivi e, quando avremo la grazia di discuterne qui o almeno in Commissione, vi spiegheremo perché. C'è bisogno di azione, signor Presidente; c'è bisogno di capire che non basta venire qui a parlare bene di Europa e di clima in quei pochissimi secondi - tra l'altro - in cui lei ne ha parlato.

occorre ridurre il consumo della benzina e del gasolio; occorre lavorare per il riuso; occorre lavorare sulle rinnovabili, sulla rigenerazione urbana, contro il consumo del suolo. La scorsa settimana milioni di giovani in tutto il mondo hanno dato vita a una straordinaria manifestazione. Li ha uniti il coraggio, l'esempio, la determinazione di Greta Thunberg, una giovane ragazza di sedici anni.

la questione della firma del *memorandum* d'intesa con la Cina, detta anche Via della Seta, ha tenuto banco nelle ultime settimane e ha coinvolto tutti gli attori della politica italiana in un sano dibattito sul futuro delle relazioni internazionali del nostro Paese, sul ruolo dell'Italia e all'interno dell'Alleanza atlantica. Per noi e per il nostro Gruppo la firma del *memorandum* d'intesa rappresenta un'importante opportunità di sviluppo commerciale del nostro Paese. La Cina sta effettuando un percorso di trasformazione economica e sociale interna, che sta portando l'emersione di una classe media corposa e un aumento della domanda dei prodotti europei. È nostro dovere, Presidente, per il bene del nostro Paese, intercettare questa domanda e aumentare la quota di esportazione italiana verso il mercato cinese. Ci tengo particolarmente a sottolineare, signor Presidente, che l'Italia esporta in Cina prodotti e beni per 13 miliardi di una quota di esportazione irrisoria, se confrontata con l'interscambio commerciale che gli altri Paesi europei hanno con il Paese asiatico. Faccio due esempi: la Francia ha esportazioni in Cina per un valore di 20 miliardi l'anno, la Germania esporta beni e prodotti per ben 87 miliardi annui. Ci chiediamo, allora, se l'Unione europea e gli Stati membri che stanno criticando il *memorandum* non temano, in realtà, una sana competizione con il nostro Paese; sana competizione che vede nel *made in Italy*, nel mercato agroalimentare e in quello del lusso dei beni fortemente richiesti dalla crescente domanda proveniente dalla Cina. L'obiettivo del Governo - e l'intesa sul *memorandum* ne è la riprova - è di attirare investimenti sicuri per il nostro Paese. Anche in questo caso sono i numeri che ci dimostrano un enorme squilibrio all'interno degli Stati europei. Nel 2018, dei circa 50 miliardi di dollari che la Cina ha investito in Europa, la Gran Bretagna ne ha assorbiti la metà, mentre la Germania si è aggiudicata una quota pari al 22 per cento, molto superiore a quella dell'Italia, stimata intorno a 15 punti percentuali. È un *trend*, questo, che il Governo si impegna a cambiare e che dimostra come sulle politiche commerciali l'Unione europea sia ben lontana dall'avere un approccio sistemico. Ci fanno sorridere, signor Presidente, i timori che arrivano da Bruxelles e che riguardano la possibile comparazione tra la situazione dei nostri porti di Trieste e di Genova e quella del Pireo in Grecia. Voglio ricordare che la Grecia è stata costretta a svendere il proprio patrimonio pubblico proprio perché lasciata sola da quell'Europa che, con le folli politiche di austerità, ha devastato il tessuto industriale della Grecia stessa. L'Italia e questo Governo - come ribadito più volte nelle ultime settimane - non hanno alcuna intenzione di svendere il patrimonio pubblico e le nostre infrastrutture strategiche. e M5S).* Ci tengo a ribadirlo a nome di tutto il Gruppo, affinché sia chiaro. L'Italia non svenderà mai nessun *asset* strategico. Per concludere, rispondo alla critica che si è sentita negli ultimi giorni e lo faccio ribadendo con forza il concetto già espresso nel corso di queste settimane. È confermato da tutte le azioni che questo Governo ha effettuato: l'Italia rimane saldamente ancorata all'Alleanza atlantica, che rappresenta la cornice naturale del sistema delle alleanze del nostro Paese; è uno strumento di assoluta importanza in termini non solo di sicurezza, ma anche di integrazione e cooperazione militare europea. Questo Governo si è dimostrato uno dei principali alleati degli Stati Uniti e non sarà questo accordo commerciale, che rientra nel perimetro dei principi di cooperazione economico-commerciali presenti in tutti i documenti europei, a modificare la naturale alleanza con Washington e ad allontanare l'Italia dal blocco occidentale e dall'Alleanza atlantica. Concludo, signor Presidente, confermando quanto detto nel mio intervento. L'obiettivo principale del nostro Gruppo in merito all'accordo in questione è investire sul rilancio del *made in Italy* e conquistare maggiori quote di un mercato - quello cinese - che rappresenta già uno sbocco importante per le esportazioni di altri Stati membri. L'Italia non fa altro che competere lealmente per sviluppare le proprie relazioni commerciali. Siamo sicuri che questo sia un bene per il nostro Paese. Allo stesso tempo, manterremo alta l'attenzione sugli investimenti e sulla difesa delle nostre infrastrutture. Il nostro Continente, che si trova proprio in mezzo a due giganti, è stato e sarà la culla della democrazia, del commercio e del turismo, ma oggi si riprende l'opportunità di non subire finalmente le scelte altrui.

Penso alla crisi economica, all'immigrazione, alle tematiche ambientali e al terrorismo. A tali sfide l'Europa di oggi non sembra in grado di dare tempestivamente le giuste risposte e ciò sta causando un significativo aumento di sentimenti di scetticismo nei confronti dell'istituzione in tutti i popoli che ne che ne fanno parte: scetticismi, paure o difficoltà oggettive che, se non adeguatamente governati, portano a scelte scellerate e potenzialmente disastrose. Penso allo spettacolo indecoroso a cui stiamo assistendo nel Regno Unito, prigioniero della Brexit, che sarà oggetto del vostro incontro, signor Presidente, e che dovrebbe rappresentare un monito per noi che abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare i nostri cittadini. Non si va da nessuna parte se si cavalcano solo le paure e non si affrontano in maniera seria e competente i problemi che pur ci sono. Venendo ai punti salienti dell'incontro a cui lei parteciperà, rappresentando gli interessi di tutti gli italiani, un ruolo preminente sarà rivestito dai temi economici, come è giusto che sia data la situazione. Signor Primo Ministro, proprio su temi economici nessuno che abbia un minimo di cognizione di causa può pensare che l'Italia, da sola, possa ottenere dei risultati veri e concreti per i nostri concittadini. Abbiamo ancora tutti negli occhi il ridicolo braccio di ferro che avete fatto e perso con la Commissione per la vostra manovra economica e pertanto auspichiamo, sin da questo Consiglio europeo, una nuova fase di dialogo e confronto con i nostri *partner*, che vuol dire non accettare supinamente i *Diktat* - come avete fatto - ma confrontarsi su provvedimenti seri e concertati. Per farlo bisogna, però, dire cose credibili e - soprattutto Come ho avuto modo di chiedere recentemente alla commissaria europea Vestager, il tema della concorrenza deve essere al centro del dibattito. Non è possibile che in Europa persista il fenomeno del *dumping* fiscale, ovvero di Paesi europei che fanno concorrenza sleale a colpi di ribassi sulle tasse, che tanto danneggia le nostre imprese. Cosa intendete fare per questo? Glielo chiedo, signor Primo Ministro, perché la vostra ultima impresa è - a quanto pare - consegnare il Paese in mano ai cinesi. Ma come, non siete orgogliosamente sovranisti? Sovranisti cinesi, forse? Dovete specificarlo, e qui mi rivolgo agli amici della Lega. Come potranno le nostre imprese, i nostri lavoratori e i nostri artigiani competere contro il gigante asiatico che non rispetta le nostre regole e che, quindi, riesce a offrire prodotti di scarsa qualità a basso prezzo? È maggiore l'*import* dell'*export*. Quindi, bene aprirsi agli investimenti cinesi, ma che ciò venga fatto con trasparenza. A proposito, se avrete la compiacenza di dirci qualcosa di più su questo accordo, non sarebbe male. Mi sembra che ci siano degli accordi bilaterali che lei oggi non ha citato (mi riferisco ai porti di Trieste e Genova). Occorre tutelare i nostri *asset* strategici, soprattutto nel rispetto dei nostri *partner* europei e delle nostre storiche alleanze. Veniamo ai temi ambientali, che finalmente sono al centro del dibattito. Voglio citare Sant'Ignazio di Antiochia, che ci dice: «Si educa molto con quello che si dice, ancor più con quel che si fa, molto di più con quel che si è». Vede, Presidente, noi rappresentanti delle istituzioni dovremo essere di esempio per i nostri concittadini. Ma, se poi un Ministro della Repubblica va in televisione a dire che ha comprato un SUV a *diesel,* come potete pretendere che gli italiani vi credano quando parlate di tematiche ambientali e chiedete loro di fare sacrifici sacrifici in questo senso? L'alternativa al *diesel* c'è e si chiama trasporto ferroviario, di cui però non si parla in nessuna delle 227 pagine della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che ha redatto il precedente Ministro degli affari europei. A proposito, signor Presidente del Consiglio, le deleghe agli affari europei le manterrà lei? Per quanto tempo? Glielo chiedo, perché avremmo parecchie questioni da affrontare, specialmente per quanto riguarda la nuova programmazione dei fondi comunitari e le relative trattative in corso, che si stanno svolgendo a Bruxelles. di trasporto ferroviario, che tutto il mondo, tranne i consulenti del ministro Toninelli, sa essere il mezzo più ecologico ed efficiente. Quindi parliamo di TAV che, in termini di competitività, creazione di posti di lavoro e miglioramento delle condizioni ambientali, è un'opportunità straordinaria che state boicottando. Come intendete rafforzare le relazioni europee se venite meno ad accordi presi? Parliamo di fatti: nell'era della globalizzazione e delle sfide ad essa legate, l'Italia da sola purtroppo non ha alcuna possibilità, mentre ora, a causa vostra, è isolata nel contesto L'apparente improvvisazione con cui avete messo in campo recenti iniziative commerciali rischia di compromettere la nostra fondamentale alleanza con gli Stati Uniti. Mi avvio alla conclusione, rivolgendovi l'invito, signori del Governo, di uscire dal *bunker* in cui vi siete rinchiusi, di smetterla di ascoltare cattivi consiglieri e di far riprendere all'Italia il suo ruolo di misura ed equilibrio nello scenario internazionale.

oggi è la festa del papà: approfitto per fare i miei migliori auguri a tutti i papà presenti in Aula e colgo l'occasione per fare gli auguri al nostro presidente, Giuseppe Conte, per il suo onomastico. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio, desidero incentrare il mio intervento sul problema del lavoro e dell'occupazione, sul problema del lavoro e dell'occupazione, visto che tra i temi che i *leader* europei affronteranno c'è proprio quello dell'occupazione, della crescita e della competitività. Le politiche di austerità hanno creato barriere sociali tra le economie più deboli del Mediterraneo, in cui lo Stato sociale è stato poco a poco smantellato, e le economie dell'Europa settentrionale, in cui i sistemi di protezione sociale hanno invece tenuto. Per il raggiungimento della convergenza economica non si sono messi in campo meccanismi e strumenti di solidarietà a livello europeo, determinando l'esplosione del fenomeno del *dumping* sociale, con un flusso migratorio intracomunitario di lavoratori verso Paesi con sistemi di *welfare* più generosi. Uno dei principi fondatori dell'Unione europea è la solidarietà: per questo è necessario creare sistemi di garanzia sociale armonizzati in tutti gli Stati membri dell'Unione europea; strumenti di sostegno al reddito, politiche occupazionali inclusive, servizi universali di assistenza e lotta alla povertà, al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei, in controtendenza rispetto alle fallimentari politiche neoliberiste e di austerità, che difficilmente potranno rilanciare l'economia nazionale. Il rilancio e la crescita europea non possono prescindere dalla tutela del lavoro nella sua accezione più ampia. La tutela del lavoro implica tanti fattori interconnessi, che vanno dalla domanda all'offerta, alla produzione industriale, alle politiche economiche, alle condizioni ambientali, alla tutela dei diritti dei lavoratori in ogni latitudine, alla conservazione dello Stato sociale. Il rilancio della crescita europea non può non porre attenzione alla protezione del lavoro e in particolare alla deflazione salariale, che agisce negativamente sulla domanda interna del Paese. Un modello di sviluppo delle relazioni industriali che vede il taglio dei salari dà solo apparentemente maggiore competitività alle aziende, ma diminuisce i diritti dei lavoratori che vengono di fatto sottopagati. Pertanto, signor Presidente, noi chiediamo che l'Europa tutta, le sue istituzioni e gli Stati membri, lavorino in sinergia con l'obiettivo dell'inclusione sociale per una crescita equa, condivisa e sostenibile, con più occupazione, lotta alla povertà, rilancio dell'economia nazionale, attraverso investimenti finalizzati alla ricerca ed allo sviluppo del tessuto economico. Particolare attenzione, signor Presidente, deve essere rivolta alle piccole e medie imprese, che sono e rappresentano il vero tessuto connettivo ed il volano

non intervengo sul dibattito, anche perché c'è varietà di opinioni ed è comprensibile; a me preme semplicemente riassumere, anche per doverosa trasparenza nei confronti del

Vorrei precisare a questo riguardo che ci siamo premurati di questa prospettiva:

con dovizia di particolari per tutti i cittadini e le imprese che potrebbero essere interessate. Poiché allo stato non sappiamo se ci avviamo a una prospettiva *no deal*, cioè a un'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo, ci siamo anche premurati con uno strumento normativo: abbiamo uno schema di decreto-legge che porteremo già domani all'esame del Consiglio dei ministri e, ove necessario, abbiamo predisposto le necessarie misure per l'ipotesi in cui non si dovesse neppure arrivare a un differimento del termine del 29 marzo e quindi ci siamo preparati anche a informare tutti i cittadini

dare sostegno e forza anche ad una nuova economia, a una nuova occasione. Gli impegni precisi, presidente Conte, sono molto chiari. Lei sa - lo ricordava prima il collega del Partito Democratico - che rispetto agli obiettivi che l'Unione europea si era data per il 2030 vi è stato un passo in avanti compiuto dal Parlamento

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del Consiglio europeo, i punti sono diversi. Il primo concerne l'occupazione, la crescita e la competitività. Presidente Conte, noi le chiediamo di andare in Europa

Con un po' di umiltà l'Unione europea dovrebbe pensare che le politiche di austerità tenute finora sono sbagliate e che la ricetta di Trump, invece, ha funzionato. La ricetta è molto semplice: investimenti pubblici, riduzione delle tasse, semplificazione e lotta alla burocrazia. Questa è la ricetta che Fratelli d'Italia chiede all'Italia e all'Unione europea.

dello scorporo delle spese di investimento nel computo dei parametri *deficit*-PIL, in modo che l'Italia e l'Unione europea possano fare investimenti massicci senza avere il problema dei vincoli di bilancio e senza andare in *deficit* per finanziare iniziative magari poco utili alla crescita. La riduzione delle tasse non è di competenza dell'Unione europea, ma dei singoli Stati. Come, però, qualcuno ha detto prima di me, si può, in sede europea, porre almeno il problema della concorrenza sleale intraeuropea di Paesi che utilizzano un *dumping* fiscale per una concorrenza europea interna che non giova all'Italia. Su semplificazione e burocrazia, noi tentiamo di fare la nostra parte in Italia, ma l'Europa non ci aiuta, avendo creato, in questi anni, burocrazia su burocrazia. Altra ricetta della strategia Trump è la guerra alla concorrenza sleale dei Paesi terzi. Sotto questo aspetto, uno dei punti del Consiglio europeo sarà proprio quello delle relazioni esterne con la Cina. Sarà l'occasione per porre il problema del *dumping* salariale e sociale che l'Europa subisce da Paesi terzi: certo, non solo dalla Cina, ma anche dalla Cina. Questo comporta che, senza quelli che Fratelli d'Italia chiama dazi di civiltà, le imprese europee avranno solamente due scelte: adeguare al ribasso la politica salariale e la politica sociale riducendo anche le spese per la tutela dell'ambiente,

salariale, sociale e ambientale che viene posto in questa fase all'Occidente. Passo ora, velocemente, alla questione Cina. Cina. Abbiamo sentito in questi giorni un po' di tutto, come il pericolo della penetrazione commerciale cinese in Occidente. Segnalo a tutti che, nel 1816, un tal Napoleone aveva detto: quando la Cina si sveglierà, il mondo tremerà. però, due secoli fa. Adesso, nel 2019, prima di parlare del pericolo cinese, magari uno dovrebbe andare a leggere alcuni dati. Stati Uniti e Cina hanno un interscambio di 600 miliardi di dollari l'anno; la Cina detiene mille miliardi di debito pubblico americano. La Cina è diventato il primo *partner* commerciale della Germania. Germania e Cina hanno

che invece andavano poste. La prima riguarda le infrastrutture strategiche. Il ministro Salvini ha detto: le chiavi di casa le teniamo noi. Giustissimo. Segnalo, però, che questo Parlamento ha bocciato sistematicamente le proposte di Fratelli d'Italia che chiedevano il possesso pubblico delle infrastrutture strategiche italiane. È una clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale su tutte le infrastrutture strategiche, sia in mano, domani, ai cinesi, che in mano, oggi, in gran parte, ai francesi. Abbiamo chiesto una visione complessiva. Anche qui, chiedo a lei, *premier* Conte: come possiamo parlare di Italia *hub* della Via della Seta e poi

di questa opportunità per porre il problema della concorrenza sleale cinese a casa nostra. Le imprese cinesi a casa nostra, in gran parte del territorio, compiono atti di palese illegalità e di elusione ed evasione fiscale che la Guardia di finanza stima in un miliardo di euro nella sola zona di Prato. Prato. Questa era l'occasione per porre anche questi problemi. Per tali ragioni Fratelli d'Italia voterà contro la risoluzione della maggioranza, non perché non capiamo l'utilità del dialogo con la Cina, ma perché reputiamo che questa sia stata un'occasione persa per porre sul tavolo, in sede europea e in sede nazionale, questi problemi.

Quante bugie. Ricordo bene le bugie sui presunti costi dell'Unione europea, le bugie sull'invasione di immigrati nel Regno Unito, le bugie sull'ingresso della Turchia nell'Unione europea. Così come ricordo benissimo le promesse: la Brexit - diceva un mio collega del Parlamento europeo dell'UKIP - porterà 350 milioni di sterline a settimana al sistema sanitario inglese; rimarremo nel mercato unico europeo e sarà un gioco da ragazzi firmare nuovi accordi commerciali con tutti i *partner* del mondo. Falso, tutto falso

così commentò l'esito del *referendum*: «Evviva il coraggio dei liberi cittadini di Gran Bretagna!!! Il cuore, la testa e l'orgoglio hanno battuto le bugie, le minacce e i ricatti. Grazie UK, ora finalmente cambierà l'Europa, ora tocca a noi». È stato un disastro. La Brexit è stata un disastro, vice presidente Salvini! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Sarebbe bello se lei lo ammettesse perché in politica si può sbagliare ma quando si sbaglia si deve avere l'onestà di ammetterlo. Ora siamo in un *cul-de-sac*. Alcuni *media* internazionali ci attribuiscono anche il ruolo di Stato membro che si opporrebbe ad una soluzione che consenta un rinvio nel Consiglio europeo. Io sono convinto che non sia così: lo dica chiaramente, presidente Conte. Il Governo italiano lavori insieme agli altri Paesi europei affinché, se ci sono le condizioni, ci sia il rinvio, se non si può completare entro il 29 marzo la Brexit.

le aziende italiane che fanno affari nel Regno Unito e le 700.000 persone italiane e gli altri europei che risiedono nel Regno Unito e che si vedrebbero, da sera a mattina, senza diritti. Stiamo parlando di una cosa esplosiva, non di un gioco da affrontare con sufficienza. Presidente, gli altri due temi sono stati trattati efficacemente dai colleghi Ferrazzi e Alfieri. Mi spiace osservare che lo spazio da lei dedicato nel suo intervento introduttivo al tema dell'ambiente e della transizione ecologica ed energetica non sia andato oltre i dieci

Vi è un punto nel Consiglio europeo che riguarda la crescita. È giusto spingere l'Europa a fare sul versante della crescita, ma il Governo italiano deve fare la propria parte. Come si può pensare

Qual è la risposta del Governo sulle zone economiche speciali? Poi viene Salvini nella mia Regione e dice: «Ma quanto è difficile arrivare in Basilicata!»; certo, se tu col tuo Governo non stanzi 450 milioni per l'elettrificazione della tratta tra Salerno,

che siamo affezionati al nostro Paese, come lo è lei, e vogliamo che il suo lavoro porti risultati positivi all'Italia e all'Europa, ma attraverso una posizione chiara e con una doppia consapevolezza.

di questo Governo e io aggiungo che forse è l'ultimo, dato che manca poco al rinnovo delle istituzioni europee. Lei invoca un autentico spirito europeo anche in questo Consiglio e siamo d'accordo con lei, perché i temi da affrontare sono certamente rilevanti, ha appena detto il collega Pittella. Vi è il doloroso distacco della Brexit, innanzitutto, con la tutela dei nostri connazionali e dei nostri interessi in quella terra e anche con uno sguardo agli effetti che essa comunque produrrà, alcuni dei quali sono stati descritti. Non sono così pessimista, però: penso che comunque il Regno Unito, un Paese di solidissime tradizioni democratiche, commerciali e culturali saprà trovare diventare un importante *competitor*, perché riuscirà a muoversi su altri terreni e accordi commerciali e internazionali che non vorrei rendessero vane tutte le nostre preoccupazioni in ordine alla Brexit.

Grazie. organizzare, che va sotto il nome di intelligenza artificiale, di economia digitale e di un cambio di paradigma totale delle nostre vite e quindi della nostra economia. Non sono dunque così convinta che quel tempo della collaborazione con la Cina, che anche in anni e decenni recenti ci ha visti protagonisti, oggi sia così

che quel grande accordo commerciale prevedeva, quindi, un dialogo con quello che poi sarebbe diventato il nuovo accordo commerciale dell'area degli Stati Uniti, del Canada e del Mexico, quello che un tempo chiamavamo il sistema commerciale più importante del mondo.

Quell'accordo commerciale vigeva proprio in un'area del mondo dove, fino a qualche tempo fa, l'Europa invocava una supremazia culturale, filosofica e politica dei diritti, della giustizia sociale delle conquiste sociali, ma invece non è in Europa e non è certo nemmeno in Cina che si è cambiata la denominazione di accordo di libero scambio. Ci è voluto Trump per definire per la prima volta - è già stato ricordato in quest'Aula - che uno scambio di libero commercio, prima di essere libero, deve essere giusto. Per giusto si intende che quel capitale umano alla base di ogni relazione economica non può essere pagato uno o due dollari. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Giusto vuol dire che quel capitale umano deve avere il giusto riconoscimento del proprio lavoro. Pertanto, nell'epoca di quell'economia così rinnovata, che somiglia tanto e forse di più a una rivoluzione industriale (che ci fa passare rapidamente dal *soft power* degli accordi internazionali allo *sharp power*, cui prima ha accennato il collega Bagnai con approfondite valutazioni), alcune guerre non si giocano più con gli strumenti tradizionali; oggi si giocano attraverso l'utilizzo anche dell'informazione di strumenti legati all'economia digitale. Questo cambia e cambierà il valore dei nostri accordi internazionali. Io so bene, come lei, signor Presidente del Consiglio, che questo accordo è solo un semplice accordo e non di più deve essere. Diversamente, gli interessi del nostro Paese entrerebbero in rotta di collisione con quell'alleanza storica che ha fatto non solo del nostro Paese ma dell'intera Europa un continente liberato dal nazismo e dal fascismo. Ci sono volute migliaia e migliaia di vite umane di giovani americani venuti su queste terre a morire anche per noi. anche per noi. Questo va annoverato nel conto economico - mi permetta di dirlo - di quell'accordo internazionale che ci vede cedere alla Cina importanti aziende

leggendo tutte le pagine di questo Consiglio europeo salta agli occhi l'ennesima contraddizione. Prima il professor Monti ha usato parole molto forti nella difesa della nostra bandiera. Bene, anche in questo Consiglio europeo ci sono ben due pagine di normative ci sono ben due pagine di normative che entro la metà del 2019 devono diventare effettive. Sono due pagine che riguardano tutta la finanza.

europea, e la nostra bandiera - che evidentemente lei e chi prima di lei e insieme a lei non ha saputo difendere per il nostro Paese - ha perso in queste due pagine di raccomandazioni, direttive e regolamenti

così come ci ha ricordato molto bene il Governo Renzi col suo decreto-legge sulle banche popolari, perché lì si doveva arrivare: far sì che il sistema del credito non fosse più dei territori, non fosse più del nostro sistema economico e sociale, ma fosse invece di questa grande finanza, di questo mercato unico della finanza che poi vede nella Cina, e forse anche in altri, il suo più pericoloso nemico. Per questo noi, votando convintamente la proposta di risoluzione di cui è prima firmataria la collega Pucciarelli, le auguriamo, il miglior lavoro possibile per la difesa di quella bandiera - professor Monti - che noi abbiamo nel cuore e stampata sulla carne.

purtroppo negativo. Prima di entrare nel tema principale di questo intervento e di questa sessione - noi abbiamo chiesto con insistenza che si parlasse anche e soprattutto della Cina, che prima non era stato nemmeno prevista devo dire che anche il nostro Gruppo invita tutti a meditare sugli esiti problematici e fallimentari della Brexit, perché quello che sta accadendo nel Regno Unito non ha precedenti: non sono riusciti né a uscire né a rientrare; rinvii, bocciature, un Governo che sopravvive a esiti parlamentari disastrosi; nemmeno la presenza di un'autorevole, tradizionale storica monarchia è riuscita a risolvere sin qui il problema. Questo lo diciamo per una meditazione. Questa Europa può non piacere, può essere da criticare, ma uscirne diventa difficile, se non impossibile, oltre che dannoso e pericoloso. Voglio dire anche al Governo, su altri temi, che ci sembra singolare il fatto che giorni fa un esponente della Lega abbia preso un'iniziativa anche simpatica e condivisibile: una certa quantità di spazio alla musica italiana. Io ascolto solo musica italiana (tra l'altro basta sintonizzarsi su una di quelle radio che fanno solo musica italiana e il problema è già risolto alla radice),

collega Morelli fa parte della Camera e non del Senato, ma occorrerebbe una via di mezzo. Se volete l'autarchia musicale, potremmo trasmettere solo Al Bano e Toto Cutugno, in senso di solidarietà per l'aggressione che hanno subito sul piano internazionale. Invece dico al Governo: difendiamo il *copyright*, il diritto d'autore, che vuol dire proprietà intellettuale, vuol dire cultura e vuol dire anche combattere le *fake news* e tutelare anche l'informazione corretta, quella che voi state sterminando con interventi sull'editoria liberticidi. Volete soltanto la Rete degli insulti, delle minacce e delle bugie, salvo poi lamentarvi quando vi si ritorce contro in maniera anche inaccettabile (e lo abbiamo visto). Dopodiché, c'è la questione del sovranismo. Io non ho capito e nessuno di noi l'ha capito; l'ha detto anche prima la collega Testor: siete sovranisti a giorni alterni, perché un giorno volete il sovranismo italiano ed europeo, e un altro giorno la subalternità. Noi abbiamo chiesto che si discutesse anche della questione cinese,

«Non è stato fatto un passaggio in Parlamento per il semplice motivo che si tratta di un testo che non costituisce un accordo internazionale e che non crea obblighi giuridici». Quindi non si sa che cosa

«Stiamo parlando» - diceva il *blog* di Grillo - «di una strategia silenziosa e lungimirante di egemonia culturale, economica, commerciale e geopolitica, che quando giungerà a maturazione sarà tanto invasiva quanto Questo sul *blog* di Grillo. Poi all'improvviso va tutto bene. Di Maio fa un paio di viaggi in Cina, c'è anche, ahimè, un Sottosegretario, credo che sia della Lega, Geraci, che non ho capito se è Sottosegretario del Governo italiano o del Governo cinese in rappresentanza in Italia,

ci vuole prima un'intesa tra l'Unione europea e gli Stati uniti sulla sicurezza digitale, un'iniziativa europea non equivoca e non frammentata in tanti piccoli

Invece noi abbiamo avuto l'atteggiamento del Presidente del Consiglio che non voleva discutere in Parlamento. Abbiamo gli Stati Uniti che reagiscono. Giorni fa hanno ipotizzato che informazioni riservate potrebbero non essere più comunicate ai nostri Servizi segreti. Con il terrorismo fondamentalista in giro, isolarsi dal sistema di sicurezza

Tra l'altro di Maio è stato a Matera, perché ci sono le elezioni in Basilicata, e ha scoperto che Matera è in Basilicata e non in Puglia. Complimenti anche a Di Maio perché nel tempo si imparano tante cose.

Ora non so se questo sia un principio giusto. Deng Xiaoping disse molti anni fa che la democrazia è una cosa troppo complicata per applicarla in Cina e che cinesi erano troppi per poter utilizzare la democrazia Noi difendiamo la democrazia e vogliamo una reciprocità di diritti con un Paese che nega diritti essenziali ai propri lavoratori e che inquina l'ambiente. Questo a noi preoccupa di questa intesa, di questo negoziato e di questo misterioso dato di fatto. Vi ricordiamo che oggi abbiamo una bilancia commerciale che vede importazioni in Italia dalla Cina per 31 miliardi ed esportazioni per 13 miliardi. Siamo certi che il *memorandum* migliorerà un dato che vede la nostra bilancia commerciale in forte passivo o arriveranno qui altri prodotti dalla Cina? Poi questa Via Via della Seta (la chiamo in italiano) è una strada di collegamento (chiamiamola strada); voi siete favorevoli come Governo a collegare l'Estremo Oriente con il cuore dell'Occidente e poi non volete fare qualche

Pechino fino a non so dove va bene, ma le merci che arrivano a Genova o che arrivano a Trieste come viaggiano verso l'Europa? Arrivati a Chiomonte ci si ferma perché c'è la pausa di riflessione: è un'assurdità. Volete le connessioni a nostro svantaggio per farci colonizzare e non volete invece le connessioni

che se Greta andasse in Cina la arresterebbero, visto il livello di inquinamento e di inerzia sul piano ambientale. Abbiamo adesso in Europa il fenomeno di discussione dell'ecologismo precoce che va bene. Allora vediamo che succederebbe se andasse in Cina. Noi abbiamo il dramma di Taranto, dove il lavoro si scontra con la salute, dove nel quartiere Tamburi le stesse famiglie hanno paura della chiusura della fabbrica siderurgica, che potrebbe cancellare il lavoro dei propri familiari, ma hanno anche paura del tumore, dei fumi e dei residui. Allora noi la Cina la vogliamo richiamare al rispetto dei protocolli ambientali internazionali, che non rispetta, portando qui acciaio che costa la metà del nostro perché prodotto inquinando e sfruttando senza nessun diritto il lavoro dei cinesi? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Mi avvio a concludere, Presidente, abbiamo anche altri impegni nella serata. Noi non abbiamo né la cinofobia, perché bisogna confrontarsi con la Cina (lo si fa da qualche millennio), ma neanche la cinofollia, che mi sembra vi abbia colpito. Noi siamo preoccupati - e per questo difendiamo le nostre nostre risoluzioni - dalla scarsa credibilità della vostra oscillante politica internazionale. Lo dico anche agli amici della Lega, che condividono con noi tradizionalmente posizioni più serie. Noi stiamo facendo caos sugli F-35. Costano molto, sì, ma non avere più una difesa aerea nel futuro per un Paese che nel Mediterraneo è esposto alle minacce del terrorismo fondamentalista, è una scelta lungimirante secondo voi? È una scelta occidentalista? Abbiamo un Governo che non ha ancora riconosciuto in Venezuela il legittimo Governo perché siete amici di Maduro, gli ultimi castristi del mondo seduti su quei banchi. Che vergogna! C'è quindi un riposizionamento che ci porta lontani dall'Occidente, un giorno a fare i camerieri dei cinesi, un giorno a fare gli apologeti di Maduro, un giorno a negare le appartenenze alla NATO e alle alleanze occidentali. Noi siamo per il sovranismo vero, quello dell'Italia e quello dell'Europa, non subalterno a nessuno. Qualcuno pensa di avere una corona in testa dai cinesi? Avrà un collare per essere trascinato al guinzaglio e noi a questo diremo sempre no.

18,48)** DI NICOLA *(M5S)*. Signor Presidente del Consiglio, condividiamo pienamente la sua visione sull'agenda dei problemi all'esame del Consiglio europeo, soprattutto apprezziamo che lei abbia illustrato la necessità, per l'Unione europea, di farsi guida dei processi di cambiamento in atto non solo sul continente, ma anche su scacchieri internazionali più complessi e globali. Dai cambiamenti climatici ai temi posti dalle pratiche di disinformazione, che vedono protagonisti non solo singoli individui, ma anche Stati di primaria importanza, ma soprattutto sul fronte dell'economia e della competitività, che con il fallimento delle ricette economiche neoliberiste, piegate all'austerità, pone all'ordine del giorno l'urgenza di un cambio di approccio e visione sugli andamenti dell'economia mai come oggi bisognosa di politiche espansive fondate sul sostegno della domanda, sul rilancio degli investimenti e sul contrasto alla disoccupazione e alle povertà. Un cambio di passo tanto più necessario alla luce dei mutati scenari internazionali, che negli ultimi mesi hanno visto la ricomparsa di vere e proprie guerre commerciali Paesi che, a causa della globalizzazione dei mercati, hanno velocemente minato la stabilità economica internazionale. Scenari sempre più multilaterali che impongono la necessità di governare gli inevitabili processi di apertura ai nuovi mercati, come quello cinese, che rappresenta un'occasione imperdibile per le nostre aziende e le nostre economie. Plaudiamo perciò alla decisione del nostro Governo di voler regolamentare e guidare queste ineludibile cooperazione avendo come obiettivo la salvaguardia del nostro interesse nazionale e dei valori e principi su cui si fondano le nostre economie e la nostra società. Un'iniziativa necessaria, come si vede, che ha tuttavia suscitato critiche da parte europea, americana e da parte delle opposizioni. Critiche incomprensibili e infondate, a ben vedere. Vediamo perché. alle critiche in ambito europeo, l'approccio italiano, lungi dall'essere una fuga in avanti al di fuori dell'approccio comune europeo, getta le basi per una migliore cooperazione Europa-Cina, formalizzando, anche a livello bilaterale, la cornice legale multilaterale europea di tutti i futuri accordi economici e commerciali. Nessuno ha protestato quando altri 14 membri dell'Unione europea hanno stipulato analoghe intese con la Cina. Si pensi solo a quella greca sul porto del Pireo o quando la Germania - pensate, la Germania ha fornito alla Cina il *terminal* ferroviario europeo della nuova Via della Seta. Forse a qualcuno disturba l'idea che l'Italia accresca l'*export* verso la Cina, erodendo fette importanti di mercati altrui. sul fronte americano, il *memorandum* in questione non è un accordo politico internazionale, ma un'intesa economica e commerciale che non mette assolutamente in discussione la fedeltà atlantica del nostro Paese, né favorisce in alcun modo le strategie di non solo perché non c'è alcun risvolto geopolitico militare, ma nemmeno alcun rischio per la sicurezza italiana e alleata. Ma forse la cooperazione con la Cina in ambito delle telecomunicazioni rappresenta un problema per gli interessi commerciali delle grandi aziende americane (telecomunicazioni peraltro escluse da questo *memorandum*). Sulle critiche delle opposizioni, lungi dallo spalancare le porte a invasioni, colonizzazioni e svendite, noi stiamo mettendo regole e paletti a una penetrazione economica cinese in Italia che è stata avviata dagli ex presidenti Renzi, Gentiloni Silveri e Berlusconi, anche in settori strategici. Pensiamo al porto di Vado Ligure, alle partecipazioni cinesi in Ansaldo Energia e Autostrade, tralasciando le partecipazioni nella moda e nel calcio. Infine, il *memorandum* garantisce esplicitamente cooperazione economica e commerciale con la Cina per le imprese italiane; per il *made in Italy* rappresenta un'occasione imperdibile di aumento dell'*export* verso un mercato in crescita come quello cinese, dal quale sia detto senza infingimenti - ci aspettiamo, in un tempo congruo, la capacità di mettersi in linea con i migliori *standard* europei in tema di equa concorrenza e garanzie sul lavoro. Dei tanti altri, fondamentali temi oggetto del Consiglio europeo, vorrei soffermarmi, nel breve tempo rimasto, sull'equità economica e sociale; tema fondamentale per il MoVimento 5 Stelle e per l'azione del Governo del cambiamento da lei guidato. Riformare, ridistribuire in forme più eque il reddito: ecco le parole d'ordine che possiamo e dobbiamo portare al centro del dibattito europeo. La riunione del Consiglio che tra un paio di giorni la vedrà impegnato è sicuramente l'occasione giusta per allargare e rafforzare questo nuovo corso. un nuovo corso per l'Europa. Dobbiamo avere il coraggio, l'orgoglio di dirlo e invocarlo; un nuovo corso in cui l'Italia può farsi levatrice e tutrice, consentendo a chi all'Europa vuole continuare a mantenere davvero fede, di tornare a credere allo spirito delle origini, agli ideali e ai capisaldi del Manifesto di Ventotene, per rinnovare l'impegno di pace e giustizia sociale tra i popoli, liberati dagli equivoci della peste mercatista che ha visto idolatrate le merci e i capitali e la loro libera circolazione e sempre più sacrificati e calpestati i diritti sociali sociali di cittadinanza, nonché i livelli di vita e la capacità di reddito di milioni e milioni di cittadini. Nel nome della concorrenza senza regole, signor Presidente, del mito del profitto sfrenato, per aziende e imprese che stanno perdendo sempre più di vista la loro funzione sociale, vediamo come stanno andando le cose nel nostro Paese (anzi, come sono andate sino a questo momento), dove questa competizione sleale, che abbisogna sempre più di abbattimenti di costi, si è scaricata infine soprattutto sulla parte debole delle sue componenti economiche, quella del lavoro e del suo valore; una componente che, complici cedimenti sindacali e la mancanza di rappresentanza politica, continua a pagare i prezzi più alti. Una situazione aggravata certo dall'introduzione dell'euro, causa gli accordi di assoluto svantaggio contrattati dagli allora nostri rappresentanti di Governo, con quegli effetti finali drammatici sulle retribuzioni citati dal Presidente del Consiglio, come come ha chiarito qualche giorno fa un rapporto della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, che ha messo a confronto le attuali retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti italiani con quelle del passato, paragonandole anche alle altre dei grandi Paesi europei. Morale: in Italia, nel periodo compreso tra il 2010 e il retribuzioni annuali hanno subito una perdita di 1.059 euro, mentre quella del lavoratore dipendente tedesco è salita - al contrario - di ben 3.825 euro l'anno. Stando così le cose, signor Presidente, ci chiediamo per quanto tempo ancora potremo reggere il quadro squilibrato delle competizioni globali di un sistema di regole che ai Paesi dell'Unione impedisce di utilizzare gli strumenti tradizionali per rilanciare l'economia in crisi. Per colpa degli assurdi vincoli di bilancio derivanti dal *fiscal compact* non c'è più la possibilità di rilanciare l'economia in *deficit,* tanto più nel nostro Paese, dove il nodo scorsoio del debito pubblico rischia di ipotecare persino il destino delle prossime generazioni. È per queste ragioni, signor Presidente del Consiglio, che dall'Europa ci aspettiamo un colpo d'ala, quel famoso nuovo corso di cui parlavo in precedenza. Con gli impegni da lei presi oggi in quest'Aula, siamo sicuri lei saprà portare avanti con determinazione le nostre istanze sia nel vertice bilaterale, sia in quello previsto dall'agenda europea per il prossimo 9 aprile con gli esponenti del Governo cinese, i cui contenuti saranno anch'essi oggetto del prossimo Consiglio europeo.

Colleghi, nella giornata di oggi, a causa di un incidente durante una competizione motociclistica in corso di svolgimento in Algeria, Grazie. rispetto alla quale vorrei esprimere il cordoglio e la vicinanza di quest'Assemblea alla senatrice Stefani e a tutti i suoi familiari. Nella certezza che la senatrice saprà superare questa difficile prova con lo spirito che l'ha sempre contraddistinta, invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento.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

nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*, per il reato di cui all'articolo 605, commi primo, secondo, numero 2, e terzo, del codice penale (sequestro di persona aggravato) trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania il 23 gennaio 2019». La relazione è stata stampata e distribuita. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio attesa la sussistenza nel caso di specie dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. Informo che sono state presentate due relazioni di minoranza, da parte del senatore Grasso e del senatore De Falco. Chiedo al relatore, senatore Gasparri, se intende integrare la relazione scritta. elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea del Senato il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore e ministro Matteo Salvini, perché, come illustra e motiva la mia relazione, riteniamo che ci sia stato il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, come dice una legge costituzionale del 1989, alla quale la Giunta ovviamente ha fatto riferimento. Come illustreremo, ci sono molte motivazioni che hanno portato a questa scelta, che la Giunta ha preso con un'ampia maggioranza. Ovviamente l'ultima parola su questo caso spetterà all'Assemblea del Senato,

non perché il Senato non ne sia consapevole, ma per chi dovesse seguirci, che questi lavori hanno una certa importanza, perché in epoche recenti non abbiamo precedenti di questa rilevanza e la discussione è sicuramente importante anche per il futuro. Vorrei ricordare che fino al 1989 esisteva la Commissione inquirente, che in Parlamento si occupava delle vicende che investivano in termini giudiziari i membri del Governo; ci fu un *referendum*

ha ridotto la tutela della casta, non l'ha ampliata, poi successivamente sono state abolite anche altre forme di immunità; sono rimaste quelle previste dall'articolo 68 della Costituzione, che non vanno confuse con quelle di cui stiamo discutendo e che riguardano le opinioni che noi parlamentari esprimiamo nell'esercizio della nostra attività. Questa di cui all'articolo 96 della Costituzione, un altro capitolo. Abolendo la Commissione inquirente, una sorta di giustizia speciale - chiamiamola così per semplicità - per i membri del Governo, questi sono stati affidati al giudizio della magistratura ordinaria, proprio per un senso di maggiore equilibrio nel rapporto tra le istituzioni. Tuttavia, per riequilibrare questo affidamento alla magistratura ordinaria ed evitare che denunce pretestuose o iniziative non fondate ostacolassero l'azione di un Governo, si è introdotto un filtro un filtro che è costituito dal tribunale dei Ministri, composto da alcuni magistrati estratti a sorte nelle varie realtà territoriali, tra coloro che hanno cinque anni di esperienza nei tribunali, ai quali viene affidata una valutazione. questo tribunale dei Ministri ha ritenuto di delegare alla Camera di appartenenza, cioè al Senato, la valutazione del comportamento del senatore ministro Salvini. Devo dire che la procura della Repubblica di Catania, come è noto, aveva chiesto l'archiviazione di questa vicenda, non ritenendo che ci fossero né reati ordinari né reati ministeriali,

il compito del Parlamento è verificare se sussistano dei requisiti indicati con precisione dalla legge n. 1 del 1989, una legge costituzionale che ha introdotto questa procedura. Mi accingo leggere la parte di questa legge che, all'articolo 9, comma 3, stabilisce che l'Assemblea, in questo caso del Senato «può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Faccio questa premessa per chiarire anche all'opinione pubblica che non siamo di fronte al privilegio di un'immunità assoluta e che non facciamo una votazione solo politica, in base ad appartenenze; c'è una valutazione anche di ordine giuridico, come la relazione motiva

il testo di 16 pagine di atto parlamentare (era necessario argomentare e motivare). Noi dobbiamo quindi trovare queste motivazioni per cui la Giunta ha ritenuto ci fossero fossero un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante oppure il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. La prima decisione che ha dovuto prendere la Giunta è stata quella di dire se si è trattato di un reato ministeriale oppure no. connesso alle funzioni di Ministro dell'interno; dopodiché non è che qualsiasi reato ministeriale può essere affidato a questa procedura. Nella relazione ci sono degli esempi: se un Ministro prende dei soldi per autorizzare un'opera pubblica, è un reato ministeriale, perché è la qualifica di Ministro che gli ha consentito di svolgere quell'azione illegale ma non potrebbe mai eccepire un preminente interesse pubblico, che non potrebbe mai esistere di fronte all'appropriarsi di soldi per interessi illeciti privati.

sia un valore che possa prevalere su altri aspetti, mentre una lesione irreversibile dei diritti (la morte di una persona o altri effetti non più recuperabili) non avrebbe potuto consentire di applicare l'esimente. Noi abbiamo quindi che certamente ci fosse una ministerialità del reato e questo credo che sia abbastanza ovvio; abbiamo ritenuto, però, che sussistessero poi le condizioni per le esimenti. Abbiamo discusso anche in Giunta sul fatto che, ripeto, non tutto può essere coperto dalle motivazioni esimenti previste dalla legge del 1989: ci deve essere un bilanciamento dei fatti. Richiamo l'attenzione - lo ripeto per la seconda volta a chi dall'esterno dicesse che il Parlamento vuole autoassolversi - sul fatto che il procuratore della repubblica di Catania Zuccaro aveva chiesto l'archiviazione, non ritenendo che ci fossero, né reati comuni, né ministeriali. Il tribunale dei Ministri ha pensato diversamente, ma rispetto a quella che sarà l'opinione del Senato, che sarà decisa con il voto di domani nell'uno o nell'altro senso, voglio dire che non dobbiamo avere il complesso dell'illegittimità delle nostre scelte, perché anche la magistratura ha discusso al suo interno con orientamenti diversi.

tale nave poteva considerarsi un luogo sicuro, essendo ancorata in porto ed essendo costantemente assistita da medici e rifornita dei generi di prima necessità occorrenti, quindi con le tutele necessarie. Va inoltre menzionato che alcuni immigrati che erano in precarie condizioni fisiche o minori non accompagnati sono stati fatti sbarcare durante quella fase. In altri termini, non sono noti danni irreversibili che siano stati subiti. Dopodiché bisogna anche dire che l'immigrato che arriva in Italia con queste modalità non ha una totale libertà di circolazione: deve andare negli *hotspot,* deve essere identificato, per cui anche il concetto di libera circolazione ha delle limitazioni che le stesse convenzioni internazionali hanno tranquillamente ritenuto praticabile (penso all'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Non c'erano quindi diritti irreversibilmente lesi. Per quanto riguarda le altre questioni si è anche detto che, ad esempio, non c'era un atto collegiale del Governo. Il Governo non avrebbe preso una decisione e non ci sarebbe un pezzo di carta che registra questo.

trattenuti, hanno preso le mille strade che hanno scelto. Ma anche il trasferimento dall'*hot spot* di Messina a Rocca di Papa non avvenne per loro scelta. Furono messi su dei *pullman* e portati lì. A chi contesta la

E non cito, per economia di tempo, le frasi di totale condivisione della politica del Governo in materia di immigrazione in riferimento al caso Diciotti. Quelli che dicono che non ci sono gli atti di collegialità, dicono una castroneria,

Quindi, c'è un intervento del Presidente del Consiglio, molto chiaro, di piena e totale condivisione collegiale del Governo. Lo sottolineo perché è importante, ai fini della motivazione che la legge costituzionale Le frasi del presidente Conte le trovate nella relazione, ma voglio anche ricordare che il Presidente del Consiglio è più volte intervenuto sul tema dell'immigrazione nelle politiche del Governo, e ne ha parlato anche oggi, in verità. Era intervenuto il 5 giugno 2018, quando si è insediato, qui nell'Aula del Senato; il 27 giugno, in vista di un Consiglio europeo; il 16 ottobre, sempre del 2018 e l'11 dicembre 2018. Egli è intervenuto molte volte sulle politiche di immigrazione, ribadendo indirizzi più severi rispetto a quelli dei Governi precedenti.

agli eventi. Avviandomi alla conclusione e dovendo necessariamente rinviare alle considerazioni scritte, rilevo che la memoria del ministro Salvini contiene considerazioni importanti, incluse le preoccupazioni che dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza (nel mese di agosto, a Ferragosto, se ne tiene una tradizionale riunione) erano emerse circa il rischio di

anche nella precedente legislatura. Quindi, noi riteniamo che tutto ciò (gli interventi del Presidente del Consiglio, la memoria del ministro Salvini, l'esame dei fatti, le circostanze che la legge ci invita a guardare) sia chiarissimo.

pienamente rispettato. In alcune altre relazioni vedo citate sentenze della Corte costituzionale che riguardano l'articolo 68 della Costituzione. Ho visto giuristi illustrissimi confondere giornali l'articolo 51 del codice penale, che qui non c'entra, con l'articolo 96 della Costituzione. Ma di questo avremo tempo di scrivere e di parlare. Abbiamo raccolto una serie di gemme giuridiche veramente fenomenali, che dimostrano come non si sia valutata la questione specifica. Ma questo lo scriveremo in letteratura, quando sarà tempo. Ora, però, dobbiamo giudicare la sussistenza di questi requisiti, come la legge ci impone. Quindi, questa non una è decisione puramente politica, come qualcuno ha detto e scritto, ma una valutazione che deve fondarsi sul rispetto di quell'area grigia, dove potrebbe esserci un reato, se non ci fosse, però, un principio di interesse preminente che va a bilanciare

riunioni dove ciascuno ha potuto prendere la parola più volte affinché, poi, l'attività istruttoria arrivasse in Aula svolta con grande serietà e precisione. Io mi auguro che non ci siano casi futuri, saranno giudicati con il rigore che ogni caso deve avere. Signor Presidente, ho concluso e la ringrazio per la pazienza, ma il caso ha una sua rilevanza. abbiamo scritto questa relazione, per la quale ringrazio molto gli Uffici che hanno dato una grande collaborazione in termini di competenza e di sapienza giuridica. Voglio dire anche a lei, signor Presidente, a orgoglio del Senato, che, oltre a noi senatori, a noi senatori, che facciamo la nostra parte, gli Uffici, che fanno ricerche giuridiche e approfondimenti, sono preziosi. Noi riteniamo di aver scritto una relazione che anche ai fini con cui si guarderà questa vicenda, potrà rendere orgoglioso il Senato del suo lavoro e delle sue valutazioni. Confido, quindi, nei colleghi per l'approvazione della proposta della Giunta, che come relatore vi ho illustrato, di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore e ministro Matteo Salvini.

integrarla e spero di avere lo stesso tempo concesso al relatore di maggioranza ai fini dell'illustrazione. Onorevoli colleghi, il tribunale dei Ministri di Catania ha ravvisato nei fatti del caso Diciotti un'ipotesi di reato e su quella chiede a quest'Assemblea se autorizzare o meno il procedimento penale nei confronti del ministro Salvini. Le conclusioni della relazione di maggioranza presentano, a mio avviso, errori di valutazione e costituiscono un precedente che, a vantaggio di tutti, è bene che non si crei. Il delitto contestato è il sequestro di persona aggravato, l'articolo 605 del codice penale che protegge, ai sensi degli articoli 2 e 13 della Costituzione, come diritto inviolabile della persona, la libertà personale, che non può sopportare alcuna restrizione «se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». In particolare, i giudici ritengono che il ministro Salvini abbia commesso un sequestro di persona ai danni dei naufraghi della nave Diciotti con l'ordine impartito verbalmente di non farli sbarcare,

e di completare il coordinamento dell'evento con l'indicazione di un luogo sicuro o di una località sulla terraferma dove le operazioni di soccorso si considerino concluse. Nella sua relazione, il presidente Gasparri ha svolto, a sostegno del diniego di autorizzazione, argomentazioni, con tutto il rispetto, a mio avviso infondate, per giustificare il perseguimento di un preminente interesse pubblico rispetto alla privazione della libertà personale. Non vi erano, nel caso Diciotti, i presupposti di alcuna controversia internazionale che giustifichi il blocco dello sbarco e comunque un eventuale contenzioso fra l'Italia e Malta avrebbe dovuto essere trattato secondo le norme e le consuetudini, ad esempio attraverso un arbitrato o il ricorso alla Corte internazionale di giustizia. Ebbene, non risulta che l'Italia abbia intrapreso alcuna di queste iniziative. In realtà, le Autorità italiane chiedono ai Paesi membri dell'Unione europea di attuare una redistribuzione dei migranti a bordo della Diciotti e la relazione del presidente Gasparri individua proprio questo come l'obiettivo perseguito dal Governo, cioè il tentativo di superare il Regolamento di Dublino a favore di politiche che prevedano logiche diverse di distribuzione a livello europeo dei migranti. Questo è condivisibile e legittimo, ma trattenere esseri umani a bordo di una nave italiana per fare pressione politica sull'Europa al fine di cambiare i regolamenti, ebbene, è del tutto illegittimo. La prova dell'intento di strumentalizzare il caso Diciotti è data dal fatto che i contatti, a livello europeo, iniziarono ancor prima che la nave fosse ormeggiata a Catania, sin dal 16 agosto, come risulta dagli atti, per ottenere in modo forzoso la «volontaria redistribuzione», senza peraltro riuscirci. Solo il 25 agosto, quando si acquisisce la disponibilità dell'Albania, dell'Irlanda e della CEI, veniva data l'autorizzazione allo sbarco. Risulta quindi dagli atti in maniera incontrovertibile che l'ordine di non far sbarcare i naufraghi sia stato emesso per esercitare una pressione nei confronti degli altri Stati dell'Unione europea. Una forma di coazione morale che potrebbe arrivare a configurare il reato di sequestro di persona a scopo di coazione previsto dall'articolo 289-*ter* del codice penale. Diversamente dal presidente Gasparri, che la qualifica come preminente interesse pubblico, il ministro Salvini utilizza nella sua memoria difensiva proprio la tesi, già smentita, della controversia internazionale, ma per giustificare la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante. Come può farlo, quando, proprio attraverso il comportamento del Ministro, si sono violati gli obblighi internazionali del salvataggio in mare, che assumono un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna, proprio ai sensi degli articoli 2, 10, 11 e 117 della Carta costituzionale? Anche ammettendo la tesi della controversia, rimane il fatto che l'Italia era la titolare dell'evento SAR (*search and rescue*), ossia del salvataggio mare, e doveva portare a compimento le operazioni proprio con l'indicazione del posto sicuro e il conseguente sbarco.

che interrompe una procedura amministrativa, posta in essere dal ministro Salvini soltanto sulla scorta di valutazioni e finalità politiche. Il Ministro non avrebbe pertanto dovuto né potuto interferire nelle determinazioni del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, se non per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, rientranti - questi sì - nelle sue funzioni. Eppure lo fece, senza alcun atto scritto né alcuna palese motivazione, in assenza di qualsiasi emergenza di sicurezza nazionale o di infiltrazione terroristica. Perché l'ha fatto? Cosa l'ha spinto ad autorizzare lo sbarco solo il 25 agosto, dopo ben dieci giorni dal salvataggio? L'obiettivo, fallito miseramente, era sin dal principio quello di mostrare i muscoli in Europa, di tenere come ostaggi i naufraghi per affermare la svolta politica in materia di gestione dei flussi migratori. I diritti fondamentali delle persone riconosciuti dall'ordinamento possono essere limitati, ma solo se lo impongono esigenze insopprimibili di rango costituzionale e non una qualsiasi forma di strategia politica, per di più di medio e lungo termine. Sulla natura ministeriale del reato il relatore Gasparri propone una tesi bizzarra e priva di precedenti giurisprudenziali, che contrasta frontalmente con l'intero *corpus* normativo. Perché un reato possa qualificarsi come ministeriale devono verificarsi due circostanze: l'autore del reato nel momento in cui questo è commesso dev'essere un membro del Governo o il Presidente del Consiglio e deve sussistere un rapporto di connessione tra la condotta che configura l'illecito e le funzioni esercitate dal Ministro. È quindi paradossale sostenere che la configurazione di ministerialità di un reato si arresti sulla soglia della lesione dei diritti fondamentali, quando il bene protetto dalla norma che si assume violata è proprio uno di quei diritti come la libertà personale. Non si può giustificare che per un fine politico un membro del Governo possa privare qualcuno della propria libertà personale o della libertà di circolazione per un tempo apprezzabile, anche se non in maniera irreversibile, senza poi affrontare un processo. La tesi del relatore sembra motivata più da opportunismo dialettico-politico che da motivazioni giuridiche, alle quali il Senato deve invece rigorosamente attenersi. Spetta all'Assemblea, in difesa del principio della separazione dei poteri, valutare se la condotta del Ministro che in astratto configura reato (se lo sia in concreto poi è prerogativa del potere giudiziario deciderlo) sia giustificata da un interesse pubblico di rango costituzionale preminente, vale a dire prevalente su quello violato dalla condotta. Questo non è assolutamente il caso perché si è dimostrato ampiamente che l'interesse alla sicurezza delle frontiere che si è inteso tutelare non entra affatto in gioco quando la scelta è se fare sbarcare da una nave militare italiana - territorio dello Stato - 177 disperati e non invece cannoneggiare un invasore che stia sbarcando sulle nostre coste con carri armati e artiglierie. I rischi connessi a un'erronea valutazione da parte del Senato sono altissimi. Si sarebbero fatte le stesse valutazioni se il caso di specie non fosse relativo ad alcuni cittadini stranieri su una nave, ma a una scuola piena di studenti? Sono ipotesi che ci dobbiamo porre. Sottrarre il ministro Salvini al giudizio della magistratura - badate bene, al giudizio, non alla condanna - rischia di trasformarsi in un precedente, a mio avviso, pericolosissimo. non possiamo sapere chi e per quali finalità in futuro utilizzerà questo precedente, che genera una sostanziale immunità per giustificare azioni simili o addirittura peggiori. La libertà personale - lo ribadisco - è un diritto inviolabile e come tale preminente rispetto a qualsiasi fine politico. Per questi motivi - qui solo accennati, ma trattati più ampiamente nella relazione depositata propongo ai colleghi senatori di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini.

Presidente, intendo integrare e illustrare brevemente la relazione che ho depositato. Presidente e colleghi, la discussione e la votazione sulla richiesta di autorizzazione a procedere sono un momento cruciale della vita istituzionale e politica di questo Paese, non tanto e non solo per quel che riguarda la ipotizzata responsabilità giuridica del ministro Salvini, come in conclusione diceva il relatore che mi ha preceduto, che non spetta al Senato dichiarare, ma per i principi e fondamenti stessi dello Stato che questo caso mette in discussione. La legge costituzionale n. - cui ha fatto riferimento anche il senatore Gasparri - ha profondamente modificato il sistema previgente della cosiddetta Commissione inquirente con una procedura che escludeva totalmente l'intervento della magistratura ordinaria. Con la modifica il Parlamento assume oggi un ruolo di difesa della funzione ministeriale. Il Senato è chiamato oggi a decidere solo se il comportamento di cui è accusato il Ministro sia coperto dalle scriminanti previste dall'articolo 9, presupposti - noi lo sappiamo - sono la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo: Per riconoscere l'esistenza dell'esimente si deve effettuare una comparazione, come è stato detto, tra il sacrificio dei diritti compressi ed usati come mezzi rispetto al fine perseguito, verificando in concreto la prevalenza (se c'è) di quest'ultimo. in questo caso la sottrazione al giudice naturale costituisce una deroga compatibile con i principi fondamentali dello Stato democratico di diritto. La comparazione deve essere effettuata secondo criteri di ragionevolezza, razionalità e proporzionalità e per una durata temporale limitata allo stretto indispensabile. Si tratta di effettuare un'operazione, per così dire, di pesatura obiettiva degli interessi in gioco, che però nella relazione di maggioranza, di fatto, non esiste assolutamente. La relazione lascia intendere che la semplice azione di Governo sia di per sé interesse pubblico preminente; ed era ancora più chiara in questo senso la prima versione (ma il nascondimento è molto modesto). Siamo di fronte a una concezione del potere che tenderebbe a essere svincolata da ogni criterio obiettivo e quindi da ogni controllo di legge, non sottoposta al principio di responsabilità. Tale principio è il cardine di ogni Stato di diritto, nel quale le regole contano più dei voti. Nessuno, neppure il Governo, neppure la maggioranza parlamentare *pro tempore* che lo sostiene, è al di sopra delle leggi. La scriminante politica è volta a difendere la funzione ministeriale in relazione a un interesse pubblico concreto, specifico, sempre che si verifichi anche che questo interesse sia preminente. Per la relazione di maggioranza, invece, qualunque azione posta in essere dal Governo concretizzerebbe un interesse pubblico, addirittura sempre preminente, con l'effetto paradossale - uno dei tanti paradossi della relazione di maggioranza di far incarnare nel Governo, che è il vertice dello Stato-apparato, l'interesse generale dello Stato-comunità, con una evidente torsione di senso che non sembra di poter reggere a un esame appena attento della lettera e dello spirito della legge costituzionale n.1 Di fatto, si introdurrebbe un nuovo concetto, quello di interesse governativo, del tutto disancorato da qualunque confronto e paragone che possa consentire di stabilire se vi sia o no la necessaria preminenza. La voluta confusione concettuale e terminologica giunge alle estreme conseguenze, di fatto dissolvendo non solo il concetto di «preminente», ma anche quello stesso dell'interesse pubblico, che viene assimilato senza alcun sostegno giuridico né logico a un interesse governativo, ovvero un interesse di parte, con la capacità di comprimere anche diritti essenziali, senza fare alcun bilanciamento tra diritti compressi e interesse,

e di agire secondo il proprio arbitrio anche sequestrando forse fino a 177 persone, costrette a rimanere per giorni sotto il sole nel periodo più caldo dell'anno su una nave militare non attrezzata a ospitare tante persone per un periodo così lungo qual è la nave Diciotti. Questo nonostante il meritorio interesse, tra l'altro, del comando di bordo, che ha cercato in tutti i modi possibili di alleviare le sofferenze dei naufraghi. Relativamente alla questione della responsabilità collegiale del Governo nella vicenda della nave affermata dal presidente del consiglio Conte, dal vice presidente Di Maio e dal ministro Toninelli, osservo che la Costituzione ritiene responsabili collegialmente il Presidente del Consiglio e i Ministri nel Consiglio dei ministri. Infatti i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro Dicasteri. Non vi è stato alcun Consiglio dei ministri nei giorni della vicenda Diciotti. Il senatore Gasparri ritiene di poter sostenere la tesi - a me pare piuttosto avventurosa secondo la quale non sarebbe necessario un formale Consiglio dei ministri per affermare che vi sia una responsabilità collegiale del Governo, ma va tenuto conto del fatto che, comunque, l'eventuale responsabilità politica del Governo non rileverebbe dal punto di vista penale, e l'eventuale responsabilità politica può essere anche del solo Ministro dell'interno, qualora si tratti di atti del suo Dicastero. Insomma, non si tratta di censurare un atto politico del Governo, ma un uso illegittimo di una potestà amministrativa tecnica, delegata peraltro dalla struttura competente del Ministero delle infrastrutture (Italian maritime rescue coordination centre) al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno in ordine a una decisione, non libera ma obbligata, di indicare il *place of safety* (POS) per poi effettuare lo sbarco dei naufraghi. Si tratta quindi di un atto interno a un procedimento amministrativo che, come mostrano tutte le testimonianze, il ministro Salvini ha bloccato per avere egli dapprima negato l'autorizzazione a indicare il POS già deciso,

quella nave), per aver disposto il divieto di sbarco in modo sempre e soltanto informale. L'intervento del Presidente del Consiglio rende chiaro che si tratta di una richiesta di fiducia mascherata. Il Presidente del Consiglio, ma soprattutto il capo politico del Movimento, anche attraverso il Presidente del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle del Senato, stanno minacciosamente minacciosamente avvertendo i senatori che dovessero ritenere di votare a favore dell'autorizzazione a procedere, facendoli indebitamente sentire responsabili della tenuta del Governo. Questo è grave, molto grave. Questa minaccia politica è un'arma impropria, al contrario di quello che fa pensare la relazione di maggioranza. Infatti, noi non stiamo giudicando il Governo, men che meno la sua politica dell'immigrazione o i suoi rapporti con l'Unione europea. Non stiamo nemmeno giudicando il Ministro. Dobbiamo verificare soltanto se debba essere riconosciuta al Ministro l'immunità, in quanto si sia però in presenza delle scriminanti che abbiamo legittimato la compressione del diritto di libertà di 177 persone, uomini, donne e bambini, detenuti a bordo tra il 20 e il 25 agosto del 2018. Spostare il quesito da questa amara concretezza relativa all'inutile violenza subita da 177 persone («persone» è una parola che quasi mai sembra essere presente; né nella relazione del senatore Gasparri, né nei fatti precedenti) a una questione invece astratta e generale è del tutto improprio ed evidenzia come sia impossibile non autorizzare la magistratura a procedere se ci si attiene semplicemente, si dovrebbe, ad esaminare i dati di fatto rilevanti: non a condannare, ma a valutare e a giudicare. Rimando alla relazione scritta per la disamina puntuale delle convenzioni che regolano i soccorsi in mare ricordando che l'obbligo di salvare vite umane in mare è un preciso dovere che grava su tutti gli Stati. L'ha già detto il senatore Grasso: prevale su qualsiasi altra norma, avendo l'Italia aderito alle convenzioni internazionali che regolano la materia e che, peraltro, conseguono a prassi consuetudinarie. Quindi, sono già, al di là della convenzione, diritto pubblico consuetudinario, quindi Neppure il legislatore ordinario, quali noi siamo, può eventualmente derogare a quegli obblighi. Nessuno può derogare a quegli obblighi. L'operazione di soccorso, che comprende il salvataggio, deve essere portata all'ulteriore e ultima conseguenza dello sbarco in un luogo sicuro, il che significa sbarco in un luogo dal quale le persone possono essere portate poi alle successive destinazioni. La nave non è un luogo sicuro: lo escludono espressamente le convenzioni internazionali. Non è vero quello che dice la relazione di maggioranza al riguardo. Semplicemente non è vero. Qui mi voglio limitare a ricordare il punto nodale della vicenda, ossia la mancata concessione del POS e la successiva imposizione del divieto di sbarco. Inizialmente il POS doveva, a ragione, essere individuato da Malta nel proprio territorio, essendo un luogo sicuro più vicino all'area in cui erano iniziate le operazioni di soccorso, come previsto dal regolamento dell'Unione europea n. 656 del 2014. Tuttavia, le autorità maltesi non hanno in alcun modo inteso accogliere la richiesta italiana. Poiché l'IMRCC, il Comando generale delle Capitanerie di porto, aveva ricevuto la notizia e coordinato i soccorsi, era comunque tenuto a individuare un POS nel territorio nazionale in ossequio al principio della necessaria integrità dei servizi SAR. Non ci può essere una zona vuota. Il 15 agosto e successivo 17 agosto sono state reiteratamente effettuate richieste di POS dal Comando generale delle Capitanerie verso il Dipartimento Nell'inerzia di questo Dipartimento, che è un ente tecnico delegato, lo stesso IMRCC - sembra su disposizione del ministro Toninelli - ha disposto che la nave Diciotti attraccasse a Catania, in adempimento, di fatto, degli obblighi posti dalla risoluzione MSC 167(78). A tale decisione rispose il ministro Salvini con uno dei tanti provvedimenti *social*, imponendo il divieto di sbarco dalla Diciotti. La Diciotti, come ha detto già il senatore Grasso ed è importante ripeterlo, è nave militare, è territorio italiano, a maggior ragione nelle acque interne di un porto come Catania. Quella gente era già in Italia, vietare lo sbarco non aveva alcun senso. Sbaglia ancora una volta la relazione di maggioranza quando afferma che il salvataggio dal mare si concluda quando il naufrago è a bordo. Non è così, lo abbiamo detto e lo voglio ripetere. I naufraghi sono stati usati come impropria merce di scambio in un doppio scontro con Malta e l'Unione europea, scontro che tra l'altro ci ha visti perdenti in entrambi i casi, non ottenendo né che Malta indicasse un POS, né che vi fosse una redistribuzione dei naufraghi. Il ministro Salvini aveva anche inizialmente sostenuto la tesi che sulla nave italiana vi fossero fra in naufraghi presi a bordo possibili criminali o terroristi. Questa tesi presto è stata abbandonata dal Ministro, ma fu ripresa brevemente da anonimi funzionari del Ministero il 29 gennaio scorso, funzionari che avevano addirittura sostenuto, in un comunicato stampa alla Adnkronos, che i magistrati inquirenti non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni da loro rese in tal senso. Lo stesso ministro Salvini successivamente, il giorno 31 dello stesso mese, rispondendo alle domande più volte reiterate da un giornalista, non poté sostenere che vi fossero specifici elementi relativi alla

c'è di ogni…». Secondo l'ordinamento costituzionale la sottrazione alla giurisdizione ordinaria costituisce una deroga compatibile con i principi fondamentali dello Stato solo se in concreto il comportamento che integra la fattispecie di reato sia volto a tutelare un bene giuridico costituzionale preminente rispetto a quello compresso, sulla base di una comparazione effettuata secondo criteri di ragionevolezza, razionalità e proporzionalità. Non è possibile, in assenza di questi criteri della valutazione e della comparazione, sottrarre il ministro Salvini all'accertamento dell'autorità giudiziaria. Inoltre, la relazione del presidente Gasparri, con la sua fluidità ed incertezza, appare certamente idonea a creare un precedente veramente molto pericoloso dato che la compressione dei diritti che essa sostiene potrebbe ovviamente non limitarsi solo al caso di specie o all'azione spregiudicata di un Ministro *pro tempore* ma essere invocata in futuro, in situazioni diverse ma analoghe, da altri Ministri

e dignità), che comportino temporanee limitazione della libertà personale. È quindi auspicabile che il Senato della Repubblica riaffermi che l'Italia è ancora uno Stato di diritto e conceda l'autorizzazione a procedere, permettendo al ministro Salvini di difendersi nel processo e non dal processo, dinanzi al giudice precostituito per legge, circostanza che, come aveva egli stesso chiarito, non lo spaventa. Andiamo avanti dunque.

le domando se ci sono notizie del vice presidente Salvini. Credo sarebbe stato rispettoso nei confronti dell'Assemblea del Senato se fosse stato qua

La Presidenza sicuramente si farà latrice delle sue richieste. Intanto le chiedo di proseguire nel suo intervento. Signor Presidente, io farò il mio intervento, però ribadisco: credo che sia interesse innanzitutto della Presidenza del Senato, ma anche del Governo tutto, tutto, fare in modo che il vice presidente Salvini possa ascoltare gli interventi su un tema così delicato, in termini politici, in termini di diritti costituzionali, in termini di funzione delle istituzioni: del Governo, che fa e porta avanti la linea politica, ma anche del Parlamento, che esprime i voti rispetto a questa vicenda. *(Applausi dal Gruppo PD).* Signor Presidente, continuo il mio intervento, però le chiedo, gentilmente, ma in termini rigorosi e istituzionali, di prendere contatto con il ministro Salvini e di fare un appello accorato affinché sia presente durante il dibattito su tale questione così rilevante per il nostro Paese, per il nostro Governo, per il nostro Parlamento.

credo che riguardi tutti noi italiani. Io ho ascoltato con attenzione tutte le relazioni: le due di minoranza mi sono apparse molto più convincenti di quella di maggioranza. Così come mi sembra che il dibattito all'interno della Giunta abbia avuto i giusti toni e i giusti approfondimenti, ma che le conclusioni del presidente Gasparri non ne tengano conto. Il diritto, ma anche la logica politica e il rispetto istituzionale avrebbero dovuto portare il relatore di maggioranza a conclusioni molto diverse, rispettando, peraltro, l'iniziale volontà del vice presidente Salvini, che aveva, nell'immediatezza della vicenda, dichiarato la propria disponibilità - giustamente, dico io - a sottoporsi al giudizio che veniva richiesto. Siamo preoccupati perché la vicenda rientra in una fase politica complessa. Alcuni hanno parlato di un voto di scambio, della vicinanza tra il voto su questa questione così delicata e la richiesta di sfiducia individuale al ministro Toninelli. Sarà un caso, signor Presidente, rappresentanti del Governo, ma questa contiguità ci fa un po' Gruppo PD)*. Ne prendiamo atto, ma non è certo la nostra preoccupazione principale, perché - ahimè - siamo abituati ormai da questa maggioranza a meccanismi di *do ut des*, cioè di scambio di di nomine, poltrone e scelte politiche, tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle, anche se prendo atto che oggi la maggioranza, su una questione così politicamente rilevante, di fatto si è allargata. La preoccupazione principale, ad esempio, è il rispetto della nostra Carta costituzionale, signor Presidente. La Carta costituzionale su questa vicenda è stata sconvolta e io direi offesa più di una volta; lo è stata, ad esempio, sull'articolo 67. Protagonisti di questa offesa sono stati tutti i parlamentari del tutti i parlamentari del MoVimento 5 Stelle, perché hanno aderito a una scelta che va chiaramente contro il dettame costituzionale. «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

di votare, come prevede la Costituzione, secondo scienza e coscienza, rispettando le carte che sono state presentate alla Giunta delle elezioni ne dovrebbe pagare le conseguenze politiche. Signor Presidente, ciò è inaccettabile. Dobbiamo tutti insieme fare un ragionamento su tali questioni e difendere la Costituzione, il Senato della Repubblica e il nostro ruolo, a tutela della democrazia. Purtroppo,

ultimi mesi di Governo, da parte di questa maggioranza. Non voglio ritornare sulla tristissima vicenda dei brogli legati all'elezione

la disponibilità del patrimonio del bene più prezioso che ogni individuo ha, ossia la propria libertà individuale. Si è trattato di una vicenda che non ha precedenti in un Paese democratico.

di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

debba essere processato o no, se la magistratura abbia o no il diritto di giudicarlo, se egli abbia il dovere di affrontare un processo trasparente, chiaro e limpido di fronte agli italiani, se gli italiani abbiano o no il dovere di sapere cosa è successo in quelle ore, se la verità del Gabinetto del Ministro sia nella prima o nella seconda versione (che gli è stata fatta cambiare) se le posizioni prese dal Presidente del Consiglio e dal ministro Toninelli siano state o no frutto di forzature politiche successive. Queste sono le cose delle quali il ministro Salvini dovrebbe rispondere di fronte a un tribunale. Ha deciso di non farlo, ha deciso di ricattare la maggioranza e ha deciso di coinvolgere Forza Italia su un passaggio delicato come questo, formando - ahimè - una nuova maggioranza in Parlamento. Il Partito Democratico stasera interverrà con tutti i suoi parlamentari per dimostrare che ci vuole fermezza, trasparenza e chiarezza nei confronti del Paese. Il Governo ha il diritto e anche il dovere di portare avanti le proprie politiche, anche sull'immigrazione. Sono politiche che il Partito Democratico non condivide, ma questo diritto il Governo ce l'ha.

del nostro Parlamento e faccio un appello a tutti i colleghi, alla loro sensibilità e al loro attaccamento all'Istituzione che rappresentano. C'è tempo: ognuno guardi dentro se stesso, si prenda il tempo di guardare le carte e saprà quale decisione prendere. *(Applausi

come le è noto il Ministro ha facoltà di non essere presente. La Presidenza si fa comunque doverosamente carico di rappresentare la sua richiesta, politicamente motivata, della presenza in Aula del Ministro.

Grazie. se reputa che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico

individuare nella difesa dello Stato e nella difesa della Patria, a norma dell'articolo 52 della Costituzione, l'interesse costituzionalmente rilevante e preminente rispetto ai diritti costituzionali dei migranti e dei funzionari italiani trattenuti a bordo della è però chiarissimo che essi non costituivano in nessun caso una minaccia per la sicurezza dello Stato e dei cittadini italiani e dunque che il loro sequestro a bordo della nave militare italiana non era affatto funzionale ad ottenere questo obiettivo. Risibile poi è la controprova rappresentata dalla fuga di alcuni di loro dopo lo sbarco. Quel comportamento non è certo la prova della minaccia incombente di alcuni - forse decine? - di migranti, ma solo l'evidenza, forse, di un'inefficienza degli apparati di sicurezza che non erano stati apprestati. Vede, non sono una marziana e quindi mi è ben chiaro il contesto in cui si svolge questo dibattito quali siano gli interessi che hanno circondato e circondano questa vicenda, e che forse circonderanno anche quella in corso, di cui parlano le cronache in queste ore,

un braccio di ferro politico-diplomatico con altri Stati membri dell'Unione europea. E si è voluto semplicemente usare quelle persone e quelle di oggi come leva o capro espiatorio o scudo umano - o come lo volete chiamare per questo fine che quindi non è, signor relatore, un interesse costituzionalmente rilevante. È semplicemente in opera una ragion di Governo, che non è neppure la già discutibilissima ragion di Stato. In questo caso è proprio una semplice ragione di Governo, per cui di fatto fatto si sacrifica tutto, anche la libertà personale, non solo dei rifugiati ma anche dei funzionari della Marina militare, tenuti in ostaggio per un fine che, peraltro, non è neanche stato raggiunto. Stiamo ricominciando oggi con la nave in vista del porto di Lampedusa? Tutto questo mi porta a dire al signor Ministro - credo anche per buona educazione e per la dignità del Senato stesso - che almeno da quanto ricordo io

- qualcuno glielo dirà - a prescindere dallo stentoreo proclama di qualche giorno fa - mi processino pure - che si è tramutato velocemente in «non mi faccio processare»

che non c'è alcun motivo per cui venga utilizzato questo privilegio, questo scudo che esime un cittadino italiano in funzione governativa dalla strada dalla strada processuale che milioni di italiani, magari anche per reati minori, affrontano tutti i giorni e forse per tanti anni. Io penso che

esercizio è passato anche al Viminale e qualcuno deve avergli detto che non è possibile procedere perché non ci sono i trattati di rimpatrio, tant'è vero

gli irregolari e li stiamo aumentando, perché è una banalità che sono finiti gli sbarchi: in effetti, forse sono diminuiti da noi, ma la medaglia è che sono aumentati i detenuti rifugiati nelle carceri libiche, sia private che pubbliche, tutte persone sottoposte a stupri e torture

quindi una politica un po' più seria, un po' più ragionata, di integrazione degli irregolari che abbiamo. Smettiamola di foraggiare dittatori di tutte le stampe e risme. vada a difendersi nel processo come succede a milioni di cittadini italiani; non usi il privilegio di esserne esentato, perché questo è solo davvero un privilegio e parla qualcuno che, nella difesa dello Stato di diritto, non ha mai ceduto da nessuna parte ad alcun tipo di giustizialismo, ed è garantista per storia, cultura, per vita, per lotte, dal caso Tortora in poi. Non c'è niente di tutto questo nelle mie parole: c'è solamente il rispetto della legge e, se possibile, anche del buon senso. Grazie.

il voto che siamo chiamati a esprimere non riguarda solo la sorte del ministro Salvini e non è neanche un semplice scambio di favori e di poltrone tra Lega e MoVimento 5 Stelle: riguarda in modo molto serio e molto drammatico la tenuta delle garanzie democratiche previste dalla nostra Carta costituzionale. Non siamo infatti chiamati soltanto a decidere se negare o meno l'autorizzazione a procedere nei confronti di un Ministro. Siamo piuttosto chiamati con il nostro voto a chiarire quali siano i confini tra l'indirizzo politico e la Costituzione. La posta in gioco, dunque, è molto più alta della sorte di un singolo uomo ed è molto più alta mi permetto di ricordarlo ai senatori del MoVimento 5 Stelle - della salvaguardia degli equilibri politici all'interno dell'attuale maggioranza o forse dovrei dire alla prosecuzione del sequestro politico dei 5 Stelle da parte della Lega. Sì, cari colleghi, quello della Diciotti non è l'unico sequestro che aleggia in quest'Aula. Stiamo assistendo ancora una volta, infatti, all'inquietante metamorfosi di una forza politica che era entrata in Parlamento al grido di onestà e che ci appare, oggi, prigioniera di convenienze politiche che la spingono a rinnegare tutto ciò per cui era nata. Ma le italiane e gli italiani, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle, vi hanno eletto in Senato illusi dalla vostra falsa promessa di cambiamento e non per scardinare la democrazia costituzionale. I cittadini vedono quello che sta accadendo e sono certa che se ne ricorderanno. Il voto di oggi rappresenta un precedente pericoloso. Il rischio è dimostrare che la politica può tutto, che non esistono limiti al potere della maggioranza, che il Governo può infrangere a suo piacimento valori e principi costituzionali, perfino ponendo in essere condotte di rilevanza penale, come è avvenuto di fronte al porto di Catania; questioni di rilevanza penale, dove fatto vuol dire condotta. E le condotte del ministro Salvini sono state deplorevoli, penalmente rilevanti, in particolare una condotta che ha come elemento soggettivo del reato il voluto ritardo della comunicazione alla Diciotti del porto sicuro attrezzato per lo sbarco e l'accoglienza, come prevedono le convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese. Sta riaccadendo. Sta accadendo, in questi minuti, in queste ore, un fatto analogo, a Lampedusa.

rimpalli di responsabilità e, addirittura, la minaccia di far arrestare chi ha rispettato solo la legge del mare, che impone di accogliere a bordo passeggeri di imbarcazioni in difficoltà, trasbordandoli nel più vicino porto sicuro. La posta in gioco in questo nostro voto, colleghi, è l'individuazione dei confini dell'azione di Governo, del punto fino a dove la politica può spingersi per perseguire i propri fini. Questi confini devono essere dettati dai parametri di ragionevolezza e congruità dell'atto e dalla reale difesa della sicurezza nazionale; elementi tutti mancanti tutti mancanti nella condotta del Ministro dell'interno; una condotta dettata solo da motivazione e conseguente vantaggio politico: una condotta illecita, perpetrata da un Ministro in perenne campagna elettorale e ripeto in perenne campagna elettorale! L'articolo 96 della Costituzione e la legge costituzionale n. 1 del 1989 sono molto chiari su questo: la deroga alla giurisdizione è eccezionale e l'immunità del Ministro è guardata con disfavore. Tant'è che il voto parlamentare può solo intervenire per ostacolare il normale *iter* di giudizio sulla condotta del Ministro da parte del giudice. Come sottolineato da Leopoldo Elia - voglio citare il grande professore Elia - proprio in quest'Aula il 27 gennaio del 1988, quella riforma fu il frutto di una spinta egualitaria, che Elia stesso fece risalire addirittura al grande Tocqueville. Come ogni altro cittadino, il Ministro è soggetto alla giurisdizione e solo in casi eccezionali l'autorizzazione a proseguire il procedimento penale può essere negata; casi eccezionali, che nulla hanno a che vedere con il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. Come disse sempre Leopoldo Elia, quella delle Camere è una valutazione non sull'operato del Ministro, del Ministro, ma sulla sussistenza degli straordinari presupposti che escludono l'ordinaria competenza della magistratura. Su questo vi voglio sentire: voglio sentire gli interventi dei colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega su questo rapporto tra ordinario e straordinario. Questi presupposti - noi lo sappiamo - sono la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo: non l'interesse elettorale della Lega e del suo capo Salvini. In entrambi i casi è la Costituzione, non la politica, che deve guidare la nostra valutazione. L'interesse dello Stato deve essere costituzionalmente rilevante e il perseguimento dell'interesse pubblico deve avvenire nell'esercizio di una funzione di Governo, funzione di Governo che è *ab origine* contenuta nei limiti che la stessa Costituzione ci pone. Diceva bene, di nuovo, Leopoldo Elia: a guidare la valutazione delle Camere deve essere non la ragion di Stato, ma la ragion di Costituzione e in questo caso non è così. Dobbiamo guardarci, colleghe e colleghi, dalla tentazione di interpretare da un punto di vista di partito interessi che invece sono collettivi, che sono dello Stato, che questo Parlamento dovrebbe rappresentare, perché con il nostro voto rischiamo di mettere in discussione i fondamenti etici della democrazia; ragion di Costituzione, quindi, e non realizzazione di promesse elettorali, come invece il ministro Salvini addirittura ha rivendicato, cercando di giustificare l'opacità e la gravità del suo operato; ragion di Costituzione che - come ribadì alla Camera un altro grande del nostro diritto costituzionale, Gianni Ferrara - si identifica anche - e io dico soprattutto - con la protezione della dignità umana e dei diritti fondamentali. Quella dignità e quei diritti sono stati negati da Salvini non solo all'equipaggio della Diciotti - tutti militari e marinai italiani - ma anche a quelle 177 persone disperate, fiaccate da giorni e giorni in mare, trattate come rifiuti da respingere, da un comportamento politico indegno di un Ministro della Repubblica e mi spingo a dire con grande rispetto, non equivocate come al solito - indegno di un uomo politico credente, che addirittura ha più volte sventolato nei suoi comizi il Vangelo e il Rosario. Ma forse, per per i nostri sovranisti, la solidarietà è solo a senso unico, vale solo tra di loro, bianchi, cattolici, meglio se sposati e certamente eterosessuali. Oggi siamo tutti chiamati - o forse voi siete chiamati perché noi non abbiamo mai avuto dubbi dal primo giorno non abbiamo mai avuto dubbi dal primo giorno - a scegliere tra politica e Costituzione, tra gli interessi di una maggioranza politica e la tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Carta. Un precedente di questo genere domani legittimerebbe, infatti, violazioni sempre più gravi dei diritti e della dignità delle persone, perché sarebbe infinitamente più semplice giustificarli di nuovo. Affermare che l'esercizio della funzione di Governo può spingersi fino ad infrangere impunemente - perché voi lo salverete dal processo - la legalità penale significa rinnegare secoli di costituzionalismo; significa colpire a morte la nostra Carta repubblicana. Non stupisce che un atto così grave provenga da una maggioranza che si autodefinisce populista e sovranista. Fin dal primo giorno del suo mandato, il Governo ha dato larga dimostrazione di non possedere una cultura delle garanzie costituzionali. Come dimenticare che il presidente Conte ha avuto il coraggio di dire di fronte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che la nostra Costituzione è sovranista e populista, perché l'articolo 1 afferma che: «La sovranità appartiene al popolo». Ci sarebbe da ridere, ma a me viene da piangere. Come dimenticare tutte le volte in cui abbiamo ascoltato da Salvini e da altri esponenti del Governo che tutto è concesso a chi ha dalla sua parte 60 milioni di italiani. Non è così, non è così. Lo dico al presidente Conte, perché l'articolo 1 non finisce a quella frase, e lui da giurista lo dovrebbe sapere. L'articolo 1 dice che la sovranità che la sovranità appartiene al popolo, ed è vero, ma anche che il popolo: «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», quei limiti che voi violerete con questo voto. Non è così. Lo dico all'assente, al latitante, all'impaurito e fugace ministro Salvini: non avete e non avrete mai il consenso del 99 per cento degli italiani

maggioranza, ma è governo della maggioranza nei limiti della Costituzione, che limita l'esercizio del potere per garantire i soggetti più deboli e le minoranze politiche rispetto all'arbitrio.

La proposta del relatore Gasparri, dal punto di vista giuridico, è a mio avviso ineccepibile e possiamo riassumerla Il delitto di cui è stato accusato il Ministro dell'interno è grave (sequestro di persona aggravata, *ex* articolo 605 del codice penale).

espresso in Senato dal presidente Conte e anche nei contatti con l'Europa, è stato chiaro: il Governo ha previsto una diversa regolamentazione e gestione dei flussi migratori; la responsabilità è comune con l'Europa, chi sbarca in Italia sbarca in Europa; vi è una redistribuzione dei costi e dei migranti. Pertanto, peraltro e comunque, si è trattato dell'atto di tutto un Governo

Credo tuttavia - e tornerò tra poco sui motivi strettamente giuridici - che, sotto sotto, questo dibattito riguardi altri aspetti, secondo quanto ho sentito dagli interventi dei colleghi. In realtà, si torna a parlare del tema dell'immigrazione, che abbiamo trattato diverse volte in quest'Aula, evidentemente con visioni politiche molto diverse, che corrispondono a visioni storiche, intellettuali e anche religiose in senso lato,

Il tema dell'immigrazione, come altri temi caldi al momento, genera normalmente discussioni e divisioni molto profonde e dibattiti in cui sono presenti anche dosi di cattiveria, cinismo e violenza verbale esagerata.

Penso, però, che ognuno abbia diritto di fare i propri congressi e quel popolo farà il suo, perché là si discute di *gender*, di utero in affitto e di altre cose molto gravi che avranno conseguenze future deleterie, perché sono contro natura. «Dio, patria e famiglia» è un motto di vita per la maggioranza degli italiani e non quell'altra cosa che abbiamo visto scritta su cartelli che sono Tutto ciò avviene per colpa del relativismo e del nichilismo imperante. Io sono un ammiratore della *lectio magistralis* di Ratisbona di Benedetto XVI. il relativismo e, sopratutto, con il nichilismo tutto può essere vero e ognuno può fare ciò che vuole e ciò distrugge la possibilità delle Nazioni occidentali di sopravvivere come comunità e civiltà negandone le regole, la storia e la verità. i fatti della Diciotti, 177 migranti sarebbero rimasti cinque giorni in più ancorati nel porto di Catania, nave c'erano anche l'equipaggio, i viveri e i medicinali. È possibile che le donne e i bambini che arrivano siano sempre tutti malati? Gli uomini no? C'erano i servizi a bordo? Erano in numero esatto? Quelle persone a casa loro avevano i servizi? Prima di venire a esprimere un tale parere, nei giorni scorsi peregrinando nel mio collegio di Cuneo, nella città di Alba, che frequento di più, e nel mio paese che si chiama Priocca, ho chiesto alle persone che ho incontrato cosa devo votare e come devo comportarmi. Sono paesi dove ci sono una tradizione cristiana, il senso del dovere e l'amore per il lavoro. Faccio una sintesi, traducendo dal dialetto piemontese quanto ho sentito affermare perché, se dicessi tutto, verrebbe giù il soffitto di questa Aula. ed è ora di cambiare; la politica lo deve capire e deve decidere a tutela dei cittadini più deboli, che pagano di più la diminuzione dei fondi e del sistema dello Stato sociale e condividono con masse più numerose sempre lo stesso tesoretto; devono dividere gli spazi, il lavoro, anche in nero, con mucchi di persone che arrivano qui, sostano in posti non congrui e si comportano in modo non corretto. Non sono tutti, ma la percentuale è molto alta. Non abitano in centro gli italiani deboli, non hanno delle professioni intellettuali e qualcuno li deve difendere e stranamente la difesa viene dal centrodestra.

Se agiamo così, secondo il piano Sophia si devono accomodare tutti: i migranti perseguiti, quelli economici, i terroristi per dare possibilità di lavoro e lucro alle ONG, alle cooperative, agli imprenditori italiani senza scrupoli. Questa è la verità che ho il coraggio di dire. Ma questo è lavoro? Qualcuno dice che lo è. È un *business* sporco, inutile e dannoso a carico dei contribuenti e per gli interessi di pochi e per futuri eventuali voti. Nel

un calo drastico impressionante del 90 per cento - e, quindi, meno morti. Sono iniziate le espulsioni in numero significativo. Sono stati sgomberati dei campi che sono strutture di violenza e di sporcizia di ogni genere. Tornando alle motivazioni giuridiche, per decidere su questa problematica bisogna parlare della divisione dei poteri. La magistratura è un ordine che esercita un potere giudiziario autonomo e indipendente ai sensi degli articoli 106 e 107 della Costituzione - la citiamo anche noi - garantito dalle nomine per concorso e dalla inamovibilità. Questa è la tutela della magistratura, ma il potere esecutivo come opera? Opera secondo discrezionalità. Allora è l'interpretazione della discrezionalità che fa la differenza. Cos'è la discrezionalità dell'azione politica? Prima di decidere il Governo deve chiedere alla magistratura? Quali sono gli interessi superiori che devono tutelare gli italiani? Sennonché è successo questo: la politica negli ultimi anni - lo riconoscono studiosi seri

Ha deciso di non decidere; ha ristretto i suoi confini a favore degli altri poteri o ordini (magistratura, burocrazia, tecnocrazia) che, per un principio fisico, hanno occupato quegli spazi. Oggi l'opinione pubblica vuole una politica che decida, che governi, che non deleghi, e la giudicano in tempo reale su questi aspetti. Se la politica non è in grado di fare questo, non vuole, non è capace, chi difende gli interessi nazionali? Ma allora qualcuno dice: tanto vale abolire la politica; decidano le corti nazionali e internazionali. Poiché non è così, riprenda la politica - in questo caso attraverso il voto del Senato - le proprie prerogative a favore di un modo di operare che tuteli i cittadini, tuteli gli italiani. Forza Italia è garantista sempre e si comporterà di conseguenza, con queste ed altre motivazioni che saranno espresse dai miei colleghi. Avrei detto: ministro Salvini, tenga duro sulla nave Mare Jonio, ma forse è andata diversamente; non ne conosco le ragioni, doveva andare così.

che, per abuso di potere, con l'aggravante di essere un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ha privato della libertà 177 persone, alcuni minori tra l'altro, e violato deliberatamente le norme nazionali e convenzioni internazionali. Non era mai accaduto nella storia della nostra Repubblica che un Ministro dell'interno e la sua maggioranza che lo sostiene chiedessero di negare l'autorizzazione a procedere in nome di un supposto e preminente interesse pubblico, negandosi così a un principio di responsabilità e al principio di legalità, principi cardine dello Stato costituzionale di diritto. Il voto di oggi ha dunque solo per oggetto una vicenda giudiziaria, che che è anche rilevante, ma anche una visione dello Stato, del nostro Paese, dell'Italia. L'obbligo di salvare una vita umana in mare - lo ricordo - è un preciso dovere che grava su ogni Stato e su qualsiasi altra norma. L'Italia ha aderito alle convenzioni internazionali che regolano la materia, le quali, oltre a discendere dal diritto pubblico internazionale consuetudinario, costituiscono un limite insormontabile per il legislatore statale che, nel rispetto degli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione, non può derogarvi poiché esse entrano nell'ordinamento attraverso norme costituzionali, e assumono quindi rango gerarchico superiore alla legge ordinaria. Questo è successo. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, poi, stabilisce che ogni Stato aderente deve esigere che il comandante di una nave autorizzata a battere la sua bandiera, sia essa dello Stato o privata, presti soccorso a chiunque in mare sia in pericolo. Ebbene, oggi, in nome di una supposta superiorità dell'interesse pubblico, tutto questo è venuto meno; è venuto meno tutto quanto è stato costruito in tutti questi anni per la credibilità del nostro Paese. Tutti ci riconoscono quanto noi diamo aiuto anche nelle missioni internazionali. Eppure, oggi è venuto meno tutto questo, e per salvare che cosa?

Se si volevano cambiare le regole dell'immigrazione, lo si doveva fare là dove era giusto farlo e dove era giusto intervenire. Negli organismi europei c'era la Commissione per cambiare il Regolamento di Dublino; peccato che non c'era mai l'attuale Ministro dell'interno, che era sempre in giro a fare politica. *(Applausi dal È stato il più assenteista. Ci sono state venti Commissioni per disciplinare il Regolamento di Dublino, ma non era mai presente qualcuno della Lega: lo hanno detto i nostri europarlamentari. È lì che si dovevano di fatto regolare le cose, non come si sta facendo adesso. È successo che il nostro Paese sta rimanendo isolato da tutto. Non siamo stati

di criterio e non ho capito perché mostriate una disumanità di questo genere, con i «me ne frego» e con la voglia di andare avanti, tanto non ve ne importa niente. Non si pensa che la vita è il valore più prezioso per ogni persona; persona: anch'io lo voglio dire, perché davvero le persone hanno la loro importanza, qualsiasi colore abbiano.

Non è individuando tutti i giorni un nemico che si possono vincere le elezioni. Prima o poi verrete anche voi alla resa dei conti. Non è così che si fa e comunque le proteste degli ultimi giorni - lo ricordo - come la grande manifestazione del 2 marzo a Milano sono state una grande risposta a tutto quello che sta succedendo e a tutte le azioni che sta facendo

Purtroppo per la sopravvivenza di questo Governo, il Ministro, se aveva coraggio, doveva difendersi nel processo e non dal processo. Il nostro è ancora uno Stato di diritto, come hanno ben detto prima i miei colleghi. Come tutti i cittadini, si sarebbe dovuto sottoporre alla giustizia e difendersi, come era giusto che facesse se pensava

insieme a me e alla senatrice Tesei, in Giunta hanno approfondito la vicenda, studiando nel dettaglio le carte che vengono portate oggi in Aula. Non dobbiamo e non vogliamo entrare nel merito della vicenda, perché non spetta a noi farlo. Non spetta a quest'Assemblea giudicare nessuno. Noi ci dobbiamo limitare ad alcune valutazioni di carattere strettamente giuridico previste dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Sostanzialmente dobbiamo dare risposta a tre domande molto semplici. La prima: il ministro Salvini era o non era nell'esercizio delle sue funzioni di Governo quando ha portato le condotte oggi sotto l'esame di quest'Assemblea? La risposta è pacifica: certamente sì, stava comportandosi da Ministro, stava nell'esercizio delle sue funzioni di Ministro e addirittura era nell'ambito di una decisione assunta da parte dell'intero Governo, come ci è stato confermato più e più volte dalle dichiarazioni del presidente Conte in questa stessa Aula, anche prima che uscisse la notizia che il ministro Salvini era indagato. Quindi, siamo pacificamente nell'alveo di una condotta ministeriale. Dobbiamo rispondere poi ad altre due domande, se cioè il ministro Salvini, nelle sue condotte, abbia tutelato o meno l'interesse dello Stato costituzionalmente garantito ovvero se abbia tutelato un interesse pubblico. Queste sono le domande alle quali dobbiamo dare risposta. Quanto alla seconda e alla terza domanda, dobbiamo forse, per dare una risposta compiuta, fare una valutazione che sia di merito limitatamente, come ho detto, a queste domande, e poi di metodo. La prima valutazione di merito: esiste ed è un'affermazione la mia - una normativa di rango costituzionale (articolo 52 della nostra Costituzione) e esiste anche una normativa legata alla legge ordinaria all'articolo 4, comma 3 del testo unico sull'immigrazione, che regolamenta l'ingresso nel nostro Paese di cittadini di altri Stati. Non è infatti possibile per uno Stato di diritto consentire l'accesso indiscriminato nel proprio territorio di cittadini che provengono da altri Stati. Questo è pacifico ed è dunque pacifico che chiunque, a partire dal Ministro dell'interno fino all'ultimo dei pubblici ufficiali in servizio nel nostro Paese, abbia un preciso non solo diritto, ma direi dovere di applicare la legge e di pretendere il rispetto delle disposizioni normative che prevedono che l'ingresso nel nostro Paese debba avvenire in determinate circostanze e secondo determinati presupposti. Nel merito, quindi, c'era sicuramente un interesse, che è da valutarsi come pubblico, anzi vorrei dire un dovere che il Ministro aveva di escludere dall'accesso nel nostro Paese cittadini stranieri che non avevano il diritto di entrarvi. Nel metodo, Nel metodo, dobbiamo però anche valutare se questa esclusione sia stata bilanciata dalle circostanze mi porta a denunciare un equivoco che per anni è stato artatamente diffuso, perché amici e colleghi, è giuridicamente molto diverso il concetto di salvataggio in mare da quello di asilo perenne nel nostro Paese, perpetuo e indiscriminato. Se io incontro un ferito per strada, ho l'obbligo giuridico di soccorrerlo, non di adottarlo. Su questa confusione di concetti si è inserita l'opera dei trafficanti di esseri umani, che hanno negli anni costruito un sistema ben collaudato che costringeva il nostro Paese a equivocare tra questi due concetti e quindi ad accogliere indiscriminatamente persone. Qual era questo sistema? Mi piacerebbe che ciascuno di voi avesse avuto l'opportunità di leggere quei quattro faldoni di carte, perché da quei quattro faldoni emerge con chiarezza questo sistema collaudato, che ora finalmente è stato disarticolato, per cui queste persone venivano caricate su barconi malsicuri che nessuna autorità preposta al controllo della navigazione mai autorizzerebbe all'uso in mare, venivano portate in mezzo al Mediterraneo con una rotta precisa su Malta, venivano accolte davanti alle acque maltesi da due motovedette e un aereo della Guardia costiera, che si premurava di dare loro la nuova rotta verso Lampedusa (era una rotta precisa al millimetro, al grado nautico) e quando si arrivava in prossimità delle acque territoriali, questi barconi immediatamente toglievano il tappo e dichiaravano l'emergenza così da poter essere soccorsi. Con l'emergenza, poi, venivano fatti sbarcare e non appena fatti sbarcare ovviamente queste persone si dileguavano. Questo tipo di operazione costringeva lo Stato italiano ad essere con le spalle al muro, cioè a scegliere tra il naufragio e la perdita di vite umane in mare e l'accesso indiscriminato nel nostro Paese. Questo sistema è stato disarticolato da una precisa politica che, senza fare un solo morto, anzi salvando vite umane - sto parlando della decisione che è stata assunta dal Ministro - ha permesso di distinguere le due fasi e questo non perché ci sia una volontà politica di chissà quale caratura, ma semplicemente perché sono le stesse Convenzioni internazionali che ho sentito citare in quest'Aula a sostegno della tesi di chi vorrebbe il ministro Salvini a processo, che dichiarano espressamente quando le Convenzioni SAR e SOLAS non si applicano. Leggo il testo perché dobbiamo rimanere in un ambito strettamente giuridico: «Le «Le questioni diverse dal salvataggio relative a richiedenti asilo, a rifugiati e allo stato di migranti sono oltre il mandato delle Convenzioni internazionali e oltre le finalità delle Convenzioni SOLAS e SAR».

non significa neppure porto sicuro; significa posto in cui le persone sono in sicurezza.

può essere o la terra o anche a bordo di una unità di salvataggio, quale era esattamente la nave Diciotti. Leggo: *may be aboard a rescue unit*. I migranti I migranti che, loro malgrado, si trovavano a bordo della nave Diciotti già si trovavano al sicuro e la loro vita è stata soccorsa, è stata messa in sicurezza, sono state garantite loro cure mediche, assistenza psicologica, c'erano a bordo mediatori culturali e sono stati rifocillati e seguiti in tutto. Quindi, da una parte abbiamo l'interesse giuridico che lo Stato italiano ha di permettere che nel Paese entrino solo persone che lo possono fare, e questo, perdonatemi, ma credo che tutti noi dobbiamo convenire che è certamente un interesse pubblico; dall'altra parte, non possiamo permetterci di perdere vite in mare. Ma la domanda è: si perdono più vite in mare autorizzando e chiudendo gli occhi su queste modalità antiumane, utilizzate per anni dai trafficanti di esseri umani che, contando sull'emergenza, cercavano in quel modo di far sbarcare il loro carico pagante, anche a prezzo di persone che sono affondate nel Mediterraneo, oppure paga di più, proprio in termini di salvaguardia della dignità della della dignità della persona e delle vite umane, il fatto di mettere in chiaro fin da subito che noi soccorreremo chiunque (a differenza di quello che fa Malta) e non accompagneremo nessuno in acque territoriali di chicchessia senza avere prima garantito la vita e la sicurezza? *(Applausi dai

il fascicolo è disseminato di atti formali del nostro Governo, che hanno cercato - affannosamente, direi di affrontare la crisi. C'è una lettera del presidente del consiglio Conte datata 14 luglio, che mette in allarme l'Europa sostenendo l'impossibilità per l'Italia di continuare ad accettare questo traffico di migranti; c'è una nota a verbale del 19 agosto che, proprio in relazione alla nave Diciotti, chiede che l'Europa sia coinvolta nella vicenda e che si dia luogo alla redistribuzione dei migranti; c'è una lettera del Ministero degli esteri del 21 agosto, che chiede nuovamente una riunione; c'è una riunione riunione preparatoria del 23 agosto, sempre del Ministero degli esteri; c'è una riunione per il ricollocamento del 24 agosto, il giorno prima dello sbarco. Tutto questo nel più totale naufragio - questo sì di un'Europa che è scomparsa dall'orizzonte, lasciando sola l'Italia, salvo poi - le chiedo ancora un minuto, Presidente, perché

«Siamo stati molto chiari nei mesi scorsi nel sottolineare che naturalmente, quando serve, la detenzione può essere utilizzata per facilitare l'identificazione dei migranti e per impedire che svaniscano anche durante le procedure di asilo. Abbiamo chiesto a tutti gli Stati membri, inclusa l'Italia, di fornire allo scopo centri di accoglienza adeguati,

Questa è la situazione davanti alla quale il ministro Salvini si è trovato ad agire. Io sono persuaso - e credo di averlo ampiamente dimostrato - che il compito del Ministro fosse esattamente quello che è stato portato avanti: nel preminente interesse pubblico e nell'esercizio delle funzioni di Governo, garantire il rispetto dell'articolo 4, comma 3, del testo unico dell'immigrazione e garantire il rispetto di una linea politica concordata col Governo, decisa con gli italiani, votata dagli italiani, stabilita dagli italiani come linea per affrontare le questioni della immigrazione.

Viene da chiedersi come mai non siano qua altri Ministri di Governi precedenti che, viceversa, hanno di fatto disapplicato il testo unico sull'immigrazione e consentito quella deportazione di massa che forse poteva essere evitata già qualche anno fa, come abbiamo dimostrato essere possibile oggi. Forse, sotto processo dovrebbero andarci loro.

un voto che non riguarda solo il destino giudiziario del singolo Ministro, ma che attiene allo stesso ordinamento giuridico del Paese. votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini significa di fatto affermare: sì, in Italia oggi esiste qualcuno che può infischiarsene della legge e questo qualcuno siede tra le fila del Governo. Quello di domani sarà un voto spartiacque, che rischia di segnare il passaggio tra l'essere uno Stato di diritto, nel quale tutti

Colleghi la discussione sta proseguendo. Chi vuole lasciare l'Aula lo faccia, per cortesia, in silenzio. Prego anche i colleghi di allontanarsi dal banco del Governo, anche se tutti noi esprimiamo solidarietà al sottosegretario Candiani. nel quale tutti siamo chiamati a rispettare la legge, o se invece vogliamo diventare un Paese nel quale qualcuno si ritiene autorizzato a violare le leggi, magari adducendo il fatto di essere legittimato dal voto popolare. motivo, signor Presidente, mi unisco ai colleghi del mio Gruppo che mi hanno preceduto e ai relatori di minoranza per chiedere in modo chiaro e netto che il ministro Salvini non si faccia inopportunamente scudo con l'immunità parlamentare

il ministro Salvini viene chiamato in causa dal tribunale dei Ministri di Catania, che è l'organo costituzionalmente preposto a vigilare su eventuali reati commessi dal Governo. La richiesta che abbiamo ricevuto è espressione di quel sistema di pesi e contrappesi di cui il nostro Paese si è dotato costituzionalmente, proprio a garanzia dell'esercizio democratico dei poteri, perché nessuno è tenuto ad abusare del proprio ruolo, neppure il Governo e men che meno un singolo Ministro. Dunque, non si tratta di un cruccio o uno schiribizzo dell'uno o dell'altro magistrato. Il tribunale di Catania non sta facendo altro che il proprio dovere:

nostro dovere, onorevoli colleghi, fare sì che questo processo si tenga. È esattamente dovere dell'Assemblea fare sì che se il ministro Salvini sia innocente o meno venga stabilito nella sede opportuna, che è quella del processo. Tra l'altro, l'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento potrebbe essere eventualmente negata soltanto nel caso in cui il Ministro avesse agito per per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, oppure per il perseguimento di un preminente interesse pubblico, cosa che il Ministro, all'interno della memoria

un'altra. Qui c'è la consapevolezza nei colleghi di maggioranza e purtroppo anche in quelli di Forza Italia e di altre forze politiche, che si affiancano alla Lega e al MoVimento 5 Stelle, che se

i colleghi che adesso sostengono di non voler concedere l'autorizzazione a procedere andrebbero semplicemente a casa, ci sarebbe la caduta del Governo e la legislatura sarebbe finita.

chi si nasconde dietro l'immunità parlamentare sono le stesse forze politiche che per anni hanno demonizzato l'immunità parlamentare, ne hanno teorizzato addirittura l'eliminazione

si tenga. All'improvviso, quelle stesse forze politiche che per anni hanno negato e demonizzato l'immunità parlamentare, adesso smentiscono *in toto* quelle loro dichiarazioni. Questo perché, come dicevo prima, è lapalissiano che rispetto ad una condanna il Governo cadrebbe. La cosa è ancora più imbarazzante per i colleghi dei 5 Stelle, signor Presidente, perché non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia.

consultazione del tutto nebulosa su una piattaforma non trasparente, una vera e propria messa in scena costruita ad arte per creare un capro espiatorio a cui attribuire la responsabilità di essere dei voltagabbana;

perché nel frattempo, per mero interesse, si piegano a qualsiasi disonestà; inoltre, proprio quelli che dicevano di voler aprire il Parlamento come se fosse una scatoletta di tonno, adesso si sono piegati e stanno diventando i lustrascarpe dei loro alleati di Governo PD)*. Onorevoli colleghi, noi oggi votiamo per decidere quale Paese vogliamo essere e anche quale Paese non vogliamo diventare. Quanto è avvenuto con il caso Diciotti ha offerto uno spettacolo indegno del nostro Paese agli occhi del mondo. la maggioranza non vuole ritornare sulla propria scelta, ma vuole evidentemente difendere il ministro Salvini dal processo e non nel processo e si spinge addirittura alle minacce. Ci sono forze politiche che si spingono a minacciare i loro componenti se non si atterranno a questo pseudovoto espresso appunto dalla piattaforma Rousseau. Rousseau. Questo è molto grave. Come diceva il relatore De Falco, è grave quanto viene fatto nei confronti dei colleghi. Io mi auguro che ci si possa ancora ripensare e faccio anch'io appello, come il nostro presidente Marcucci, affinché alcuni colleghi riconsiderino la loro decisione.

pretenderà di trincerarlo dietro l'immunità parlamentare, vorrà dire avallare il principio secondo cui il potente di turno riterrà di poter fare quello che vuole e questa è una grave lesione per il nostro Paese e per la democrazia. Io mi auguro che questo non succeda, ma se così dovesse accadere sarebbe davvero molto grave. *(Applausi

proverò allo stesso tempo a seguire la traccia che il presidente Gasparri e prima di lui la Corte costituzionale dal 2012 a qualche mese fa hanno suggerito: pedissequamente sul tema, non divagare sulla politica dei migranti, Salvini qui, il Ministro di là, il presidente Conte da un'altra parte ancora. Il tema è stato sviscerato da più parti, ma la domanda segue soprattutto una risposta al contenuto della legge costituzionale n. 1 del 1989. È lì il punto e lì casca l'asino. È già stata rappresentata doppiamente una visione naturalmente antitetica, tanto che abbiamo due relazioni di minoranza ed una relazione di maggioranza, circa la valutazione sull'interesse pubblico preminente e naturalmente l'atto costituzionalmente rilevante. Se stiamo a quanto abbiamo letto, la mia opinione naturalmente è che vi siano fondatissimi elementi per ritenere le due relazioni di minoranza assolutamente ottime nel supportare la tesi che l'autorizzazione a procedere che riguarda il Vice Presidente del Consiglio possa essere legittimamente e coerentemente conferita e concessa. Il punto debole della difesa del ministro Salvini, che in maniera precisa ha ripetuto più volte nel tempo, è il seguente: Salvini sostiene che la scelta fatta in attuazione dell'indirizzo politico costituisca di per sé espressione di un interesse pubblico a tutela della sicurezza nazionale. Non esiste memoria di una considerazione di questa natura: non soltanto non esiste memoria, com'è evidente, nelle relazioni di minoranza, ma trovo molto debole anche la memoria in in opposto presente all'interno della relazione del presidente Gasparri e questo perché non sta scritto da nessuna parte che la motivazione politica assuma un rilievo nella legge costituzionale n. 1 del 1989. Quel che è certo, invece, ed è assolutamente inequivocabile, è che le garanzie costituzionali proteggono le libertà e l'incolumità delle persone contro gli abusi dei Governi. La volontà politica, né in questo momento, né in altro, può entrare in contrasto con la Carta e con i trattati internazionali e l'indirizzo politico - è evidente - deve sottostare al principio di legalità, avendo nella Carta e nel rispetto dei diritti inviolabili il suo naturale contrappeso. Chi ha citato l'*habeas corpus* lo ha fatto legittimamente, richiamando la madre di una storia del diritto che nel tempo, nei secoli, noi abbiamo fatto vostra, a partire dagli Statuti comunali di molte città italiane nel periodo medievale. però un punto politico che supporta, anzi, doveva necessariamente supportare la tesi prevista nella relazione di maggioranza ed è la giustificazione del comportamento di una parte della maggioranza, quella che fa capo al MoVimento 5 Stelle, che ruotava completamente non rispetto alla posizione tenuta nella legislatura precedente, a quella prevista nell'atto fondativo del MoVimento 5 Stelle. Non che io lo condivida, ma non c'è dubbio che nell'atto fondativo stia l'anima del MoVimento 5 Stelle, obbligato a ruotare per difendere il Vice Presidente del Consiglio. Per questo c'era bisogno, citando e organizzando una certa interpretazione del diritto, di argomenti plausibili, a cominciare dall'invenzione letterale della responsabilità collegiale.

rispetto alla posizione assunta dal vice presidente del Consiglio Matteo Salvini. Quindi non capisco la differenza tra il cinguettio del ministro Toninelli o del vice presidente Di Maio, che ho mandato a memoria, e riunioni su riunioni o esternazioni su esternazioni, con nessuna delle due posizioni supportata, però, da un atto amministrativo, da un provvedimento collegiale tale da far ritenere l'atto sconsiderato di un Ministro come l'atto di un intero Governo. Quell'atto non esiste; se c'è, bisogna che venga tirato fuori.

È un fatto che siano state rovesciate due posizioni: quella del ministro Salvini, prima propenso a farsi giudicare e, successivamente, con evidente esempio di camaleontismo, propenso, invece, a farsi proteggere dall'Assemblea. Il punto vero, però, è l'aver rinnegato, da parte del MoVimento 5 Stelle, una parte consistente della loro anima circa il giudizio sulle immunità. Ho anche io una sfilza di citazione possibili se mi vengono richieste, le consegno agli atti per ragioni di tempo. Opporsi all'autorizzazione a procedere è un ribaltamento secco della posizione da voi tenuta nel corso degli anni. stato detto, lo ha fatto anche il presidente Conte, in questo caso in veste di giurista, e ne sono preoccupato, che «chi tira in ballo le immunità non sa di cosa parla». sapeva di cosa parlava un suo maestro. E poiché la generazione mia e del presidente Conte è la stessa, noi ci siamo formati, pure se in facoltà diverse, sullo stesso testo, che è quello di Costantino Mortati. Costantino Mortati inseriva nell'articolo 96 della Carta tutto ciò che attiene alla giustizia politica. Ed è l'articolo 96 della

Il caso che esaminiamo oggi, signor Presidente, è un modello classico studiato dalla scienza della politica. È il problema che si pone ai movimenti populisti quando vanno al Governo. una cosa è promuovere campagne elettorali permanenti sulla base di *slogan* ad effetto, altra cosa è assumere responsabilità istituzionali e, per farlo, muoversi dentro la cornice costituzionale. Può accadere, come in questo caso, che si sia travolti anche da un corto circuito; che comportamenti di quando si è all'opposizione vengano rinnegati una volta al Governo; che l'onorevole Di Maio debba esibirsi in acrobazie da funambolo. Certo che può accadere. Tuttavia, se si rinuncia ai principi fondanti della propria storia, se si contravviene a uno degli ideali bandiera, la storia si vendica sempre. E, prima della storia, si vendicano, decisamente, gli elettori. Oggi dobbiamo registrare, comunque, un fatto nuovo. In questo Parlamento seggono due tipi di maggioranza diversa: una maggioranza larga, fondata sull'articolo 96 della Costituzione, ed una maggioranza, invece, fondata sull'articolo 94 94 della Costituzione. Ho concluso. Ho letto più volte le carte, per chiedermi se il mio garantismo entrasse in conflitto con il voto a favore sulla concessione dell'autorizzazione a procedere. La risposta è stata non facile, ma è stata che non c'è conflitto. E non c'è conflitto perché le libertà individuali, l'incolumità delle persone, i diritti fondamentali prevengono, cioè vengono prima. Inoltre, poiché questo è un tempo dove dilaga il diciannovismo, non possiamo, quando dilaga il diciannovismo, fare dei diritti civili carne di porco. Non si può tentennare. Anzi, sono sorpreso che l'anima liberale di Forza Italia non si sia ribellata. Mi rivolgo al senatore Perosino, che ha citato il Papa Ratzinger di Ratisbona e il dialogo tra Manuele II Paleologo e il dotto persiano. Suggerisco, invece, al senatore Perosino di leggere Papa Wojtyla che accettò, come evoluzione della scienza e dei diritti, tale Darwin e il darwinismo, che Papa Ratzinger, naturalmente, a Ratisbona smentì e dimenticò.

«Per l'ennesima volta, sulla Diciotti andrò a testa alta in Senato. Facciano come credono. Se mi processano, sarò orgoglioso». La stessa ostentazione di forza è stata replicata più e più volte in questi mesi, accortamente orchestrata da un gruppo di comunicazione che il Ministro, orgogliosamente, definisce la bestia. Il quesito della procura di Catania - di questo oggi discutiamo - è semplice: su quanto avvenuto nell'agosto scorso al largo delle nostre coste, ci sono o no gli estremi per un reato che nulla ha a che fare con la sicurezza nazionale, compiuto con totale spregio di qualsiasi prassi istituzionale e senza alcuna collegialità, come dimostrano i documenti analizzati dalla Giunta per l'autorizzazione a procedere? Ministro - che non c'è - lei ha deciso sì o no di tenere in ostaggio 177 persone, immigrati, sì, persone? E ciò per un calcolo che non riguarda per niente la sicurezza nazionale ma le sue fortune politiche. È una modalità da allora divenuta prassi, dovrei dire aberrante, di questo Governo: orchestrare ad arte su qualsiasi questione seria solo dei can-can mediatici, sottraendo alla politica e alle aule parlamentari il proprio ruolo, facendo divenire qualsiasi tema esclusivo oggetto di contrattazione e compravendita ad uso e consumo dei due contraenti di Governo. Il volgare scambio è: no processo a Salvini, no sfiducia a Toninelli. Caro Ministro che non c'è, lei probabilmente a processo non ci andrà e non perché quello che ha fatto coincida con l'interesse supremo nazionale. Lei non ci andrà perché ha fatto di tutto per non andarci, perché i suoi alleati di Governo, un tempo campioni di giustizialismo, sono divenuti felicemente suoi complici. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Mentre ancora fingono, da anime belle, di essere diversi in un vergognoso gioco delle parti, non possono smentirla se non smentendo se stessi e questo Governo. La salveranno dal processo ma non dal giudizio politico, un giudizio per noi indiscutibile. Dobbiamo ricordarle quanto affermato in diretta Facebook il 24 gennaio commentando la richiesta dei giudici; quello che ripeteva il 27 gennaio il ministro Luigi Di Maio quando diceva: «voteremo sì all'autorizzazione a procedere per Salvini, lo vuole anche lui». «Salvini ha detto "io mi voglio far processare", quindi il MoVimento 5 Stelle non gli farà un dispetto e voterà sì alla richiesta di autorizzazione a procedere. E al processo sarò il primo a dire che fu una decisione di Governo». A quanto pare di tanto coraggio non ci sarà alcun bisogno, rilassatevi. Dunque, il Ministro si salverà dal processo, come già anticipato dalla decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere. La salveranno i suoi alleati di Governo che a loro volta, per salvarsi la faccia, hanno esibito la commedia di una finta consultazione *on line* e ascolteremo dalla voce di volenterosi parlamentari, forse perché l'Aula è vuota, del tutto piegati a esclusive logiche di potere, le giustificazioni conseguenti. Esattamente quello che sulle memorie ha scritto il Presidente, avvocato Conte, e che abbiamo ascoltato da ministri come Toninelli, Bonafede e Di Maio, ovvero che una decisione presa in totale autoreferenzialità e abusando del suo ruolo, contravvenendo a precise norme nazionali e internazionali, assunta in nome e per conto di uno Stato che lei ritiene a immagine e somiglianza di un movimento politico che sul rancore e la paura del diverso ha fatto la sua fortuna elettorale, è stata presa collegialmente o meglio è collegiale in quanto risponde ad una linea politica indicata nel contratto e dunque lei non è perseguibile perché ha difeso il superiore interesse nazionale. Il collega Bonifazi ha già chiarito con precisione e puntualità nella Giunta le ragioni per cui il Partito Democratico ha votato per il sì all'autorizzazione a procedere: noi non abbiamo cambiato idea per due ragioni. Rifiutiamo di pensare che l'interesse nazionale potesse risiedere - allora, come ora - nel tenere segregate in mare per cinque giorni 177 persone, che avevano attraversato il deserto per mesi e mesi e sostato nelle carceri libiche, tra cui 29 minori non accompagnati, cinque uomini affetti da scabbia, altri malati di tubercolosi o polmonite e 11 donne stuprate - sì, stuprate - nei *lager* libici, mentre il Ministro degli esteri del Governo di accordo nazionale libico affermava la Libia non avrebbe accettato in alcun modo il rimpatrio di migranti illegali verso i Paesi del Nord Africa da cui erano venuti. Colleghi, l'interesse nazionale di quest'Assemblea e questa maggioranza di Governo coincideranno con il reato di umanità? Fatevi questa domanda, domani, quando voterete.

Il divieto di sbarcare non si è tradotto in atti ufficiali, ma in una pericolosissima sospensione del diritto nel rispetto di leggi nazionali e internazionali, mentre il Ministro ha tenuto in ostaggio 177 disgraziati, il diritto, le norme, le convenzioni internazionali, il codice della navigazione, il Governo e il Parlamento italiano, nonché la politica. Ha sospeso il diritto e l'umanità, riducendo quello che dovrebbe essere la politica per l'immigrazione di un Governo a un miserabile gioco di rapporti di forza, e questo sulla pelle di uomini, donne e bambini che potevano solo aspettare e pregare di riuscire a sopravvivere e non morire. *(Applausi dal Gruppo PD).* E vengo alla seconda considerazione: in un sistema costituzionale e democratico ci dev'essere o no un limite all'agire politico, a garanzia stessa della democrazia e dell'inviolabilità dei diritti fondamentali? L'essere stato votato dal popolo, come dice, la mette al di sopra della legge e le consente di giocare con la vita umana? *(Applausi dal Gruppo PD).* Per giustificarsi, lei ha automaticamente assimilato a terroristi la vita di persone profughe: un'altra bugia, ma quella vita non poteva e non doveva essere sequestrata e messa a rischio. Lei ha detto più volte che era finita la pacchia, riferendosi a persone per cui la pacchia non è mai cominciata; così dicendo, ha legittimato comportamenti aberranti, la cui gravità è sotto gli occhi di tutti ed è alimentata dalla sua bestia. È una responsabilità, la sua, inemendabile e imperdonabile. L'immigrazione - che non governeremo, finché non ne assumeremo per intero tutte le implicazioni e non saremo capaci di ridiscutere i rapporti di scambio - non è una questione di ordine pubblico pubblico che lei ha già messo seriamente in crisi chiudendo gli SPRAR); è una grande questione politica e, come tale, dobbiamo essere capaci di affrontarla, discuterla e governarla. *(Richiami del Presidente).* è evidente che non possiamo accoglierli tutti, lo è altrettanto come tutti debbano poter trovare accoglienza in Italia e in Europa, affrontando noi qui, con altrettanta serietà e responsabilità politica e umana, la scarsa efficacia, se non il fallimento, di una lettura delle cose che individua la soluzione cardine nella frontiera esterna e nei respingimenti. Lo voglio dire a quest'Aula semivuota: io, senatrice Bellanova, non mi sento meno colpevole se le persone muoiono a due metri da Lampedusa o nei *lager* libici. E di certo mi sento più colpevole pensando che stiamo pagando i carcerieri libici… *(Il microfono

Di fronte alla responsabilità lei si fa curato di campagna e dimostra il coraggio di don Abbondio. Ricordo, soprattutto a chi ha testi scritti, che si possono consegnare tranquillamente. Capisco chi deve fare un intervento orale, ma per chi ha i testi scritti il nostro Regolamento consente

vorrei rivolgere un ringraziamento, che non è formale, al Presidente della Giunta, nonché relatore, perché ho scoperto con immenso piacere che Maurizio Gasparri è una persona che ha il senso profondo delle istituzioni. Si può condividere o meno quello che dice o quello che pensa, però ha condotto i lavori con un grande equilibrio che credo gli vada riconosciuto. Tra l'altro, vorrei anche esprimergli la mia solidarietà, come abbiamo già fatto per il senatore Candiani, perché oggi ha ricevuto anche delle minacce e degli insulti via *web* e quindi credo sia doveroso. Non mi intratterrò a lungo, perché credo che il cuore ce l'abbia dato il tribunale quando ha presentato la richiesta per l'autorizzazione a procedere.

ha detto chiaramente a pagina 48 (andatevelo a vedere) che lasciava la valutazione delle ragioni politiche della condotta di Salvini alla Camera di appartenenza e, quindi, anche la valutazione della sussistenza di un preminente interesse pubblico.

il cui programma elettorale, votato democraticamente dal Paese a maggioranza, perché la maggioranza questo esprimeva, era chiarissimo riguardo al blocco degli sbarchi e al fatto che

È assurdo dire che un Ministro deve difendere le ragioni politiche nel processo: questo è pericoloso, perché le ragioni politiche le giudicano a maggioranza gli eletti democraticamente della Camera di appartenenza.

qui. Perché ha fatto bene Salvini, da un punto di vista politico, a fare quello che ha fatto? Perché non era la prima volta che il centrodestra si trovava di fronte alla questione relativa al blocco degli sbarchi.

Il ministro Pisanu, Ministro dell'interno di un Governo di centrodestra, nel 2006 venne indagato per abuso e omissione in atti d'ufficio, perché alcuni deputati di centrosinistra, in modo particolare di Rifondazione,

c'è una differenza fondamentale: quando accadde quell'episodio a Pisanu, il Governo reagì in modo corale e non vi fu bisogno di una verifica *on line* di quello che pensavano gli iscritti della piattaforma Rousseau.

che erano misure di contrasto all'immigrazione, per le quali era stato votato, anche allora, un Governo di centrodestra. Allora, per rispondere al tribunale dei Ministri,

che sono presso la Giunta, vi viene qualche sospetto a vedere degli esposti un po' pelosi. Se andate a vedere gli atti, troverete degli esposti di strane associazioni,

parte offesa nel processo contro Salvini. In più, sempre a novembre e dicembre, quindi in precedenza, considerando che la richiesta di autorizzazione a procedere era di gennaio, trovate pure una trentina di nomi, assistiti da uno studio legale, che chiedevano l'accesso agli atti, sempre perché volevano avere in mano degli elementi per poter aggredire il Ministro. Allora, mi dovete dire chi ha indirizzato una ONLUS di Napoli contro le discriminazioni per chiedere questi atti, chi ha indirizzato questi trenta degnissimi cittadini eritrei per organizzarsi e fare un'operazione di questo genere.

coerente con le sue opinioni. Anche se non ne condivido l'impostazione, sicuramente comprendo il suo voler svolgere una relazione di minoranza.

Presidente, era il 27 agosto quando il Ministro dell'interno, Matteo Salvini, sosteneva che era pronto a essere processato sul caso della nave Diciotti: «Se il tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire», diceva allora il Vice Presidente del Consiglio. Quando poi il tribunale dei Ministri ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere, Salvini ha in breve cambiato idea e nella lettera che ha inviato al «Corriere della Sera»

«in questo non c'entra la mia persona» (ci mancherebbe). «Innanzitutto il contrasto all'immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico», confondendo contenuti normativi e obiettivi politici, che sono due questioni profondamente diverse, tant'è che il ministro Salvini, nel giustificare il suo cambio di posizione spiega che «la vicenda giudiziaria è strettamente legata all'attività di Ministro dell'interno e alla ferma volontà di mantenere gli impegni della campagna elettorale», che però non possono essere distanti o divergenti da quello che le norme di legge dicono.

e che i giudici infatti lo accusano di aver violato la legge imponendo lo stop allo sbarco in virtù del suo ruolo di Ministro dell'interno. E il ministro Salvini, autoassolvendosi, afferma che si tratta di una decisione che non sarebbe mai stata possibile se non avesse rivestito il ruolo di responsabile del Viminale. Ma essere al Governo non significa essere al di sopra della legge. Lo Stato di diritto esiste per limitare la tirannia di chi governa: dove starebbe altrimenti la differenza fra lo Stato di diritto e lo Stato assoluto? ministro Salvini voleva farsi processare e raccontare ai giudici la sua verità; inizialmente, con dispiego di proclami video sui *social*, il Vice *Premier* era convinto di non dover chiedere che il Senato respingesse l'eventuale autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Così all'inizio diceva di voler fare Matteo Salvini e i suoi compagni di viaggio, del MoVimento 5 Stelle, gli sono andati dietro, ben contenti di sentirgli pronunciare queste parole. La senatrice Fattori: «Dobbiamo dire sì all'autorizzazione per essere coerenti con i nostri principi» (e forse sarà l'unica del MoVimento 5 Stelle che alla fine la voterà); il presidente della Commissione cultura della Camera Luigi Gallo:

«Ok a processo Salvini, lui stesso lo vuole»; il vice *premier* Di Maio: «Salvini ha detto "io mi voglio far processare" e quindi il MoVimento 5 Stelle non gli farà un dispetto e voterà sì alla richiesta di autorizzazione a procedere»; e infine il giramondo Di Battista: «Salvini rinunci all'immunità». tutte dichiarazioni del 27 e 28 gennaio scorso. Poi, fatto quanto normalmente non fa mai e cioè approfondire le carte, Salvini scopre che probabilmente se andasse davanti ai giudici qualcosa rischierebbe davvero e così cambia avviso e mette nero su bianco che pretende il pieno sostegno di tutta la maggioranza per non essere processato. Ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della legge costituzionale n. 1 del 1989, come è già stato più volte detto, il Senato nega l'autorizzazione «ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». La valutazione del Senato che noi siamo chiamati a fare è pertanto vincolata all'accertamento di due requisiti (ciascuno dei quali di per sé sufficiente a negare l'autorizzazione): la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e il perseguimento di un preminente interesse pubblico. La Giunta prima, e l'Aula oggi, sono chiamati a giudicare le azioni di un Ministro, che, come già detto, non può essere sopra la legge. E se oggi siamo chiamati a verificare la sussistenza di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un preminente interesse pubblico, l'interrogativo non può che trovare risposta nelle carte che il tribunale dei Ministri ha trasmesso al Senato e nella relazione che il tribunale dei Ministri di Catania ha inviato al Senato sul caso Diciotti si legge: «Nessuno dei soggetti ascoltati da questo tribunale ha riferito (come avvenuto invece per altri sbarchi) di informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di persone pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico nazionale». In quel passaggio il tribunale argomenta così la tesi che lo sbarco dei 177 migranti a bordo «non potesse costituire un problema cogente di ordine pubblico». Lo scrive il tribunale, nelle carte che ci ha inviato e che abbiamo letto. Dove è dunque l'interesse pubblico che lo stesso Salvini, nella sua lettera al «Corriere della Sera», richiama come elemento sufficiente per non concedere il via libera al processo, autoassolvendosi dopo aver per mesi sbandierato la tesi opposta? Diciamoci la verità: tutta l'azione del Ministro si muove per propaganda. La stessa propaganda che lo sta portando a nascondere gli sbarchi non solo ai cittadini e ai giornalisti, ma anche ai sindaci, che sono ormai quasi inconsapevoli degli sbarchi che avvengono sulle loro coste, che continuano ad avvenire sulle loro coste. Lui continua a fare l'uomo forte. Allora, Ministro che non c'è, continui a fare il forte anche di fronte alla legge. Si sottoponga al giudizio dei magistrati. Vediamo se è realmente più forte anche della legge, la stessa che dovrebbe tutelare le decisioni dei sindaci che quotidianamente si trovano a dover gestire il fenomeno degli sbarchi sulle proprie coste senza gli strumenti giusti. E questo solo perché, per l'interesse propagandistico di quello che vuole apparire come un uomo forte, si stanno sacrificando principi costituzionali sacri per il nostro ordinamento. Il ministro Salvini dimostri all'Aula la sua vera forza. Ne ha la possibilità: mostri al Paese intero il suo coraggio e la sua buona fede. È troppo facile fare il bullo con la divisa delle Forze dell'ordine e poi fuggire di fronte a quella stessa legge che tutti i giorni, combattendo e rischiando la vita, quelle donne e quegli uomini in divisa tentano di far rispettare. Un Ministro che scappa di fronte ai processi non è degno di indossare una divisa. Un Ministro che è convinto di poter autogiudicare il proprio operato, andando anche oltre il giudizio della magistratura, non è degno di servire questo Stato. Non è degno di sedere su questi banchi e infatti oggi non è qui ad ascoltare questo dibattito che lo riguarda. Il ministro Salvini ha oggi una grande opportunità. Dimostri la sua forza, così come tutti i giorni le migliaia di operatori, che sono costretti a districarsi nelle assurde norme che questa maggioranza ha scritto. Donne, uomini, volontari, sindaci, Presidenti Donne, uomini, volontari, sindaci, Presidenti di Regione, amministratori locali: per tutti loro non c'è alcuna immunità, ma dimostrano giorno dopo giorno, nonostante Salvini, nonostante questo Governo, di essere più forti di qualsiasi cosa. Ma, ahinoi, non mi aspetto e non ci aspettiamo nessun segnale positivo in questa direzione. C'è solo incoerenza, dimostrata dall'assenza fisica di questa sera. E l'incoerenza di fondo del ministro Salvini e del MoVimento 5 Stelle in questa vicenda è mossa esclusivamente dalla paura: la paura di essere processato e di essere condannato e, per effetto della legge Severino, Severino, decadere dalla carica e la paura di vedere dissolvere il Governo e la maggioranza e dover tornare a casa. Ma la paura non è mai buona consigliera. Napoleone Bonaparte sosteneva che ci sono due modi per far muovere gli uomini: l'interesse e la paura. In questa vicenda pare che sia Salvini, sia il MoVimento 5 Stelle si siano ispirati a questa massima. Ma Paolo Borsellino ci ha insegnato anche che la paura è umana e che la si combatte con il coraggio, quello che oggi manca sia al Ministro per farsi processare, sia al MoVimento 5 Stelle per essere coerenti con i loro principi.

grazie anche al Presidente della Giunta, che è presente, e ai relatori di minoranza. Io parlo, convinto che da qualche parte ci sia il Ministro; sono convinto che c'è anche in ragione della vicinanza, che è stata garantita durante i lavori della Giunta, la vicinanza dei colleghi che, ho capito, voteranno in un certo modo e in una certa direzione. Credo che questo accadrà perché c'è la presenza del Ministro, anche se noi non la vediamo. Di cosa tratta la convocazione odierna su questo punto? Lo hanno spiegato con pienezza di argomenti e di ragionamenti i miei colleghi che mi hanno preceduto. Il ministro Salvini è sottoposto ad accertamento giuspenalistico relativamente alla condotta tenuta nella sua qualità di Ministro dell'interno, riguardo alla trasformazione di una nave che ha una denominazione non casuale. Riflettiamo dedicata a Ubaldo Diciotti, non è una nave qualsiasi e non ha una denominazione qualsiasi. È la dedica a una personalità del servizio pubblico italiano, appunto il generale Diciotti, che si è distinto nel 1941 per operazioni di soccorso in mare; anche questo deve contribuire a far capire qual è il giudizio che tocca a quest'Assemblea quando ci occupiamo dell'argomento di cui ci stiamo occupando.

costosa non solo dal punto di vista della fatica che c'è, che si tocca con mano, nel rendere accettabile il giudizio che avete prefabbricato, ma anche dal punto di vista dei diritti che si stanno sospendendo sul piano della cultura dei diritti, della cultura delle regole e della legalità. Ho sentito fare ragionamenti impegnativi da parte di colleghi, i quali non credevano nel ragionamento che facevano, argomentando, ad esempio, su quella elevatissima categoria che è l'interesse pubblico prevalente: l'ordinamento si piega per rendere prevalente un interesse costituito. Su questo aspetto non c'è soltanto il diritto, che ci fa leggere, ma c'è anche la scienza della politica, la dottrina dello Stato, le dottrine politiche, tutto quello che ha scritto sulla paura che è il più grande studioso di paura dentro e contro le democrazie. Qual è stata l'operazione messa in campo qui? Un'operazione di comunicazione politica, che si nutre delle cartellette scritte del programma di Governo e che, però, per la pienezza della sua riuscita, aveva bisogno di una operazione - consentitemi, c'è un solo aggettivo - scandalistica, che determinasse una rottura,

Tra quali elementi? Quel programma di Governo, quella condotta e il sacrificio di interessi davvero rilevanti, quali sono quelli riferiti alla libertà delle persone. Non si può immaginare che si sospenda, anche solo per un giorno, la libertà delle persone di poter procedere, di spostarsi, per dare luogo alla realizzazione di quattro righe di un programma di Governo. La proporzionalità della condotta del Ministro dov'è?

(ce n'è uno che ha cultura della legge e delle istituzioni, che non vedo presente) e i molti avvocati stimati nelle loro libere professioni. Voglio fare l'esempio di un Ministro che ha leso

occupò un appezzamento di terreno di diverse proprietà private senza attivare le procedure. Lì ci fu la violazione di una regola, una norma, un bene custodito, qual è la proprietà privata, per evitare un rischio

se non della voglia di sopraffare e prevalere sul piano della comunicazione politica? Cari colleghi senatori, dobbiamo sapere che non cominciamo oggi la vita politica, giuridica e giurisprudenziale. La giurisprudenza non è giusfollia:

guardate che anche il dibattito tra Creonte e Antigone ci può aiutare: la legge dell'uomo stabilisce che tu non devi seppellire tuo padre,

soccorsi e aiutati. Ci sono i trattati internazionali, ma arrivano - starei per dire - appena dopo, perché i diritti delle persone sono preesistenti. In quest'Aula i Padri costituenti questo ci hanno insegnato: la preesistenza dei diritti fondamentali delle persone, anche davanti alla ragion di Stato. Noi abbiamo avuto molti toscani qui, anche in passato.

cari colleghi, perché c'è un costo che noi paghiamo: la lesione rimane. Che accade dopo? Perché si sta attenti a non rompere l'assetto istituzionale? Per ciò che può accadere dopo, per l'irrimediabilità.

tenere da conto il costo di quest'operazione, che vi serve, ma distrugge.

mi permetto di rilevare che, nonostante la discussione sia iniziata da quasi due ore e malgrado la richiesta accorata del nostro capogruppo, senatore Marcucci, il ministro Salvini ancora non si vede. Non credo abbia paura del dibattito. Le chiedo pertanto

se è vero che il Senato non è chiamato a decidere sull'innocenza o sulla colpevolezza del Ministro, è altrettanto vero che, per come è stato svolto il dibattito e tutte le le argomentazioni ultronee che sono state usate in quest'Aula, il tema si traduce sostanzialmente come segue: è giusto o meno che sia il giudice naturale a determinare l'innocenza o la colpevolezza, in questo caso, dell'inquisito? Questa scelta non è giuridica, ma è valoriale e culturale in una qualsiasi democrazia matura. La seconda premessa è invece una domanda: in uno Stato di diritto esistono azioni politiche sempre e comunque lecite, che sono legittimate dai voti presi o dai programmi elettorali, come abbiamo ascoltato poco fa, e che quindi possono essere sottratte al giudizio della magistratura? Ho iniziato il mio intervento con una premessa e una domanda per chiarire bene qual è il delicato contesto nel quale si muove questo dibattito, che non è quello relativo alla legge costituzionale del 1989: magari lo fosse, ma non è così. E proprio in ragione delle storture che sono state inserite in questo dibattito, in questi giorni e in questa sede, mi preme evidenziare quali sono i rischi che la Repubblica italiana e la democrazia corrono, nel caso in cui il Senato dovesse decidere di non procedere nei confronti del ministro Salvini.

luogo, la decisione investe due piani distinti: quello della libera determinazione dell'indirizzo politico dei Governi e quello dello Stato di diritto, democratico e costituzionale. I Costituenti avevano chiarito bene questo punto, in maniera inequivocabile: basta leggere l'articolo 96 della Costituzione, nella parte in cui espressamente prevede che i reati commessi nell'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere sottoposti alla giustizia ordinaria. Se questo è vero, come è vero, può chiunque affermare che l'azione politica è esente dal giudizio? Penso in maniera convinta di così come per tutti gli italiani, per i quali, nel caso dovessero commettere degli illeciti, c'è il giudice naturale. Perché per un Ministro non dovrebbe che il diniego allo sbarco è stato impartito fuori dal Consiglio dei ministri, che non è stato formalizzato e che è stato compiuto con un comunicato, se non ricordo male a margine di un vertice europeo. Subito dopo si sono precipitati il presidente Conte e altri Ministri, con lettere ed *e-mail*, in malo modo, tentando di di avallare una decisione che comunque non avevano mai preso. L'articolo 95 della Costituzione prevede per i singoli Ministri una responsabilità collegiale solo per gli atti decisi nel Consiglio dei ministri

maniera molto convinta. È bizzarra la giustificazione del ministro Salvini, che giustifica il suo diniego richiamando la norma che punisce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. È forse questo il caso? A me risulta che quelle 177 persone erano tutte controllate e tutte identificabili e sarebbero state - come poi sono state - inserite nel programma di accoglienza o addirittura portate in altri Paesi europei, quindi facendo venire meno il reato stesso al quale Salvini si appiglia. Pertanto, sebbene sia un obbligo costituzionalmente rilevante proteggere gli interessi dello Stato, quale evento catastrofico e imminente stava per accadere o sarebbe accaduto nel momento in cui quelle persone, tutte identificate, fossero sbarcate subito? Nessuno. Suggestiva è poi la tesi secondo la quale la politica, in questo caso dell'immigrazione, come è stato ripetuto anche poco fa in Aula, deve essere decisa dalla politica stessa, dal Parlamento, dai Ministri, dal Governo e non dai magistrati. Ritengo che sia troppo facile e banale dire che ciò è vero, ma detto in un contesto di questa natura, di carattere esclusivamente ed eminentemente giustificatorio, non è altro che la promulgazione perenne di un modello istituzionale, che ha eguali solo nelle dittature e in e in quei luoghi in cui l'immunità delle decisioni è sacrosanta e inviolabile. Noi siamo in un altro contesto, assolutamente diverso. Vado Vado avanti sempre riflettendo sulle dichiarazioni che ho avuto modo di leggere sui giornali. Persuasiva è la giustificazione secondo la quale l'interesse pubblico appare evidente alla luce degli atti successivamente esperiti in sede europea. È una giustificazione del Presidente della Giunta delle elezioni e delle la domanda è se il divieto allo sbarco, che con questa tesi si ammette (perché si dice che è servito per convincere l'Europa in una certa direzione), diventa lecito se altri Paesi, peraltro non assoggettati ad alcun obbligo internazionale in questa vicenda, non concordano con l'indirizzo politico del Governo. Non credo proprio e lo dico in maniera molto convinta. Una riflessione va fatta anche sul messaggio collegato a questo tipo di scelta, ovvero alla possibile decisione negativa sull'autorizzazione a procedere.

che per il potere, per mantenere le poltrone per capirci, i politici in carica sono pronti a superare ogni cosa, finanche le leggi che loro stessi votano e che a questo punto valgono per gli altri e non per loro.

produrrà danni; in particolare, in quella fascia dell'abbandono confermerà che i politici possono fare quello che vogliono. Questo è il messaggio peggiore che una classe dirigente potrebbe favorire. In caso di diniego all'autorizzazione il Senato si assumerà un'importante responsabilità nei confronti dello Stato di diritto, proprio perché in questo caso a differenza di quelli passati ci si interroga sui limiti dell'agire politico ed in particolare ci si chiede se il preminente interesse dello Stato costituzionale possa comportare la violazione degli obblighi fondamentali, quali quelli sul diritto di asilo e sulla libertà personale degli stranieri. signor Presidente, io credo che dopo questa decisione ci sia un prima e un dopo. Il dopo è il superamento non sanabile di un cardine democratico che aprirebbe le porte a percorsi inesplorati, con una buona dose di pericolosità sociale prima ancora che politica. Mi chiedo perché smantellare la nostra democrazia, la Repubblica italiana, insinuando criteri che nella democrazia non esistono.

ha rivolto al ministro Salvini sul caso Diciotti è veramente seria e grave; non è quindi possibile archiviarla né tenerla solo sul piano delle diverse o opposte opinioni politiche. Sequestrare donne, uomini, minori, limitare la libertà personale è una forma di violenza sulla persona che non può in nessuna occasione essere giustificata o considerata come effetto indesiderato delle scelte politiche di un Governo. Questo non è ammissibile. Desidero dire subito che non mi appartiene la posizione politica che identifica il ministro Salvini, o qualunque altro esponente del Governo della Repubblica italiana, come un nemico da abbattere e su cui fare cannibalismo becero, con linguaggi che alimentano odio o delegittimazione. Certo, considero le politiche di questo Governo e del ministro Salvini, *leader* della Lega, contrarie ai miei principi, a ciò che penso sia utile per l'Italia, per la sua crescita, per il suo benessere, per la convivenza civile e democratica. Ma proprio per questo non considero Salvini, lo ripeto, un nemico da abbattere, ma un avversario politico sì, da sconfiggere politicamente ma, innanzitutto, nel Paese. Io voglio sgombrare questa discussione dai toni del confronto partitico politico

da questa vicenda, perché lo riterrei un elemento qualificante della reputazione democratica del nostro Paese. È importante, però, che il Ministro accetti di essere giudicato come accadrebbe a qualsiasi altro italiano accusato di sequestro, come lui stesso aveva inizialmente affermato. Il comportamento corretto, cioè, è quello di chi si difende nel processo e non dal processo. Ma perché, ministro Salvini, lei ha cambiato idea? Lei e tutta la sua maggioranza di Governo avete preferito, con il voto di quest'Aula, il rifiuto, il diniego, di andare a processo e, quindi, di farsi giudicare nelle sedi proprie. Avete così tanta paura del merito dell'accusa che vi viene rivolta? Oppure, insieme a questo, volete un salvacondotto per proseguire, come stava avvenendo in queste ore con i quarantanove migranti a bordo della nave italiana Mare Jonio, in brutali attacchi alla dignità e libertà della persona? O, magari, ancora più in generale, per attaccare le libertà e le norme costituzionalmente garantite, che è, secondo me, il tema di merito su cui discutere?

Ministro abbia agito senza umanità, giocando con le vite delle persone, soffiando sulla paura dell'immigrazione e del diverso, come purtroppo fa troppo spesso. E per che cosa? Per qualche punto percentuale di consenso in più? Guardate che questo è davvero drammatico. Non saremo mai d'accordo con Salvini su questo. Mai la vita umana, in un sistema democratico, può essere sacrificata sull'altare di scelte politiche, quali che siano. E mai le scelte politiche di un Governo possono violare le leggi. il punto è proprio questo: distinguere politica e giustizia. Mi permetto di ricordarlo alla collega Modena, che invece ha detto che stiamo parlando di politica e che la politica non può essere affidata ai tribunali. Il punto, allora, è proprio questo: distinguere politica e giustizia, rispettando, però, gli spazi di ciascuna. Occorre distinguere il conflitto politico su una scelta, che, dal suo punto di vista, Salvini continua a difendere e che noi continuiamo a contrastare, dal giudizio penale su di essa. E solo un tribunale può decidere questo: se la decisione di non fare attraccare la Diciotti, una nave della Repubblica italiana, sia stata presa in violazione delle leggi e se, effettivamente, sia stato un sequestro. Non può giudicare il Senato su questo, non i *media*, non l'opinione pubblica, non una maggioranza parlamentare. Colleghe e colleghi, il voto cui siamo chiamati domani è questo: lasciare che le cose vadano secondo quanto è più giusto, facendo svolgere al tribunale dei Ministri il proprio lavoro, o piegare regole nazionali, costituzionali e internazionali e valori condivisi al puro interesse alla sopravvivenza di questo Governo e di questa maggioranza. Perché è di questo che si tratta, e lo sapete bene, cari colleghi della Lega, del MoVimento 5 Stelle, di Forza Italia e tutti coloro che pensano di votare no domani. Gli italiani ci guarderanno votare. Non alimentiamo l'idea di una politica che ha più diritti delle persone comuni. Non usiamo due pesi e due misure. Non facciamo passare il messaggio che basta essere un esponente del Governo per non essere sottoposti al giudizio della magistratura. Guardate che questo è un precedente gravissimo. Ministro Salvini, glielo chiedo nelle sue funzioni di giovane *leader* populista, di Ministro e di padre. Ma perché non dà un buon esempio? Si faccia processare. Rispetti il tribunale e accetti di essere giudicato come una persona sicura del suo operato, sicura di non aver infranto la legge. Semplicemente questo. Continuerò ad oppormi, con determinazione e costanza, alle sue scelte politiche, ad impegnarmi con tutte le mie forze per costruire un'alternativa al suo Governo nel Paese e poi nelle elezioni perché reputo il suo Governo dannoso per il Paese, ma guardi, Ministro, sarei la prima a congratularmi con lei se fosse assolto avendo scelto di farsi giudicare negli unici luoghi deputati al giudizio di merito, i tribunali, così come prevedono la nostra Costituzione, le nostre regole, le nostre leggi. Questa è la responsabilità che spetta a lei, ministro Salvini, a tutto il Governo e alle senatrici e ai senatori che siedono in quest'Aula. *(Applausi

Il punto è se quest'Assemblea, se il Senato della Repubblica ha deciso di spogliarsi di una prerogativa che la Costituzione gli consegna oppure no.

non è venuto a dire che domani sarà presente per difendere un interesse pubblico che abbiamo tutelato fino alla fine. No. È venuto a dire che domani sarà qui a metterci la faccia perché quella è la linea politica del Governo.

- ha portato in prossimità dell'illecito ed è da chiarire se l'operato di questo Governo sia in prossimità dell'illecito o sia dentro alle prerogative della legge e della Costituzione e non lo può chiarire quest'Assemblea. Quest'Assemblea deve solo decidere

non c'è più nessun reato perseguibile. Il senatore Pillon ci ha spiegato che poiché Salvini è a favore dei respingimenti e della riduzione degli sbarchi, ha fatto bene a non far scendere

utilizzare lo strumento della tortura per raccogliere quella informazione perché è in ballo l'interesse nazionale. Ma ci rendiamo conto, Presidente, di che cosa sta consentendo quest'Assemblea? Io penso che non sia affatto vero che la relazione del presidente Grasso

Cito: «In altri termini, affinché il Senato possa legittimamente rigettare la richiesta di autorizzazione a procedere, si deve ritenere che l'interesse pubblico che il Ministro intende difendere sussista effettivamente in concreto e sia preminente rispetto al bene protetto dalla norma» e nessuno in quest'Aula ha saputo descrivere dove sta l'interesse pubblico. Si è detto solo che noi siamo contrari ai clandestini oppure che si sta attuando il contratto di Governo. Nessuno dei due punti appartiene all'interesse pubblico. E se qualcuno in quest'Aula ha un dubbio

di questo stiamo parlando, non delle felpe né delle giacche né dei migranti, ma del fatto che un Governo possa venire prima della libertà costituzionalmente sancita di ogni individuo; questo è il punto.

C'è il rischio infatti che «poiché la valutazione cui è chiamato il Parlamento è una valutazione "politica", essa possa diventare una scusa per fare rientrare in tale concetto tutto ciò che si vuole». Ma è evidente che se ciò è ad attuazione del programma di Governo, cioè di maggioranza, di fatto stiamo scudando l'Esecutivo di un Paese,

non mi rivolgo al MoVimento 5 Stelle e agli amici e colleghi della Lega, in relazione alle loro dichiarazioni e a ciò che hanno sempre detto di intendere, di volere e di pensare: no, quello lo fanno i giornali e la polemica politica.

Ecco, non credo che la questione sia questa, ma che sia giusto che gli organismi di questo Senato e della Costituzione e la Repubblica vedano le garanzie e le prerogative costituzionali garantite a tutti, compresi i parlamentari e i senatori. però c'è una domanda evidente, alla quale non vogliamo rispondere, e cioè il fatto che quest'ipotesi di reato, commesso da un Ministro, lede in maniera evidente un principio costituzionale: l'autorità giudiziaria deve andare a verificare se tale reato è stato commesso o meno, perché oggi è solo un'ipotesi.

alla valutazione espressa da cittadini che, tramite una piattaforma gestita da chissà chi, hanno detto che questa autorizzazione non ci doveva essere. c'è stata una valutazione di documenti - ripeto che la sua relazione mi trova in profondo disaccordo, ma è frutto sicuramente di un lavoro serio che voglio riconoscerle

non è stata messa nella condizione di fare il proprio lavoro seriamente o, meglio, questi membri hanno deciso di non farlo; hanno deciso di offendere le istituzioni. Hanno preferito rinunciare a un ruolo che gli veniva dato dai cittadini e, quindi, hanno offeso anche il Senato; hanno invalidato un lavoro serio, ma noi proviamo a continuare a essere persone serie e vogliamo provare a spiegare invece il perché delle nostre motivazioni. La Giunta prima e l'Assemblea poi sono chiamate a verificare se sussista una delle due ragioni *extra ordinem*, che qui sono state descritte bene, previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ossia - è stato ripetuto più volte ed è giusto ripeterlo - se l'interessato «abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

ma se l'ipotetico e allo stato non ancora dimostrato reato sia giustificabile alla luce di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero di un preminente interesse pubblico. Non siamo giudici qui e nessuno di noi vuole emettere sentenze

Lei ha affermato che la Giunta non è chiamata a disquisire sulla natura politica o amministrativa di un atto, salvo poi però arrivare a conclusioni che non possiamo accettare. Il primo punto debole che vogliamo evidenziare è il fatto che la relazione si fissa nell'affermazione dell'esistenza del perseguimento di un interesse pubblico governativo. La legge di riferimento, però, come abbiamo provato a ricordare e come provo a ripetere come un mantra, utilizza altre parole e altri aggettivi, proprio perché la rinuncia alla verifica giurisdizionale può essere attuata solo in nome di interessi tali da compensare questo agire *extra ordinem*. Non basta. Nella relazione del presidente Gasparri, dopo aver escluso la sussistenza di un interesse personale (per esempio, qualora ci fosse la ricezione di denaro per un atto d'ufficio), si estende questa esclusione anche all'interesse partitico, come se la Lega non avesse interesse partitico nella lotta contro l'immigrazione. È il suo cardine: non vuole risolvere il problema perché senza quel problema non ha consenso perché ha costruito tutto il suo consenso sul caos creato proprio dal problema dell'immigrazione. È su questa esclusione che la relazione incorre in quello che io ritengo una sorta di inciampo logico: nell'intento di coprire e superare la falla di questo impianto, restituisce però la vera finalità della condotta del Ministro. Cosa dobbiamo seguire in questa richiesta? Una semplice domanda: il contrasto all'immigrazione è un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero un preminente interesse pubblico? La risposta è confusa anche da parte della maggioranza. Lo ha detto la piattaforma Rousseau che, posta di fronte a questa domanda, non ha dato percentuali bulgare, ma alquanto mescolate tra di loro. E sappiamo benissimo

La condotta posta in essere dal ministro Salvini è stata funzionale a tutelare quel presunto interesse pubblico? Solo ed esclusivamente con quella condotta era possibile tutelare quel preminente preminente interesse pubblico non potendosi adottare nessun altro comportamento? Va da sé che la conclusione è palese e sotto gli occhi di tutti, perché con questa condotta non si è contrastata l'immigrazione, e lo si è visto anche oggi. visto anche oggi. Esistono ancora navi che sbarcano; esistono ancora navi in mezzo al mare, quindi quella condotta non ha contrastato il fenomeno. Sono paradossi, lo so, ma questi paradossi servono a dimostrare come le conclusioni presentate dal presidente Gasparri non siano congruamente motivate, perché non portano a compimento il tentativo di quella sorta di *maquillage* di quell'evidente interesse del partito di Salvini che è il preminente interesse pubblico. Questa similitudine non c'è, le due cose non coincidono. Questo, sia chiaro, non significa che il Ministro sia responsabile di sequestro di persona. Questo - e lo ribadisco - non significa che il Ministro sia responsabile del reato di sequestro di persona. Nessuno di noi è tenuto qui a dirlo, ad accusare e a saperlo. Intendo però ribadire che l'assenza di questa evidenza nei termini indicati dalla legge di riferimento non può in alcun modo consentire l'attivazione di una garanzia che non è ragionevole.

perché è proprio l'articolo 9 a concedere un potere a questa Assemblea nel negare l'autorizzazione a procedere al ministro Salvini, per quello che è stato un reato ministeriale. Ma l'articolo 9, nel definire le esimenti, le scusanti, come è già stato rappresentato, che creano indubbiamente quegli spazi di discrezionalità politica che altri colleghi hanno richiamato, incontra dei limiti nei principi della cultura giuridica nazionale, posta sia dall'ordinamento interno che dalle norme delle convenzioni internazionali. Sono proprio questi principi che delimitano il confine del giudizio a cui quest'Aula dovrà attenersi. Il giudizio e questi principi sono posti a tutela di un sistema valoriale in grado di creare fortunatamente una gerarchia di tutele e di garanzie delle libertà fondamentali delle persone. Spetta a noi oggi e domani, dunque, il nostro giudizio domani sarà non più appellabile da altri poteri e da altri soggetti. Quindi abbiamo una grande responsabilità. Nel caso di specie, l'interesse pubblico indicato dal ministro Salvini a giustificazione della sua condotta

allo specifico della privazione della libertà personale di 177 persone trattenute illegittimamente per sei giorni a bordo di una nave della Marina militare italiana nel porto di Catania. Il Ministro doveva cioè dimostrare che quell'interesse preminente non poteva essere perseguito in altro modo; e si doveva dimostrare che la condotta stessa non avesse ecceduto quanto strettamente necessario per realizzare quello stesso interesse pubblico. non mi appare nemmeno condivisibile la tesi espressa dal presidente Gasparri nella sua proposta, secondo la quale in teoria non potrebbe mai configurarsi un reato ministeriale in relazione a fattispecie criminose che ledano in modo irreversibile diritti fondamentali. Paradossalmente non è la reversibilità del reato, infatti, a qualificarlo come ministeriale, perché in teoria si potrebbe arrivare anche al compimento di un reato grave, quindi a ledere in modo irreversibile dei diritti, qualora vi fosse una concreta e attuale minaccia di un interesse supremo dello Stato quale la sicurezza pubblica o la salute, per esempio, di una comunità. comunità. Vi doveva essere quindi una situazione di reale pericolo dell'integrità dello Stato, una minaccia concreta dei diritti costituzionali dei cittadini che il Ministro non ha saputo argomentare. In tale quadro quello che ci pare indiscutibile, al contrario, è che non può essere adottata in alcun modo la finalità di un obiettivo politico di governo e di attuazione di impegni del contratto di maggioranza, quali le politiche migratorie ridotte a mero strumento di propaganda, come scriminante generale in sede penale, in quanto tale tesi - è stato sottolineato anche dai miei colleghi porterebbe la ragion di governo ad autorizzare sempre violazioni di diritti garantiti dall'ordinamento nazionale e internazionale. La ragion di governo costituirebbe in tal solco una vera minaccia allo stato di diritto e alla nostra democrazia. Presidente, nella memoria depositata dal Ministro dell'interno, non emerge alcun pericolo o minaccia tale da giustificare la compressione di diritti fondamentali, tantomeno una minaccia paventata alla sicurezza pubblica, considerato che nessun protocollo di protezione della sicurezza o ordine pubblico è stato mai attivato. Senza dubbio, pertanto, la limitazione della libertà personale con un atto amministrativo compiuta dal Ministro rappresenta una scelta gravissima che si colloca su una linea di frattura rispetto al principio generale posto dall'articolo 13 della Costituzione, per il quale la libertà personale è inviolabile, quindi anche la libertà personale di migranti e richiedenti asilo, e può essere limitata solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Riteniamo pertanto che la limitazione della libertà di 177 persone rappresenta un precedente del tutto inaccettabile per i principi del nostro ordinamento giuridico democratico fondato sul diritto. Riteniamo che l'autorizzazione debba essere concessa e che il Ministro abbia il diritto di difendersi nel processo, ma non dal processo, anche se il Ministro non sembra averne il coraggio. Presidente, oggi noi abbiamo una grande responsabilità che può costituire un precedente. Non concedere l'autorizzazione in nome della ragion di governo significa trasformare l'immunità ministeriale da strumento di tutela di funzioni proprie istituzionali a un privilegio. Voi della cittadinanza, dove uno vale uno, state solcando una pericolosa frattura, un'ulteriore distanza tra chi governa e il popolo governato. Voi oggi, per un mero scambio tra controparti di governo, voi che dicevate di demolire la casta, ne state rafforzando la difesa e l'inviolabilità: siatene consapevoli. finestra") *(PD)*. Signor Presidente, ci troviamo oggi a trattare un tema che è un fatto unico per la storia repubblicana: il tribunale dei Ministri ha chiesto l'autorizzazione a procedere per il ministro Salvini in virtù di una valutazione che riguarda l'aspetto che contraddistingue la sua attività di Ministro, quindi relativamente all'abuso dei poteri soprattutto nella funzione di pubblico ufficiale. Oggetto dell'abuso sono le 177 persone private della libertà. Il tema di fondo però è di ordine giuridico, come è stato trattato in maniera esaustiva in tutti gli interventi e direi

che riguarda l'attività di un pubblico ufficiale, di un Ministro in questo caso. Noi dobbiamo pensare che anche le garanzie funzionali ai servizi di sicurezza incontrano dei limiti, il limite assoluto del divieto di reati contro la persona nello specifico e quindi, se anche in quel caso ci sono dei limiti, noi dobbiamo ragionare sul fatto che perfino le attività di un Governo e di un Ministro nella gestione dei flussi migratori

Va fatta infatti una comparazione, come è stato ben spiegato in molti interventi, tra il fine pubblico perseguito e il sacrificio dei mezzi. Il Ministro, nello specifico, si sottrae alla giurisdizione solo se il comportamento dello stesso sia volto a tutelare un bene giuridico costituzionalmente preminente rispetto a quello compresso. La valutazione di questi due pesi, questa comparazione è del tutto assente nelle valutazioni che anche il Presidente della Giunta ha fatto nella sua relazione di maggioranza. Nessun atto politico può ledere la sfera giuridica soggettiva dell'individuo, l'inviolabile diritto alla libertà personale. L'articolo 13 della Costituzione spiega chiaramente che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Non può essere condivisibile il fatto che un Ministro possa avanzare il supposto perseguimento di un preminente interesse pubblico per sottrarsi al principio di responsabilità e al principio di legalità, che sono principi cardini dello Stato di diritto e non vi sono soggetti che possono derogare ai limiti posti dall'ordinamento costituzionale. Tra l'altro, in questa vicenda è paradossale, come veniva detto prima anche da alcuni miei colleghi, che il preminente interesse pubblico, che è un valore concettualmente rilevante ed importante, venga di fatto a coincidere con l'interesse della coalizione di maggioranza, con l'interesse rappresentato dal contratto di Governo ed è incredibile che non si faccia una valutazione accurata su questo aspetto. Infatti interpretare così il concetto di preminente interesse pubblico, e cioè pensare che l'azione di Governo, proprio perché persegue un interesse pubblico preminente, possa derogare ad alcuni principi e ad alcune norme di legge, ci porta ad una visione dello Stato che credo sia da contrastare; allo Stato assoluto, allo Stato come fine, allo Stato sovrano, allo Stato che è sottratto alla legge: questa è la visione che in qualche modo viene portata

In quei giorni si sono concretizzati una serie di errori e di omissioni notevoli e si è perso il senso dello Stato di diritto: 177 persone private dei diritti civili e politici sanciti dalle convenzioni internazionali sull'asilo, sulla vita delle persone. In quei giorni si è giocata una contrattazione politica molto cinica tra Governo italiano e Unione europea, senza spazio per le mediazioni diplomatiche che avrebbero potuto produrre molto di più e molto meglio e, soprattutto, si è voluta in quel modo esercitare una pressione sull'Unione europea sul tema delle politiche dell'immigrazione, quando invece sappiamo bene che l'unica soluzione per la gestione condivisa dei flussi migratori è la riforma del Regolamento di Dublino e non delle attività scenografiche utili solo per la propaganda e per il soddisfacimento dei *follower* e di coloro che poi sui *social* sono pronti a mettere un «mi piace» che non costa nulla. Appare evidente, quindi, che queste riflessioni sono rimaste sicuramente a margine delle decisioni della maggioranza; è prevalsa una subalterna fedeltà a uno scellerato contratto di Governo piuttosto che ai principi costituzionali che preordinano anche il nostro ruolo di rappresentanti delle istituzioni. Ammettetelo senza reticenze: procedere alla negazione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini non è altro che uno scambio sul piano della sopravvivenza del Governo. Nei miei appunti avevo scritto che vi era uno scambio tra il no al processo a Salvini e il "ni" alla TAV, perché di quello si è trattato. Andate avanti così, per accordi momentanei su questioni che riguardano l'attività di Governo e lo fate a danno dell'Italia. Un Paese dovrebbe essere governato con decisioni chiare e non con uno scambio continuo, che avviene tra voi che esercitate alternativamente la funzione di minoranza e maggioranza: un giorno viene sostenuto un provvedimento che è più favorevole alla Lega, e e magari c'è il finto contrasto del MoVimento 5 Stelle, la volta dopo il MoVimento 5 Stelle ha un provvedimento da sbandierare e la Lega fa una finta opposizione interna. Facendo così svilite il ruolo delle istituzioni, anteponendo l'accordo di Governo al rispetto dei principi di legalità

ma ci vuole rispetto per il Parlamento e credo sia giusto fornire il vostro punto di vista. Come potete guardare alla vostra storia senza avere un po' di imbarazzo? Nel 2014 Di Maio diceva che in Italia l'immunità è sempre stata uno scudo per la politica e mai una garanzia. parlava di Parlamento pulito come punto d'arrivo di ogni impegno politico nel nostro Paese. Con un voto voi butterete a mare tutto il vostro incessante richiamo alla onestà e alla legalità. Faccio appello alle coscienze dei parlamentari affinché si superi l'appartenenza acritica a un accordo di Governo, in ragione della suprema funzione istituzionale che ci deve spingere al rispetto delle leggi e alla tutela delle libertà individuali da queste previste. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli senatori, ciò che è accaduto lo scorso agosto e ciò che stava accadendo in queste ore apre una ferita profonda nel cuore dei sacri e altissimi valori posti a fondamento del nostro Paese e della nostra comunità. Ancor prima della violazione delle leggi e delle convenzioni internazionali suscita sgomento la grave profanazione di quei principi universali che affermano, al di sopra di ogni ragione di Stato, la difesa dei fondamentali diritti di tutti gli esseri umani.

Un tradimento del principio di eguaglianza e di pari dignità di tutti gli uomini, del rispetto e dell'amore per il prossimo, della pratica della solidarietà: valori cui la nostra Costituzione si ispira e che devono sempre illuminare l'agire delle istituzioni del nostro Paese. Il caso della nave Diciotti rimarca un grande dilemma etico e morale che attiene alla coscienza di ognuno: impedire lo sbarco di 177 esseri umani, tra cui 29 bambine e bambini, e lasciarli in mare per giorni e giorni per usarli come leva nelle negoziazioni con gli altri Paesi europei è un atto che travalica ogni ragionamento giuridico, politico e di pura umanità,

Quelle drammatiche giornate sono state l'emblema di un uso rovesciato della forza, esercitata solo nei confronti dei più deboli e mai nelle sedi opportune; di chi realizza il proprio potere per violare senza alcuna giustificazione le leggi dello Stato e le libertà fondamentali che la nostra Costituzione riconosce a tutti indistintamente; di chi si rifugia dietro il pretesto dell'ordine pubblico per alimentare la macchina della propaganda. Signor Presidente, ho l'onore e l'onere di sedere nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani umani e, alla luce di queste vicende, mi chiedo: quale credibilità istituzionale può avere questa Commissione se un membro del Governo tratta i diritti umani come merce di scambio? Qual è il valore del ruolo mio e delle onorevoli senatrici e senatori, che dedicano parte della loro esperienza e delle loro energie a questioni così delicate e urgenti e urgenti per entrare nel merito delle stesse al fine di costruire e rimarcare la linea della responsabilità comune traducendole in scelte politiche conseguenti, se poi l'Esecutivo, con i suoi atti, si dimostra difforme e arbitrario nelle decisioni, svuotando in questo modo il principio della reciprocità politica e dilatando i confini dell'azione di Governo ben oltre le coordinate istituzionali? La vicenda Diciotti sarà a lungo ricordata come uno dei momenti più bui della storia del nostro Paese, un episodio che ci auguriamo resti isolato. In quest'Assemblea potrebbe andare in scena il secondo atto di questo dramma. voi tutti - perché a noi è già chiaro - il compito di decidere se a un membro del Governo può o no essere concesso di agire elevandosi al di sopra della legge, smarcandosi dal dovere di realizzare, nel concreto di ogni specifica circostanza, il peso fecondo dei principi morali. Si tratterebbe di un pericoloso precedente di compressione dei diritti, che potrebbe essere invocato in situazioni diverse, ma analoghe. una grave ferita allo Stato di diritto della nostra democrazia affermare in maniera esplicita la facoltà, in capo a un Ministro, di derogare alle leggi nazionali e internazionali cui tutti siamo sottoposti, perché ciò vorrebbe dire arrendersi al fatto che, ancora oggi, le più elementari tutele riconosciute agli esseri umani in quanto tali e in quanto persone possono essere calpestate, travolgendo la libertà e la dignità E qualcuno deve ancora spiegarci come 177 esseri umani possano rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica se è vero che abbiamo fatto nostra - e non deve restare solo una dichiarazione di intenti quella linea d'orizzonte che vede nell'altro e nel bene della persona la destinazione del nostro impegno: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito». Deve spiegarci come mai questo trattamento sia stato riservato alle persone a bordo della nave Diciotti, mentre nell'agosto del 2018 sbarcavano altre persone nell'assoluto silenzio mediatico e in totale sicurezza. E a cosa è dovuto il cambiamento di postura politica rispetto alla prospettiva del giudizio, probabilmente frutto di forzature politiche successive, ammantate da una presunta ragion di Stato, ma - piuttosto - aventi al fondo la ragione di Governo e la salvaguardia di equilibri politici? Un Ministro della Repubblica non può perseguire interessi di parte, travalicando precisi limiti di ordine costituzionale e sovranazionale, sconfinando nella gestione arbitraria e nella sovversione dei valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. È uno scenario intollerabile per una democrazia liberale e per uno Stato civile come il nostro. Anche in questa sede, nel luogo autorevolissimo del confronto, delle decisioni e delle scelte, non dobbiamo dire le parole che vincono, ma le parole che salvano. Qui devono definirsi con chiarezza condotte politiche che abbiano dentro la forza e la bellezza faticosa e tenace di questa responsabilità: una responsabilità da viversi in nome dell'umanità tutta.

che non ha precedenti nella storia del Parlamento italiano e che assumerà una valenza generale dal punto di vista giuridico e istituzionale, prima ancora che politico. Presidente, l'autorizzazione a procedere di cui si chiede la concessione è in ordine ad un reato estremamente grave, come hanno ricordato tanti colleghi: sequestro di persona aggravato, previsto e punito dall'articolo 605 del codice penale. tribunale di Catania, chiede al Parlamento, a questa Assemblea, l'autorizzazione a processare il Ministro dell'interno, che è stato accusato di avere privato della libertà personale, per sei giorni, 177 persone, tra cui alcuni minori, in deliberata violazione di norme nazionali e convenzioni internazionali, abusando dei suoi poteri e con l'aggravante di essere un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. È un fatto senza precedenti. Nello Stato democratico e di diritto tutti sono soggetti alla legge e nessuno può derogare i limiti posti dall'ordinamento costituzionale: è un principio fondante delle democrazie, compresa la nostra. Secondo il principio di responsabilità, il soggetto che ricopre un ruolo politico risponde delle funzioni pubbliche che esercita sia in sede politica, che in sede giudiziaria e questo principio di responsabilità è connesso e deriva dai principi di uguaglianza e di legalità. L'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n.1 del 1989, più volte richiamata in quest'Aula, prevede che la Camera competente possa negare l'autorizzazione a procedere richiesta per un reato ministeriale, ma solo a precise condizioni e in particolare se reputa se reputa che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Sono chiare la *ratio* e la finalità di questa norma: la salvaguardia dell'operato del Ministro da interventi della magistratura penale quando l'operato del Ministro sia stato determinato da esigenze eccezionali. Secondo la giurisprudenza costituzionale, secondo le pronunce della Corte costituzionale che più volte è intervenuta sul tema, questa deroga eccezionale è soggetta ad una stretta interpretazione ed è limitata dal diritto positivo, dai principi di cultura giuridica alla base del nostro ordinamento. In assenza di quei requisiti, la deroga eccezionale prevista dall'ordinamento diventa un privilegio incompatibile con i principi del nostro ordinamento costituzionale Gruppo PD)*, a partire dal principio di pari trattamento nell'esercizio della giurisdizione di tutti i cittadini, Ministri compresi. intendono negare l'autorizzazione a procedere con argomentazioni vaghe e inconsistenti, senza le congrue motivazioni che devono essere alla base di questa negazione. Non abbiamo infatti ravvisato motivazioni solide nella relazione di maggioranza che abbiamo ascoltato questa sera. Assumere questo tipo di scelta e negare l'autorizzazione a procedere in assenza di motivazioni circostanziate equivale a sottrarre il ministro Salvini ai principi di responsabilità e di uguaglianza, che sono due principi cardine dello Stato di diritto. Signor Presidente, oggi non stiamo votando solo su una specifica vicenda giudiziaria, pur molto rilevante.

lo Stato è il fine e il sovrano è *legibus solutus,* è al di sopra della legge; invece, negli Stati costituzionali di diritto come il nostro, lo Stato non è un valore in sé, ma uno strumento finalizzato alla tutela della persona umana e dei diritti fondamentali delle persone; la ragion di Stato, che pure è ammessa, non può prescindere dal rispetto dei principi dello Stato costituzionale di diritto. Questa è la posta in gioco. Inoltre, il sottrarsi alla giurisdizione ordinaria è compatibile con i principi dello Stato di diritto solo se il comportamento che integra la fattispecie di reato sia volta a tutelare un bene giuridico preminente rispetto a quello compresso, ma questa valutazione deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza, razionalità e proporzionalità e per un tempo strettamente limitato: la deroga è ammessa, ma a precise condizioni e secondo precisi criteri. Sostenere, come abbiamo ascoltato in quest'Aula, che ogni interesse di natura pubblica, ogni atto politico sia di per sé preminente, equivale ad ammettere l'uso di qualsiasi mezzo per conseguire qualunque finalità governativa, senza proporzionalità e senza controllo: non è più Stato costituzionale di diritto, ma Stato assoluto; si legittima un potere assoluto e si contraddice l'essenza stessa del nostro Stato di diritto così come è scritto nella Costituzione. È questo il punto politico più rilevante della discussione odierna e della decisione che dobbiamo assumere, perché il Senato e quest'Assemblea sono chiamati a riaffermare che l'Italia è uno Stato di diritto in cui sono in vigore i principi di responsabilità e uguaglianza. Questo è il punto, signor Presidente. La maggioranza, negando l'autorizzazione a procedere, di fatto fa coincidere il preminente interesse pubblico con una ragione di Stato assoluta e fine a sé stessa. Questo è il punto, perché nella relazione di maggioranza non c'è comparazione tra i beni pubblici essenziali per individuare l'interesse pubblico preminente cui sacrificare il diritto della persona: si sacrifica un diritto di libertà senza un reale interesse pubblico preminente. Signor Presidente, avviandomi a concludere, per noi l'obbligo di salvare le vite umane in mare è un dovere che prevale che prevale e l'Italia ha aderito a convenzioni internazionali che regolano la materia. Il legislatore statale non può derogare a queste convenzioni internazionali, tantomeno un Ministro nell'esercizio delle sue funzioni può prescindere la pretesa del ministro Salvini di aver agito per difendere i confini italiani, come abbiamo letto, non ha alcun fondamento, perché questi 177 naufraghi che sono stati tenuti in ostaggio per sei giorni erano a bordo di una nave militare italiana, erano già dentro i confini della Patria, dentro i confini nazionali e non c'era alcun confine da difendere in questa fattispecie. Il principio costituzionale preminente nella vicenda della nave Diciotti è l'*habeas corpus,* la tutela della libertà personale sancita dalla nostra Costituzione, e la libertà personale di quelle 177 persone è stata compressa senza alcuna ragionevolezza, senza alcuna razionalità e senza alcuna proporzionalità. È sulla base di questi fatti che noi riteniamo che nell'azione del ministro Salvini non si possa ravvisare, né la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, né il perseguimento di un preminente interesse pubblico.

l'immunità funzionale garantita dalla legge costituzionale. Sono questi i motivi per cui noi voteremo per concedere l'autorizzazione a procedere, consentendo al ministro Salvini di fare quello di cui, almeno a parole, non ha paura: difendersi nel processo, davanti ai giudici legittimati dalla legge italiana.

Signor Presidente, penso che ci troviamo di fronte ad una vicenda grave, per ragioni sia specifiche che generali. Per ragioni specifiche, perché questa vicenda nasce dalla decisione - a nostro avviso sciagurata - di giocare con i diritti umani di 177 persone indifese. Per ragioni generali, perché, agendo nel modo in cui ha agito il ministro dell'interno Salvini e in cui ha agito il Governo, si è arrecata una grande ferita ad alcuni principi ai quali non si dovrebbe mai derogare in una democrazia ben ordinata, ben funzionante e degna del proprio nome. Si è arrecata una ferita allo Stato di diritto, e questo non lo si dice mai abbastanza. Noi sentiamo la necessità, come Gruppo Partito Democratico, anche dando vita a una lunga serie di interventi come abbiamo fatto questa sera,

Dicevo che per noi diventa essenziale riaffermare il principio che il perseguimento di un impegno elettorale non autorizza nessuno, qualsiasi sia la carica che egli ricopre, a porsi al di sopra della legge. Intendiamo riaffermare il principio che chi vince le elezioni non acquista il diritto di violare le norme penali; chi vince le elezioni non acquista il diritto di dettarsi da solo le regole e non acquista il diritto di strafare. *(Applausi dal Gruppo dover ripetere nell'Aula del Senato queste cose, ma vediamo che c'è, da parte delle forze della maggioranza e da parte del Governo, un modo di procedere che sembra dimentico, ignaro, di una delle massime fondative della civiltà democratica occidentale. Diceva Immanuel Kant che il diritto non deve mai adeguarsi alla politica e che è la politica che, in ogni tempo, deve adeguarsi al diritto. Questo principio è finito nel dimenticatoio per una parte rilevante di quest'Assemblea, e non soltanto per la maggioranza e questo sentiamo la necessità di sottolinearlo con forza. Vediamo che non ci sono gli elementi per dire che sono rispettate la lettera e la sostanza della legge costituzionale n. 1 del 1989, che disciplina la figura giuridica del reato ministeriale. Dov'è l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, che la condotta del ministro Salvini e del Governo avrebbero protetto? Dov'è l'interesse pubblico preminente? Non si vede. E non si vede, non perché è nascosto, ma perché non c'è. PD)*. Credo che noi dobbiamo seriamente interrogarci su quello che è avvenuto e anche sul modo con cui si è cercato di giustificare l'operato del Ministro e del Governo. La legge n. 1 del 1989 prevede che si possa derogare a una norma dello Stato se, appunto, si persegue un interesse pubblico preminente o un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ma prevede che si dimostri l'esistenza di interessi del genere, non che si proceda per autocertificazione. La cosa grave, e anche un po' ridicola, della discussione alla quale pezzi di maggioranza hanno dato vita è questa: si è affermato che questo tipo di interessi si possono autocertificare. Ma non esiste l'autocertificazione in questo ambito. Non c'è nessun motivo che porti a pensare che la volontà del ministro Salvini di attivare una rincorsa al consenso, tenendo in vita nel Paese una strategia della tensione che si basa sulla volontà

Anche l'assenza del Ministro stasera non è cosa alla quale noi ci rassegniamo con facilità. È un atto, politicamente parlando, sia di pavidità che di furbizia ma non di pavidità e non di furbizia abbiamo bisogno in queste Aule: avremmo bisogno di verità, di coraggio, di dibattito franco. Il Ministro, rendendosi irreperibile ai fini del nostro dibattito, viene meno anche a questo dovere e viola questo dovere, come ne ha violati molti altri. Mi sento poi in dovere di mettere in evidenza che l'episodio di cui stasera stiamo discutendo si aggiunge ad altri episodi tutti insieme, questi fatti configurano una visione della democrazia parlamentare presso le forze di maggioranza che ci allarma sempre di più. Io vedo infatti un filo rosso collegare i fatti di cui stasera dibattiamo con gli attacchi alla magistratura, con gli attacchi alle autorità indipendenti, con gli attacchi agli organi di garanzia, con il dileggio del Parlamento, con la patente violazione delle prerogative del Parlamento che abbiamo visto fare in occasione dell'ultima legge di bilancio e non soltanto. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Tutto si tiene e l'insieme non è un granché. Lasciate che lo dica. Tutto ciò che vediamo non fa che incrementare la nostra preoccupazione. Vorrei concludere dicendo anzitutto che non sentivamo la necessità di di veder costruire il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato di arbitrio e invece questo vediamo avvenire: il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato di arbitrio. Attraverso la Presidenza mi pare inoltre sia necessario concludere questo intervento - uno dei tanti che il Partito Democratico stasera ha svolto in quest'Aula con alcune domande che vorrei porre, soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, conoscendone la storia, e le affermazioni passate. La prima cosa che vorrei chiedere loro è: ma che cosa siete diventati? che cosa siete diventati? Eravate il partito del no ad ogni immunità e passerete alla storia come il partito che ha favorito l'immunità più scandalosa di tutte. Eravate il partito dell'onestà e passerete alla storia come il partito della complicità. Salvando Salvini perderete ogni credibilità: perderete ogni credibilità: perché lo farete contro la legge per le ragioni che ho detto, perché lo farete contro l'evidenza dei fatti, perché lo farete - ne sono sicuro - in molti casi anche contro la vostra coscienza, perché lo farete per salvaguardare un patto di potere e una spartizione di potere che non ha niente di nobile e che ha molto di immorale. Fermatevi perché siete ancora in tempo a fare la cosa giusta. Termino il mio intervento augurandomi che domani, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle (lo dico sempre tramite lei, Presidente) quando voterete, mi auguro che lo farete obbedendo alla vostra coscienza, lo farete in libertà, lo farete ricordandovi tutto quello che avete detto e che rischia di venir cancellato

l'argomento di questa discussione sia cosa decidere di fare con la serenità con cui lo può decidere un Senato della Repubblica: valutare che non c'è alcuna ragione per un trattamento speciale verso un cittadino italiano, che peraltro ha rivendicato con totale convinzione le proprie azioni, che probabilmente - ma questo lo valuterà la magistratura sono criminose rispetto all'attuale normativa italiana. Da garantista, sono convinto che chiunque sia innocente fino a condanna definitiva e ritengo giusto dare a questo cittadino italiano la possibilità di dimostrare la propria innocenza oppure, più probabilmente - come egli stesso ha chiesto - la sua volontà palese di violare la normativa perché le proprie convinzioni politiche lo portano a dire che è sbagliata. Certo, pensiamo che chi dispone di una maggioranza di Governo e ritiene che una normativa sia sbagliata farebbe meglio a modificarla e comportarsi nel rispetto della legge, però è una rivendicazione che egli ha fatto. quindi perché quest'Assemblea debba creare uno scudo. Che non ci fosse un interesse prevalente è stato argomentato in maniera molto significativa, non solo nelle relazioni, ma nei numerosi interventi

dell'arbitrio, non del libero arbitrio, ma di quello del potere. Tutta la civiltà giuridica che abbiamo costruito è nata, facendoci uscire dal periodo feudale e poi da quello delle monarchie assolute, sulla base dello Stato di diritto come elemento che tutela il cittadino dal potere.

Quello che stiamo valicando in queste ore è un limite, per cui domani mattina qualcuno potrebbe svegliarsi e dire che nell'interesse prevalente del Paese è possibile portare via la casa a un altro, che non potrà dire niente, perché è nell'interesse prevalente del Paese. Ognuno di noi

in un porto, sul territorio nazionale, e c'era il presidio della forza pubblica: quale era il problema? Il problema c'era ed è dovuto alla trasformazione che sta avendo la nostra democrazia, purtroppo insieme a molte altre: noi stiamo passando dalla democrazia alla demagogia e in questa contano di più i simboli, o meglio le urla, o meglio le dichiarazioni fascinose, affascinanti e coinvolgenti che toccano l'emotività delle persone rispetto alle azioni concrete e ai fatti. Per cui, se un Ministro dell'interno vuole mettere in campo delle azioni utili a governare il fenomeno dell'immigrazione non ha bisogno di fare ciò che fa il nostro attuale Ministro dell'interno; se, invece, siamo nell'era della demagogia, allora abbiamo bisogno di alzare i toni, di inventare nemici, di costruire criminali e di dimostrarci eroi che combattono contro il drago che non c'è, inventandosene uno per darlo in pasto ai cittadini e diventare eroi. Nel tempo della demagogia l'interesse prevalente che voi state provando a tutelare è il diritto alla propaganda

di chi si occupa di politica, riconosce il loro lavoro e si fa carico anche delle loro responsabilità, rischiano di essere messi nella condizione di avere indicazioni politiche che vanno contro il loro dovere di pubblici ufficiali e il loro dovere nei confronti delle leggi. Il paradosso è che poi, se si ipotizza che questa persona sia un possibile portatore di una violazione della norma, a lui non costa niente mettere gli altri contro la norma perché per lui viene alzato dalle persone che che sono contrattualmente vincolate a quel patto tra due capi uno scudo che li difende. Tutte queste questioni davvero meriterebbero una riflessione individuale di ogni singolo senatore e di ogni singola senatrice perché non si tornerà indietro

alcune ore di riflessione e una pausa. Qualcuno dice che la notte porta consiglio. Io vorrei che domani avvenisse un fatto sorprendente: che ci svegliassimo con un con un Senato che ritrova il suo coraggio, la sua libertà, la sua dignità e in cui ogni senatore e senatrice porti il proprio valore dentro questa Aula - come fa ogni giorno - e che questo Senato si sentisse liberato e senza nessuna minaccia. Non succederà niente al Governo; non succederà niente alla maggioranza e non succederà niente neanche al cittadino cui permetteremo di fare ciò che ci ha chiesto di fare: sfidare il drago; andare di fronte ai giudici e dimostrare la sua innocenza o la sua volontaria colpevolezza. Diamogli questa possibilità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro presente-assente, è doveroso eliminare ogni equivoco da questo dibattito, ogni pretesto che possa essere usato per alimentare uno scontro nel merito dei fatti avvenuti a bordo della nave Diciotti. Il Senato non deciderà se il ministro Salvini ha commesso un reato abusando dei suoi poteri, trattenendo indebitamente a lungo profughi e marinai del pattugliatore della Guardia costiera; il Senato deciderà invece se il ministro Salvini avrà la libertà di difendersi dalle accuse che gli ha mosso il tribunale di Agrigento motivando le ragioni per cui ha ritenuto di non archiviare ma, anzi, rinviare gli atti al Parlamento per la sua valutazione. Il Senato deciderà anche se le ragioni della politica, dei partiti e della tenuta del Governo sono più forti della legge e del diritto che ogni uomo ha di difendersi nel processo. Lo stesso ministro Salvini si era fatto forte di quel diritto quando, appena ricevuto l'avviso di garanzia, aveva detto di essere pronto ad andare dai magistrati addirittura il giorno dopo: «Mi costituisco», aveva detto a caldo il Ministro. Ma qualcosa è rapidamente cambiato e Salvini ha deciso che bisognava difendersi dal processo, dai magistrati che non sono stati eletti da nessuno. Non credevo che avremmo assistito a una replica sbiadita di quello scontro tra politica e magistratura che ha segnato una stagione certamente poco edificante della nostra storia recente. Per noi, nemmeno un Ministro è al di sopra della legge. Per noi, che pure crediamo sia stata compiuta una violazione grave, un abuso di potere, tocca alla magistratura ordinaria vagliare la legittimità delle decisioni del Ministro dell'interno. Non tocca a noi sostituirci alla magistratura e dichiarare prosciolto Salvini. Pensavamo che questa fosse anche la convinzione che animava quel Movimento portato in quest'Aula da un'onda popolare che gli chiedeva di farsi portavoce di istanze di giustizia e pulizia nelle istituzioni. Ci ingannavamo, al pari di milioni di cittadini che mai avrebbero creduto di vedere il partito fondato da Beppe Grillo ricorrere ai metodi del tanto vituperato Berlusconi. È tardi, ma è bene ricordare ancora ciò che è successo. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2018, la nave della Guardia costiera italiana Diciotti salvò 190 migranti nella SAR maltese. Per cinque giorni la nave rimase al largo di Lampedusa, mentre il ministro Salvini polemizzava con Malta e altri Paesi europei circa la distribuzione dei naufraghi e minacciava un respingimento verso la Libia. Da lì a poco vennero sbarcati d'urgenza solo 13 migranti in gravi condizioni di salute. Il 20 agosto - ed erano passati già cinque giorni - il ministro Toninelli indicò Catania quale porto d'attracco, ma Salvini negò l'autorizzazione allo sbarco, continuando a polemizzare con gli altri Paesi affinché si facessero carico dell'accoglienza dei migranti salvati. La nave Diciotti rimase quindi ancora nel porto di Catania con 177 persone a bordo. Il 22 agosto sbarcarono 29 minorenni non accompagnati. Gli altri furono fatti sbarcare nella notte tra il 25 e 26 agosto: undici giorni dopo. Per undici giorni un numeroso gruppo di migranti fu trattenuto a bordo; fu negata loro qualsiasi assistenza sanitaria e sociale, impedito di presentare domande per l'accoglienza. Per tutto questo la procura di Agrigento ha ritenuto di indagare il ministro Salvini per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Ora, come prevede la Costituzione, questa Camera può negare l'autorizzazione, con delibera a maggioranza assoluta, «ove» - voglio citarlo ancora - «l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante». Il presidente emerito della Corte costituzionale, Valerio Onida, ha scritto come, nel nostro caso, venga affidata esclusivamente all'Assemblea parlamentare una valutazione per cui, anche se il fatto in sé costituisce reato, essa ritenga «l'agire del Ministro giustificato dalla prevalenza dell'interesse pubblico e quindi lo sottragga sottragga alle normali conseguenze processuali e sanzionatorie». Noi tutti siamo dunque chiamati a concedere all'autorità giudiziaria competente l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro, ma la legge costituzionale del 1989 prevede pure che, a maggioranza assoluta, la Camera di appartenenza possa anche negarla, ove ritenga che l'inquisito abbia agito nel rispetto della citata norma costituzionale. L'ho ricordato: il ministro Salvini, sin da subito, dichiarava di voler affrontare a viso aperto e senza *escamotage* il processo. Oggi però il Ministro, che non ha paura di nessuno, vuole farsi scudo della norma costituzionale e invoca a sua difesa lo schieramento incondizionato di tutti i senatori della Lega e di quelli del MoVimento 5 Stelle. Quali siano gli equilibri interni alla maggioranza non è dato e neanche ci interessa sapere. Del resto, lo si è letto nelle agenzie quale sia stato l'ordine dato ai senatori del MoVimento 5 Stelle, che siedono qui privati della libertà di votare secondo la propria coscienza. La nostra è una posizione diversa, perciò facciamo un appello al ministro Salvini affinché si sottoponga, come ogni cittadino che si rispetti, al giudizio della magistratura ordinaria. Se verrà condannato in via definitiva, vorrà dire che non avrà impedito lo sbarco per ragioni di sicurezza, comprimendo le libertà fondamentali dei migranti non per un motivo lecito, ma per ragioni politiche. Non dobbiamo però essere noi a stabilire questo, chiediamo che lo stabilisca un tribunale dello Stato. Noi vorremmo che fosse qui ribadito senza esitazione che la legge vale per tutti, Salvini compreso. Mi sia permesso aggiungere un pensiero che spero potrà essere condiviso o almeno preso in considerazione al di là dei nostri schieramenti: ci troviamo in quest'Aula, che costituisce uno dei luoghi sacri della nostra democrazia, dove ogni cosa ci ricorda i nostri doveri, a riflettere su una questione che prescinde nella sua essenza da ogni valenza politica e andrebbe intesa *in primis* come tema etico, perché quando chiunque di noi, membro eletto di quest'Aula o semplice cittadino, non considera più quale bene supremo il rispetto dell'uomo e la vita dei suoi simili, in quel momento dobbiamo fermarci. Se tutto ciò non riesce più a scuotere le nostre coscienze, significa non soltanto che abbiamo abiurato a quell'imperativo categorico che determina la nostra umanità, ma che ci siamo anche lasciati alle spalle secoli di progresso sulla strada dei diritti

*(PD)*. Signor Presidente, oggi il Senato è chiamato a esprimersi su una vicenda che non ha precedenti nella storia repubblicana. Al cosiddetto *festival* dello scambio all'interno della maggioranza domani si salva il ministro Salvini e giovedì si fa lo scambio salvando magari il ministro Toninelli.

e a tutto il Governo che è responsabile di aver privato 177 persone della loro libertà e dignità, violando la nostra Costituzione e le convenzioni internazionali: vi chiediamo di farvi un esame di coscienza guardare al clima di odio e di paura che avete creato nel Paese. Purtroppo lo vediamo drammaticamente nella cronaca quotidiana. Noi vogliamo ripristinare la vigenza del diritto e dell'umanità, la legalità costituzionale e i diritti umani che il Governo ogni giorno sta violando. Per la prima volta nella storia repubblicana l'interesse della coalizione di maggioranza all'attuazione di una linea politica viene fatta coincidere con il preminente interesse pubblico, cioè con una ragione di Stato o di Governo che nello Stato democratico di diritto non può essere fine a se stessa. Il voto di oggi ha dunque per oggetto non una vicenda giudiziaria, che pure è rilevante, ma una visione stessa dello Stato perché questo è un atto politico vero e proprio, un atto di Governo, di maggioranza che in quanto tale dovrebbe prevalere - secondo voi - sull'interesse pubblico. Questa nozione di atto pubblico è stata però - come abbiamo visto già in altre occasioni, e pensiamo alle leggi razziali - esclusa dal Consiglio di Stato. Allora ci chiediamo: per poter giustificare un'azione simile, come dice il nostro patrimonio giuridico comune nello Stato di diritto - e ancora fortunatamente lo siamo ci devono essere gravi motivi di sicurezza nazionale, di pericolo reale per l'integrità dello Stato, per la vita e l'incolumità delle persone e per i diritti costituzionali fondamentali dei cittadini. Ma, come sappiamo dagli atti fin qui depositati, si fa riferimento, oltre che alla domanda di autorizzazione del tribunale di Catania, alla memoria presentata dal Ministro dell'interno alla Giunta delle elezioni e condivisa dal Presidente del Consiglio e dal Governo, da cui emerge, però, che non c'è alcun pericolo del genere. Il tribunale di Catania scrive non si comprende quale potrebbe essere l'interesse pubblico qualificato, cioè riconosciuto e tutelato come tale da norme di legge. La relazione mette in evidenza che non sussistono pericoli per il nostro Paese, dato che è stato accertato che a bordo della nave non vi erano soggetti sospettati di costituire un pericolo per tali fondamentali valori, gli unici che avrebbero potuto consentire l'invocazione all'articolo 52 della Costituzione, e cioè la difesa della Patria, mentre sì la libertà personale e la dignità dei migranti costituiscono diritti fondamentali della persona, riconosciuti come valori inviolabili della nostra Costituzione, rispetto sia ai cittadini italiani che a ogni altra persona di qualsiasi nazionalità. Sono inoltre riconosciuti come valori inderogabili da principi e regole internazionali che il nostro Paese ha sempre condiviso. Per tutte queste ragioni, la decisione che domani prenderete qui al Senato avrà un rilievo istituzionale e non semplicemente politico e avrà cioè delle conseguenze, oltre a creare un precedente, che andrà a limitare di fatto la libertà personale e, quindi, i diritti inviolabili di ogni cittadino. Chiedetevi allora cosa state facendo - avete questa notte per pensarci quale precedente si verrà a creare dopo questo voto assurdo che domani quest'Aula forse esprimerà. Pensiamo a cosa vuol dire Mediterraneo; pensiamo a cosa vuol dire parlare di una civiltà civiltà millenaria come la nostra, fatta di accoglienza, ospitalità, umanità, solidarietà. Sono parole sconosciute a questo Governo, che già parecchie volte si è venduto in uno scambio di favori reciproci. Noi non ci stiamo. Noi difendiamo i diritti e la libertà individuale, difendiamo ogni essere umano perché questo è uno Stato di diritto.

Signor Presidente, spiace anche a quest'ora dover iniziare l'ennesimo intervento nella perdurante assenza...

Le volevo dire che spiace iniziare l'intervento nella perdurante assenza del ministro Salvini che, pure se preso probabilmente da qualche sua presenza televisiva, ci auguravamo che a un certo punto si rendesse conto non

È lei, collega? Non lo avevo capito. Prego, prosegua, non è un'offesa al Partito Democratico. Non è ostentare arroganza e presunzione nei confronti del Partito Democratico. È ostentare un'arroganza e una mancanza di rispetto nei confronti di quel Parlamento in nome del quale e grazie alla fiducia del quale siede nei banchi del Governo. Governo. Vorrei partire da questo. Nella valutazione che il Senato è chiamato a esprimere oggi si incrociano ragioni e profili diversi, alcuni di carattere giuridico in senso stretto, altri invece di carattere più propriamente politico. C'è una cosa, però, che senza alcun dubbio a quest'Aula non compete, come hanno detto tanti colleghi prima di me: la valutazione sulla colpevolezza o l'innocenza di un cittadino italiano, che resta - ricorderei - per fortuna nelle mani di una magistratura indipendente e autonoma, anche se il cittadino in questione è il Ministro dell'interno in carica e *leader* di questo Governo e della maggioranza. Non è nostro compito entrare nel merito dell'accusa. Non spetta a noi giudicare la sua fondatezza o meno; tanto meno stiamo qui oggi valutando se quell'accusa sia stata sollevata in maniera artificiosa, se sia riscontrabile, cioè, un *fumus persecutionis*. C'entra poco anche l'immunità parlamentare da qualcuno evocata. Non c'entra, perché oggi dobbiamo valutare, anche qualora il fatto costituisca reato, se l'agire del Ministro sia stato giustificato dal prevalere di un interesse pubblico. Non siamo di fronte a una valutazione schiettamente politica; dobbiamo basarci su principi giuridici, che in un sistema costituzionale e democratico non sono mai nella piena discrezione esclusivamente della politica. Ecco perché non ci può bastare oggi il profilo soggettivo, cioè il fatto che il ministro Salvini, da parte sua, abbia dichiarato che, nel negare lo sbarco, vi fosse un preminente interesse pubblico. Tutti abbiamo letto con attenzione le parole che il ministro Salvini ha inviato, il 29 gennaio, al «Corriere della Sera», scrivendo che egli ha agito al fine di verificare la possibilità di un'equa ripartizione tra i Paesi dell'Unione europea degli immigrati a bordo della nave Diciotti. Con quelle parole, però, il ministro Salvini ammette più di quello che dice: rivela di considerare il contenuto di una sua promessa elettorale ben al di sopra e ben più importante di ciò che è consentito dalla legge, dal diritto del mare e dal diritto internazionale. Noi siamo in presenza di un Ministro dell'interno che sostanzialmente considera - come pure è stato già detto - la sua funzione di Ministro come un mandato del popolo, che lo pone al di sopra della legge e gli permetterebbe di piegare a proprio esclusivo piacimento interessi che hanno di per sé un valore superiore - quelli sì a partire dal rispetto dei diritti umani fondamentali, tra cui appunto quello alla libertà personale, che non possono mai - dico, mai - essere nella libera e assoluta disponibilità del potere politico. Tutto questo non solo è inaccettabile per chi ha un minimo di cura per la difesa del nostro Stato di diritto e dei suoi principi democratici e di garanzia; tutto questo è anche lontanissimo dal rendere il comportamento tenuto dal Ministro un atteggiamento accettabile alla luce del più volte richiamato interesse pubblico preminente. Volete poi farci credere che la politica del Governo sull'immigrazione sia stata una politica univoca, lineare; ma noi vi abbiamo dimostrato che non è così. Soltanto un mese prima, nel luglio 2018, tutti ricordiamo che un caso simile a quello della Diciotti terminò soltanto quando il Presidente del Consiglio ordinò lo sbarco. In quel frangente il Ministro dell'interno dichiarò esplicitamente che non condivideva le decisioni adottate dal Presidente del Consiglio; situazione che si è ripetuta con il caso Diciotti, quando il Ministro dell'interno ha minacciato una crisi di Governo, nel caso in cui la sua linea politica fosse stata sconfessata dal Presidente del Consiglio. Iniziamo a dire, quindi, che in quei giorni ci sono state iniziative assunte singolarmente dal Ministro dell'interno, in dissenso da altri membri del Governo. Altro che indirizzo governativo condiviso e coordinato! Il punto vero è che, quando è in gioco un interesse pubblico, anche l'indirizzo governativo che lo persegue dovrebbe essere improntato alla serietà, alla coerenza e alla responsabilità. Invece questi sono tutti elementi che sono mancati nelle politiche degli ultimi mesi, in modo particolare in quelle sull'immigrazione, e lo sono stati in modo palese nel caso della In quell'occasione è mancata un'iniziativa politica seria, che utilizzasse gli strumenti della concertazione e non quelli della minaccia. È mancata la diplomazia, che sarebbe stato necessario avviare, se vi fosse stata realmente una controversia internazionale tra l'Italia e lo Stato maltese. È mancata, infine, soprattutto la credibilità gli altri Paesi europei, che questo Governo ha iniziato a perdere quando il Gruppo di Visegrád, amatissimo dal nostro Governo, ci ha messo nell'angolo proprio sul tema dell'immigrazione. Quando si è trattato di modificare, su proposta del Parlamento europeo, la regola del primo ingresso, sostituendola con un meccanismo obbligatorio di ripartizione dei richiedenti asilo, le forze che reggono questo Governo sono scomparse o si sono astenute o addirittura hanno votato contro. contro. È paradossale, a proposito di indirizzo del Governo, perché, così facendo, in pratica hanno votato contro quello che loro stessi avevano scritto nel famigerato contratto di Governo. Fatemi dire che è inevitabile che vada così, perché quando usi una logica nazionalista è chiaro che, poi, alla fine, ti scontri con interessi inconciliabili, confine contro confine, e anziché suonarle agli altri - come dice di fare il nostro Governo - finisci per essere suonato tu. Allora, quando non sei più credibile con i tuoi *partner,* ti rimane soltanto l'appiglio della propaganda e degli annunci vuoti, in cui il ministro Salvini ha dimostrato eccellere in questi mesi. a cominciare dal tentativo di confondere la lotta contro l'immigrazione clandestina con il salvataggio in mare di naufraghi, che ha regole e obblighi ben precisi, a partire da quello di identificare, appunto, il porto di sbarco. Mentre discutiamo, un'altra nave - la Mare Jonio - è rimasta bloccata dall'Italia fuori dal porto di Lampedusa con 49 migranti a bordo. Si tratta di persone che, dopo aver subito torture e ricevuto botte, stanno scappando dalle prigioni libiche, mettendo in pericolo la vita pur di non tornare in quell'inferno. E il Ministro dell'interno italiano ha avuto la faccia tosta di invitarle a sbarcare nei porti libici, che - secondo lui - sono adeguati a offrire assistenza logistica e sanitaria. Cari colleghi, se non fosse drammatica, questa situazione sembrerebbe perfino poco Gli atti compiuti nell'agosto scorso dal ministro Salvini non lasciano dubbi. L'ordine di non far sbarcare i naufraghi è stato emesso per fare pressione sugli Stati dell'Unione europea. Un Governo serio si sarebbe attivato per cambiare le regole comuni con mezzi leciti. Il nostro Ministro ha invece preferito il ricatto verso i Paesi membri, trasgredendo regole e obblighi del diritto internazionale e interno e il Governo tutto gli è andato dietro, perché non ha trovato la forza politica per fermarlo. Quanto accaduto nell'agosto del 2018 sta lì a dimostrare una cosa semplice: il sovranismo a giorni alterni di questo Governo, che un giorno rivendica prerogative

ma non può produrre un indirizzo politico di Governo coerente e capace di perseguire un obiettivo. Altro che interesse pubblico: quello andato in scena nell'agosto scorso è solo una vergognosa azione di propaganda irresponsabile che il nostro Ministro dell'interno ha fatto pagare a uomini, donne e minori, che, per vedere migliorata la propria vita, avevano corso il rischio di poterla perdere e che, invece, si sono visti limitare, senza alcuna giustificazione, i propri diritti. Su quella nave non c'erano terroristi, né persone che avrebbero potuto mettere in pericolo l'incolumità pubblica; c'erano 177 persone disperate, tra cui minori non accompagnati e donne che fino a pochi giorni prima avevano subito violenza. Si tratta di persone che sono state strumentalizzate in maniera vergognosa. È per questo motivo che il ministro Salvini non può oggi opporre lo scudo che gli viene dalla sua attività di Ministro e deve poter essere giudicato da una magistratura competente e autonoma che, in piena e assoluta libertà, in ogni Stato democratico e giusto sarebbe chiamata a valutare il suo operato.

Signor Presidente, le vicende da cui scaturiscono le accuse pesantissime al ministro Salvini sono state impresse nella nostra memoria collettiva innumerevoli volte, troppe volte - voglio dire insopportabilmente troppe volte - per l'Italia, l'Europa e le nostre democrazie.

dalle convenzioni internazionali, dalla Costituzione e dalle leggi italiane, di essere tratti in salvo e condotti in un porto sicuro. Questo, invece, non è avvenuto in quei cinque lunghissimi giorni, tra il 20 e il 25 agosto in cui è stato impedito lo sbarco e il nostro Stato di diritto è stato sospeso, come dice il tribunale di Catania. Ciò è avvenuto per le 190 persone della nave Diciotti,

da dove stanno scappando. Non ce lo chiediamo mai e questo è un errore, un torto. Dobbiamo dire a voce alta, per onestà intellettuale e politica, che scappano da guerre e persecuzioni, come siamo scappati noi decenni addietro. Scappano da violenze indicibili, come quelle dei campi libici, che anzi dovremmo chiamare *lager*, dove c'è un'immane barbarie che si sta consumando e non possiamo far finta di nulla. Vanno stracciati gli accordi con la Libia. Va messa in piedi invece una missione di pace internazionale, che intervenga. Va ripresa l'attività di salvataggio nel Mediterraneo: l'indifferenza del Governo italiano è una voragine morale e politica. Il fatto che si agiti ossessivamente il tema dell'invasione è qualcosa di falso, una grande arma di distrazione di massa,

per nascondere il vuoto pneumatico sul lavoro e sull'economia, la disoccupazione che cresce e la recessione che dissangua il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*. L'Italia è un grande Paese, non merita questa vergogna e che si tengano in ostaggio persone inermi, per essere utilizzate a un tavolo di contrattazione europea. In Europa si conta per l'autorevolezza e quale autorevolezza può avere un Paese il cui vice Presidente è accusato di sequestro di persona, di abuso di ufficio e di omissione di soccorso? *(Applausi della senatrice altri ordinamenti porterebbero all'alto tradimento e all'*impeachment*. Per noi la vita umana e il rispetto della persona vengono prima di ogni calcolo elettorale, perché qui vive o muore la nostra democrazia. Dunque, non può esserci alcuna scelta politica che violi le leggi e, in questo caso, la libertà personale, che è garantita dalla Costituzione. Può questa Assemblea, signor Presidente, avallare la violazione massiccia dei diritti umani? Signor Presidente, colleghi, non possiamo, perché la nostra Costituzione figlia della Resistenza e i nostri Padri costituenti allora giurarono che non ci sarebbe stata mai più violazione dei diritti e mai più sospensione dello Stato di diritto, come era avvenuto durante il fascismo. «Difendere i diritti dei migranti significa anzitutto difendere tutti noi», ha scritto Luigi Ferrajoli ed è vero. Aggiungo che ciò significa non far arretrare i diritti degli italiani, soprattutto quelli dei più deboli tra noi. colleghi, impedendo alla magistratura di andare avanti e negando l'autorizzazione a procedere, date un colpo allo Stato di diritto e affermate che quello della politica è un potere assoluto, arbitrario e sopra la legge. Allora chiedo: se domani, anziché contro i migranti, questo potere venisse usato contro la libertà di stampa, che peraltro mai come adesso è minacciata dai vostri tagli e dalle vostre politiche, o contro le minoranze? Vi ricorda qualcosa tutto questo? Il voto su Salvini è un punto di non ritorno; uno sfregio all'equilibrio dei poteri; una minaccia a quella libertà di ogni cittadino, che è inviolabile, come quella dei 177 della nave Diciotti.

senatore che giorni fa, riferito ai parlamentari di opposizione, fece il gesto delle manette: un gesto abietto. Egli, intervistato dal «Corriere della Sera», a proposito del salvataggio di Salvini, ha detto che il Ministro dell'interno «deve essere libero libero di agire in nome e per conto dello Stato». C'è qualcosa di più inquietante e pericoloso di una frase del genere? Nessun Ministro o Capo di Governo può essere libero di agire per conto dello Stato, perché abbiamo una Costituzione e delle leggi, a garanzia dei diritti democratici di tutti, che tutti devono rispettare. I rappresentanti del Governo per primi hanno l'obbligo di farlo e anche Salvini ha quest'obbligo; quel Salvini che, qualche tempo fa, all'inizio di questa vicenda diceva: «Fatemi processare!» Lo diceva nei comizi, urlando. Quando invece poi la richiesta è arrivata, forte e motivata, è scappato dal processo. chi scappa lo fa per paura, signor Presidente, e allora il ministro Salvini ha deciso di essere salvato dal processo a ogni costo e i 5 Stelle hanno deciso di salvare Salvini. Pur di restare al potere non hanno problemi - lo stanno dimostrando - a vendersi l'anima. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Hanno urlato per anni nessuna immunità per nessuno, ma era propaganda, era presa in giro. Per un briciolo di potere, per qualche ufficio ministeriale, la prospettiva può cambiare e allora possono votare a favore delle immunità perché, se cade Salvini, vanno tutti a casa e quindi dicono sì all'immunità e no ai giudici. Allora si mette in piedi la pantomima della consultazione *on line* per giustificare il tradimento delle loro posizioni; una consultazione gestita da Casaleggio, sulla piattaforma *on line* di Casaleggio,

come due facce della stessa pessima moneta. Gridavate contro il potere; oggi insabbiate le accuse di abuso di potere e sequestro di persona rivolte a voi,

per l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, perché non c'è alcuna difesa degli interessi dello Stato nel tenere in ostaggio persone inermi, violando il principio di legalità, che è il cuore degli Stati democratici, solo per ragioni politiche, propagandistiche, elettoralistiche. è una pagina nera. Domani non potrete dire di non sapere. Noi non saremo complici; continueremo a parlare e a denunciare a voce alta; risveglieremo quelle coscienze che da troppo tempo state ingannando, ma che non potrete ingannare ancora. *(Applausi